donne; la decisione di revisionare le Province mediante un disegno di legge costituzionale di

queste sì definite, e nella loro entità e nella loro qualità, nel senso che sono entrate di competenza e di cassa, addirittura con scadenze precise. Dunque, i requisiti sono esattamente quelli che la pressione di questi giorni ci chiede,

forse contribuirebbero di più ad un clima di serenità, che è necessario per la considerazione dell'Italia all'estero. In quella Commissione, maggioranza e opposizione, mantenendo ovviamente i toni critici che differenziano il giudizio complessivo sulla legge finanziaria, hanno discusso approfonditamente, con estrema serietà e - lo dico per tutti gli altri membri della Commissione - con grande competenza la materia che avevano di fronte.

italiana: un Governo che, assumendo la specificità della crisi italiana all'interno della crisi internazionale, ha saputo provvedere in tempi certi. Dall'altra, un Parlamento che nel suo complesso, e con grande senso di responsabilità,

e dell'intero Parlamento, maggioranza e opposizione. Forse un giorno bisognerà rendere pubbliche anche le sedute delle Commissioni così da far conoscere i toni, la qualità dei parlamentari

parlamentari e a tutti coloro che in questi giorni in Commissione ed in Aula hanno lavorato per fronteggiare la più grave crisi finanziaria a memoria di vivente. Signor Presidente, non intendo replicare, perché sui documenti noti

che con grande senso di responsabilità ha saputo dare corso a tante modifiche migliorative del testo originario, testo ulteriormente rafforzato dalle ultime misure adottate dal Governo con il maxiemendamento che di qui a pochi minuti

e di lavorare per l'Italia in un momento così difficile, accogliendo in pieno sia l'appello del Capo dello Stato

A nome del Governo lo voglio ringraziare pubblicamente, perché con la sua proverbiale saggezza ha saputo dare corso a lavori che hanno subito modifiche

*(IdV)*. Non voglio turbare questo clima di falso ecumenismo da cui intendo sottrarmi.

Le chiedo, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, se abbiamo ancora tre carte, se c'è qualche carta coperta o scoperta: vorremmo capire i tempi che noi abbiamo. leggiamo - il senatore Morando ne aveva fatto menzione - che il maxiemendamento sarebbe stato depositato ieri sera o nel corso della notte, mentre il sottosegretario Gentile

il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo

Presidente, le chiedo di verificare che, assieme all'emendamento, venga depositata anche la relazione tecnica, come richiesto dal nostro Regolamento.

Onorevoli colleghi, l'emendamento interamente sostitutivo, presentato dal Governo, è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente. Il Presidente della Commissione riferirà all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria alle ore 12. Avrà quindi inizio la discussione sulla questione di fiducia, che potrà protrarsi fino alle ore 18, momento in cui avranno inizio le dichiarazioni di voto finali con trasmissione diretta televisiva. Pertanto, la chiama sul voto di fiducia sarà indetta intorno alle ore 19. Conseguentemente, sono sconvocate le sedute già previste dal calendario per giovedì 8 e venerdì 9 settembre, fatta salva la riunione del Parlamento in seduta comune domani mattina, alle ore 10. **Calendario

associati effetti finanziari e quindi noi le segnaliamo affinché quegli effetti abbiano una rispondenza nel merito del testo normativo proposto. Se è possibile occorre

è stata richiesta la corrispondenza tra questa norma e quella precedente che impone alle Regioni l'obbligo di assicurare con addizionali proprie fondi per gli eventi calamitosi e solo a seguito dell'espletamento di questi compiti la possibilità di intervento dello Stato centrale. Il Governo ha risposto che

si meravigliava del fatto che a due platee differenti fossero associate misure di esatta corrispondenza. Questa era l'annotazione che veniva fatta.

ai fornitori della pubblica amministrazione. La risposta del Governo è stata politica: il Governo non ha ritenuto di porlo nell'emendamento su cui ha posto la fiducia. Questa è stata una risposta molta chiara, non naturalmente, signor Presidente, nel merito, che non tocca a me assolutamente valutare. È stata una risposta precisa: il Governo ha ritenuto di non doverlo inserire nel testo su cui pone la fiducia. la questione di rilievo finanziario maggiore. Alcuni senatori hanno posto questo problema specifico. È evidentissimo il miglioramento dei saldi conseguente, in particolare, nella sua parte assolutamente maggioritaria, all'aumento di un punto dell'aliquota IVA ordinaria. Di fatto, i saldi migliorano dell'entità di quella maggiore entrata più piccolissime cifre. Nessuno ha fatto correttamente questioni sulla qualità di quella entrata, che è perfettamente identica a ciò che ha sostituito, perché ha lo stesso carattere di certezza e di liquidità. I senatori però hanno posto un problema di destinazione di quel miglioramento dei saldi; in particolare, uno fa riferimento alle necessità che avremo con la delega, che chiamo chiamo genericamente assistenziale e fiscale, ma che tutti sappiamo qual è. Si riteneva da parte di alcuni senatori che una destinazione di quel miglioramento del saldo a copertura di quella delega contribuisse alla solidità dell'impianto della manovra;

del saldo maggiore quanto nel verificare la solidità dell'impianto della manovra e, quindi, la destinazione di quel miglioramento del saldo immediatamente al consolidamento di entrate

la destinazione di quei saldi, così come è stata proposta, lascia comprese anche le destinazioni che vengono proposte.

essere certo il conseguimento del pareggio di bilancio nel 2013 come imposto e, quindi, una riserva di maggior saldo serve a conferire uguale certezza

Governo il suo parere sulla necessaria certezza e solidità dell'impianto complessivo della manovra come il carattere più importante per per fronteggiare le pressioni dei mercati finanziari in questi giorni.

destinazione più efficace del maggior saldo attivo - chiamiamolo così - conseguito con questa manovra. A me interessa molto, signor Presidente, ribadire questi concetti: come ho detto più volte nella relazione, la manovra è stata affrontata da tutti i colleghi della Commissione in uno spirito di assoluta costruttività

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

Signor Presidente, nella storia di un Paese ci sono dei momenti in cui non è permesso temporeggiare o rinviare

di un uomo stanco e amareggiato, che non riesce a fronteggiare una situazione figlia, in gran parte, degli errori commessi da lui e dal suo Governo e, per questo, non più in grado di guidare il Paese. Errori, dicevo: dapprima la manovra di luglio, che rinviava gli aggiustamenti alla prossima legislatura, poi una manovra integrativa caratterizzata dall'assenza di un messaggio chiaro. Norme confusamente affastellate, approssimativamente predisposte, sbagliate tecnicamente, modificate o ritirate a poche ore dalla presentazione, fino a questa mattina. II Governo stesso ha dimostrato di non credere in ciò che sta facendo. II problema nostro è soprattutto un problema di credibilità. Si è affermata nell'opinione pubblica internazionale, quella più diplomatica delle Cancellerie, almeno nel luogo pubblico, e quella più impietosa dei mercati, l'idea che l'Italia non possa farcela con una crescita troppo bassa e con un debito così elevato, e soprattutto che la maggioranza politica che guida il Governo non ne sia consapevole, e per questo siamo puniti dai mercati. Avete fatto di tutto per confermare tale pregiudizio. Dopo la famosa lettera Trichet-Draghi avete preso degli impegni, di fronte all'opinione pubblica e di fronte alle autorità finanziarie e politiche europee, e non li avete onorati, preoccupati più delle reazioni immediate di interessi parziali inevitabilmente toccati che della direzione di marcia del risanamento. Si parla molto di costi della politica, colleghi, ma non c'è costo più elevato di una politica che viene meno al dovere della fermezza e della coerenza. Bisogna rimediare. Proprio la vicenda greca dimostra che ciò che non si vuole fare oggi si è costretti a fare domani con un costo molto più elevato ed un effetto molto più debole. Le correzioni ora introdotte vanno anche nella direzione giusta per rafforzare coperture inesistenti, ma non rimediano all'insufficienza strutturale della manovra: manovra sbagliata, peggiorata ad Arcore, ora comunque inferiore alle necessità. bisognava ristabilire due pilastri ben piantati che reggono tutta l'ossatura e a cui abbiamo conformato le nostre proposte. Il primo è quello dell'equità. Se bisogna chiedere dei sacrifici, occorre che siano ripartiti secondo le possibilità con un principio di giustizia. Ed è la così evidente violazione di questo principio (che è etico, prima ancora che politico) a rendere la manovra insostenibile. La pretesa che chi chi più ha non sia chiamato in nulla a contribuire al risanamento e che gli altri debbano pagare in silenzio. Il Capogruppo della Lega ieri ha criticato il Partito Democratico per la presenza di propri dirigenti ai cortei della CGIL invece di essere in Senato. Oggi il senatore Bricolo, mentre si discute di una manovra che influisce sulle condizioni di vita di tutti gli italiani, non è presente. *Gramazio)*. Ma in piazza non c'erano pericolosi criminali. C'erano tanti cittadini italiani che hanno manifestato pacificamente contro l'iniquità della manovra. Il senatore Bricolo ricorderà con quale impegno ed attiva partecipazione i parlamentari della Lega sostenessero gli evasori delle quote latte mentre sparavano letame contro la polizia. siamo andati da un'altra parte. E, se permettete, i nostri dirigenti non frequentano, con una costanza degna di migliori interlocutori, malavitosi ricattatori, come tale Lavitola, di cui si occupano le cronache. Il secondo pilastro è la presenza di una visione chiara del Paese, di un orientamento generale che regga i singoli provvedimenti, la certezza che i sacrifici di oggi servono ad evitarne di più gravi in futuro. Ecco, questi sono gli elementi che rendono debole la manovra e nei nostri emendamenti ne abbiamo tenuto conto: più equità, maggiori misure strutturali e una maggiore attenzione alla crescita. Ed è su questo punto che desidero Bisogna agire con la revisione generale della spesa pubblica. C'entra naturalmente con il miglioramento delle potenzialità di crescita. È possibile per questa strada non solo contenere l'espansione della spesa, ma cambiarne profondamente la distribuzione nel senso di sostegno allo sviluppo. La coesione sociale è un valore per la crescita. La coesione porta con sé la concertazione, che sempre ha dato risultati positivi: più investimenti e più salari. Con le norme dell'articolo 4 non solo disperdete una convergenza acquisita tra le parti sociali, ma andate in direzione opposta e aggravate in modo intollerabile il dualismo del mercato del lavoro. la Commissione europea sottolineava, nell'esame del nostro piano per le riforme, come debolezza da correggere. Abbiamo proposto un pacchetto di politiche industriali per la crescita e avete detto di no: un pacchetto di proposte per l'efficienza energetica, la *green economy*, la tecnologia italiana e la ricerca. Con pochi fondi si possono ottenere effetti moltiplicativi importanti, compreso un allentamento del patto di stabilità per gli investimenti dei Comuni, che avrebbe un effetto espansivo importante. È importante agire sugli oneri eccessivi sul fattore lavoro. L'ultima grande operazione di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro è stata fatta dal Governo Prodi. Ora aumentate l'aliquota IVA, con gli effetti ben noti sui redditi bassi, e sprecate l'occasione: si sarebbe dovuto destinare il gettito ad abbattere il costo del lavoro e semmai a sostenere i redditi familiari per neutralizzare gli effetti negativi dell'aumento dell'IVA. I conti si sarebbero messi in sicurezza con l'introduzione di una modesta patrimoniale, imposta che non ha effetti recessivi e per cui c'è nel nostro Paese amplissimo margine. Con l'aumento dell'IVA, non accompagnato dalla riduzione di altre altre tassazioni, si incrementa non solo il *record* della pressione fiscale, il *record* della sua iniquità, ma anche il peso dell'aumento delle tasse sulla manovra, superiore a due terzi del suo complesso. liberalizzazioni e le semplificazioni, ci avete fatto sopra un Ministero, ma nulla di concreto è avvenuto. In attesa della inutile ed ideologica modifica dell'articolo 41 della Costituzione, nulla viene fatto, mentre servirebbe un disegno organico, come abbiamo proposto, per ridurre gli oneri amministrativi, stimolare la concorrenza e migliorare la regolazione dei mercati. È incredibile che non abbiate voluto accogliere gli emendamenti dell'opposizione. In molti settori a rete, essenziali per la competitività del Paese, la concorrenza resta scarsa: servizi energetici, del gas in particolare, ferrovie, poste, autostrade ed aeroporti. Abbiamo formulato proposte precise, come per i mercati dei farmaci, delle assicurazioni, delle banche, in cui i consumatori vengono particolarmente penalizzati. Per le professioni, almeno fosse stata introdotta in modo chiaro la rimozione dei vincoli attuali che impediscono l'esercizio della professione in forma societaria per accrescere la competitività delle nostre strutture sul mercato europeo! Nulla è stato accolto. Ma, senza maggiore crescita, non vi sarà risanamento strutturale, e a pagare sarebbero i soliti noti. Ma ciò che hanno visto gli italiani e l'opinione pubblica internazionale sono stati incertezza, ritardo, egoismo elettoralistico e soprattutto la palpabile assenza di una grande visione dei problemi del Paese, dell'ambizione di ricomporne gli interessi con equità. Questo soprattutto paghiamo e di questo portate la responsabilità di fronte al Paese.

credo che in Aula siamo tutti consapevoli che questa è la quarta o quinta fase o puntata di una manovra tutta da venire ancora, che voi del Governo e della maggioranza non volete fare, non potete fare, e temo, soprattutto, non sapete fare, e nei prossimi mesi, se non settimane, seguiranno le altre puntate ben più feroci, perché saremo costretti a rincorrere in condizioni ancora peggiori un pareggio di bilancio sempre più oneroso. Questa è la verità, accade perché non c'è stata e non c'è la consapevolezza della gravità e della portata della crisi, negata per mesi, sottovalutata per altri mesi; né c'è la consapevolezza del vero rischio di *default* dell'Italia e con esso della stessa Unione monetaria europea. In qualche misura non ne comprendete le cause, non le conoscete e, quando scrivete la manovra sotto vera e propria dettatura della Banca europea, neppure due settimane dopo la svuotate, facendo precipitare il Paese in uno spettacolo che non voglio neanche più commentare. commentare. Avete impersonato una sorta di poderoso *deficit* politico di consapevolezza e di comprensione politica di ciò che stava succedendo. anche le liberalizzazioni timidissime sono sparite; quelle già esistenti sono state fatte passare per nuove, ad esempio quella sugli orari di apertura dei negozi; i pochi tagli di spesa, anche quelli della politica, si sono ancora ridotti; sono salve le esenzioni ICI delle attività commerciali del Vaticano ed è salvo il finanziamento pubblico. I saldi sono adesso garantiti per oltre il 68 nel 2012 da più tasse, con evidenti effetti restrittivi sulla domanda interna; e con gli ultimi emendamenti annunciati, la composizione della manovra è ancora più squilibrata dalla parte del prelievo fiscale. Le famiglie a basso reddito saranno colpite ancora più duramente con maggiori tasse da pagare se la delega per la riforma fiscale non verrà esercitata. Come sta scritto, quasi metà della manovra, circa 20 miliardi, dovrà essere garantita dal taglio delle agevolazioni fiscali per tutti, ed intanto quelle per gli asili nido e per le persone disabili. Nelle ultime ore è stata messa una toppa perché il Presidente della Repubblica ed altre istituzioni hanno tirato le orecchie e, soprattutto, il mercato non ha bevuto la bufala dei risultati miliardari della lotta all'evasione fiscale. neanche questa toppa basterà se non affrontiamo con coraggio il macigno del debito e gli ostacoli strutturali che hanno determinato da anni, ancor prima di questa crisi, la stagnazione economica del nostro Paese. In poche parole, credo che i prestatori siano sempre più convinti che l'Italia non sarà in grado di onorare il suo debito e tanto meno di ridurlo con una crescita dello "zero virgola", con l'incapacità di affrontare con coraggio le grandi voci di spesa della previdenza, della sanità, delle riforme strutturali. Va bene mettere le mani alle pensioni. Solo che, con i nuovi emendamenti, anticipate al 2014 l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne, senza neppure prevedere compensazioni per migliorare i servizi che facilitino l'accesso delle donne al mercato del lavoro, la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, dopo che già 4 miliardi del fondo costituito a tale fine nella precedente equiparazione per le lavoratrici del pubblico sono stati scippati e sottratti a pura copertura, credo, di qualche buco. Però vi guardate bene, per il blocco della Lega, che si manifesta ormai come blocco di interessi conservativi, dal seguire dal seguire la strada maestra dell'estensione a tutti del regime contributivo *pro quota* e dell'innalzamento dell'età pensionabile in una forchetta di età da aggiornare automaticamente, che avrebbe dato sicuramente ben altro segnale di rigore e di volontà di ridurre strutturalmente la spesa pubblica. È mai possibile che non si possa mettere le mani su un riassetto del nostro sbalestrato sistema di *welfare*? Occorre insomma, come dicevo, un atto di coraggio. Per essere chiari, sto parlando della necessità di tagliare subito almeno di dieci punti percentuali, se non di più, come ha proposto qualcuno, il nostro debito pubblico. Tradotto in soldoni, sto parlando di almeno 200 miliardi, che dovremmo complessivamente reperire se volessimo davvero essere minimamente credibili. E sapete tutti - non è che me lo invento io - che dai prossimi giorni si dovrà pensare alla vera manovra, ben più dolorosa. Forse sarebbe stato meglio immaginare un prelievo straordinario sui grandi patrimoni. A tale proposito, vorrei far notare che in molti Paesi dell'Occidente ricchi illuminati hanno lamentato di essere colpiti da tasse ridicole e di voler contribuire in maniera più seria al superamento della crisi. In Italia, nonostante lo scandalo dell'evasione fiscale, non molti ricchi hanno proposto una patrimoniale, e mi verrebbe da chiedere al presidente Berlusconi, che è sicuramente uno degli uomini più ricchi del nostro Paese, perché mai non si fa promotore di un prelievo straordinario per salvare il nostro Paese dalla bancarotta: ciò sarebbe, credo, per lo meno un buon avvio.

Aggiungo a tali proposte la convinzione, apparentemente tutta solo radicale, che solo il ripristino della legalità, dello Stato di diritto, di una giustizia giusta e funzionante può essere da sostegno a qualunque misura si voglia poi adottare, perché, in questo Paese, "fatta la legge, trovato l'inganno", e questo è uno dei motivi di scarsa credibilità verso i cittadini e verso l'opinione pubblica internazionale. voglio parlare di Europa, perché ho l'impressione che, così avvitati sui nostri tormentoni, stiamo perdendo di vista, tra le altre cose, lo scenario europeo. Intanto, qualche parola di verità sull'Europa e sui *bond*, perché mi pare che scarsa sia la consapevolezza della classe politica che se l'Europa non saprà superare questa crisi, che coinvolge in modo così drammatico il nostro Paese e l'intero sistema finanziario degli Stati membri, la fine dell'euro sarà inevitabile e le conseguenze sull'economia europea neppure immaginabili. Tuttavia, bisogna che chi parla di *eurobond* dica qualche verità

siano disponibili a garantire con i soldi dei propri contribuenti degli *eurobond* dal rischio che qualche Paese non sia più in grado di onorare i propri impegni: non è pensabile, non è possibile. Come vi viene in mente? quindi dire con molta chiarezza che questi *eurobond* si possono realizzare non solo dando, ovviamente, più risorse al Fondo europeo di stabilità finanziaria, ma soprattutto rinunciando ad un pezzo non piccolo di sovranità nazionale a favore di una politica fiscale europea, di una Tesoreria unica europea, di un Ministro delle finanze europeo, di un bilancio di almeno il 5 per cento del PIL, per essere credibili. Insomma,

Da anni, abbastanza isolati, abbiamo sostenuto che era una follia creare l'Unione monetaria e una moneta comune lasciando che ogni Paese decidesse in assoluta autonomia sulla politica fiscale e di bilancio. Oggi non siamo più soli a dire questo: lo ripete con forza il presidente Napolitano, lo ha ripetuto con forza persino Trichet, lo stanno ripetendo in molti e c'è da augurarsi che, al di là delle pastoie pastoie in cui siete avvolti, la tradizione più vera, europeista, federalista di questo Paese torni con forza ad essere la punta trainante della politica del nostro Paese. Non è assolutamente con furbizie contabili o localismi fuori dalla storia che usciremo dalla nostra crisi: occorre mettere i conti in ordine, grandi sforzi, ma anche riprendere con forza la bandiera federalista spinelliana che avete, temo, troppo calpestato e dimenticato.

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, sarebbe stata necessaria una manovra che incidesse davvero sulla crisi e rilanciasse l'economia del nostro Paese, invece siamo davanti all'ennesima fiducia su un provvedimento *omnibus* che contiene norme, come quelle all'articolo 8, che nulla hanno a che fare con l'urgenza del momento. Se il merito delle norme in tema di lavoro contenute in questo provvedimento è da respingere, lo è certamente anche il metodo con il quale tali norme vengono poste in essere. La decisione di inserire queste norme in un provvedimento finanziario, per di più con carattere di necessità ed urgenza, è un'ulteriore riprova di quella scorrettezza e di quel movente tutto ideologico che sono stati il tratto caratteristico dell'azione del Ministro del lavoro in tutta questa vicenda. Quali siano i benefici che norme come quelle contenute nel Titolo III (ed in particolare nell'articolo 8) possono apportare alle finanze dello Stato non è dato saperlo. Del resto, la stessa relazione tecnica al decreto, per quanto riguarda tali disposizioni, si limita a riportarne in modo sommario il contenuto. Il decreto-legge è, per sua natura, un atto con carattere di necessità ed urgenza. Ma qual è - come ho detto prima - la necessità e l'urgenza di inserire nell'ordinamento disposizioni come quelle di cui all'articolo 8? Semplicemente, attraverso questo strumento, approfittando cinicamente della situazione nella quale il Parlamento si trova costretto ad operare, si cerca di blindare queste norme, impedendo non solo quell'ampio ed approfondito esame delle stesse, che sarebbe invece necessario anzitutto da parte delle Commissioni competenti per materia, ma qualunque serio ed ampio dibattito su di una organica riforma della contrattazione e del mercato del lavoro. Del resto, i metodi del ministro Sacconi si sono potuti ampiamente apprezzare sulla vergognosa vicenda della ventilata norma del riscatto a fini previdenziali degli anni di laurea. A tal proposito tuttavia, è necessario fare una precisazione: se le responsabilità del Ministro sono evidenti, è altrettanto evidente che scelte sciagurate come quella sono figlie anche del comportamento di certi leader sindacali i quali, in maniera assai poco responsabile, prima partecipano ad incontri clandestini con il Governo per accordarsi sottobanco su provvedimenti che nulla hanno a che fare con la tutela dei lavoratori e poi, quando si ritrovano la propria base giustamente in rivolta, si tirano indietro cercando di nascondere le proprie responsabilità o addirittura, in maniera stucchevole, di presentarsi come gli affossatori di provvedimenti che avevano condiviso fino al giorno prima. Ma veniamo ora al merito di quell'articolo 8 che è il peggiore di tutti gli interventi sul lavoro contenuti in questa manovra. In occasione dell'esame di questo provvedimento presso la Commissione lavoro, avevo rilevato la quantomeno curiosa formulazione della relazione illustrativa all'articolo 8. parla infatti di «piena coerenza della disposizione con la tradizione del nostro sistema di relazioni industriali e di lavoro». In realtà, come ho già detto, l'unica tradizione ad essere rispettata è quella del modo di agire del ministro Sacconi. Per l'ennesima volta, infatti, il Ministro del lavoro ha agito in maniera totalmente ed esclusivamente ideologica andando a toccare la materia della contrattazione aziendale e territoriale: una materia che tutte, e sottolineo tutte, le parti sociali avevano espressamente chiesto che restasse nella disponibilità delle parti senza interferenze da parte della politica. Una volta di più, nel caso ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto la dimostrazione pratica di quanto valgano per il Ministro le indicazioni delle parti sociali interessate. Le norme di cui all'articolo 8 sono di una gravità assoluta. Il senatore Castro, in un'intervista pubblicata su «La Stampa», ha parlato in toni entusiastici di «una rivoluzione con salto di Evidentemente, sì, qui siamo in presenza di un salto di effettivamente sessant'anni, ma all'indietro! E se ciò già era abbastanza chiaro a metà agosto, quando questa raffazzonata manovra è stata presentata, la maggioranza si è incaricata negli ultimi giorni di rendere la cosa ancor più palese. All'inizio si è tentato di far passare l'idea che queste norme fossero semplicemente una traduzione in legge dell'accordo del 28 giugno di quest'anno. Tutti coloro che osavano anche solo mettere in dubbio ciò venivano colpiti dagli strali del Ministro del lavoro. Tra questi, il Servizio studi del Senato, il quale aveva il grave torto di avere fatto il proprio dovere, segnalando il rischio che la normativa in questione facilitasse un possibile aggiramento delle garanzie previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Abbiamo letto su questa norma difese accorate, insinuazioni su presunte invidie di giuslavoristi dell'opposizione per non aver potuto realizzare loro una simile meravigliosa riforma, grandi discorsi sul vero liberalismo, invettive contro i "bastardi anni Settanta" (peraltro, a quanto pare, poco apprezzate). Al netto delle chiacchiere, i fatti però restano: qui si cita solo formalmente l'accordo interconfederale di giugno, ma l'intenzione lampante è quella di scardinare quell'accordo. Del resto, gli emendamenti approvati in Commissione (ed ora recepiti nel maxiemendamento) vanno esattamente in quella direzione. Paradossalmente risulta più apprezzabile la cruda sincerità di quegli interventi, che chiariscono una volta per tutte la totale derogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione, piuttosto che i patetici interventi del ministro Sacconi che fino all'ultimo ha cercato di sostenere che l'articolo 8 non avrebbe in nessun modo leso le garanzie dei lavoratori. Si stanno spostando materie delicatissime, tra cui quella del recesso dal rapporto di lavoro, ad un livello in cui le organizzazioni sindacali hanno forza contrattuale nettamente ridotta. L'inserimento dei "sindacati territoriali" (ennesimo contentino al Sindacato padano) ha come conseguenza l'aumento del rischio (peraltro già presente nel testo originario) che le aziende possano concludere accordi anche solo con sindacati di comodo. Il tutto espresso in una disposizione pasticciata ed in più parti ambigua la quale, nel migliore dei casi, non farà altro che aumentare il contenzioso. È la stessa tecnica che abbiamo già visto in occasione del collegato lavoro: il legislatore non si assume la responsabilità di dettare una normativa chiara e scarica sulla magistratura del lavoro l'onere di interpretarla. Le cosiddette garanzie che sarebbero previste sono ridicole. Siamo in piena crisi, le imprese sono in difficoltà, la manovra strangolerà i consumi e la liquidità delle aziende, e in una tale situazione si mette a punto un provvedimento che agevola la possibilità di mandar via le persone. È ovvio che, in una situazione di crisi come quella attuale, se un imprenditore viene messo nelle condizioni di poter licenziare, quella diventa la tentazione, la via più facile o addirittura la via obbligata, visto che di fatto non vengono indicate altre strade. L'argomentazione secondo la quale il contratto che verrà firmato a livello aziendale sarà frutto di un compromesso con i sindacati è ridicola. I rapporti di forza fra un'azienda che ha il coltello dalla parte del manico e i dipendenti minacciati dal fallimento sono evidenti. Ad esempio, si potrà sempre dire loro: «se non fate questi straordinari, ve ne andate a casa»; oppure: «se non consentite la deroga all'articolo 18 per tagliare quelli che reputiamo i rami secchi, si chiude». È lo stesso metodo ricattatorio che è stato usato nelle vertenze FIAT a Pomigliano e a Mirafiori, dei cui accordi ora infatti si dispone l'applicabilità generale. Anche in questo caso, siamo in presenza di una norma grave e del tutto ingiustificata, che si riduce ad un ennesimo regalo ad una dirigenza aziendale la quale, dopo aver ottenuto praticamente tutto ciò che voleva, non ha rispettato nessuno degli impegni riguardo i finanziamenti ed il rilancio degli stabilimenti automobilistici italiani. Vengono così spuntate anche le poche residue armi giuridiche nelle mani dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, facendo di fatto decadere i ricorsi già presentati presso la magistratura del lavoro. Signor Presidente, abbiamo più volte detto che non avremmo fatto sconti ed avremmo anzi dato battaglia per tutelare l'interesse dei cittadini e dei lavoratori italiani. Confermiamo anche qui questa posizione. La cosa più sbagliata che un partito di opposizione può fare in questo momento è diventare la sponda di un Governo che mentre invoca responsabilità da parte degli altri, tenta di scardinare i diritti di

infatti obbligati a modificare i nostri stili di vita, pubblici, sociali e privati, se vogliamo mantenere i diritti acquisiti, che fanno dell'Italia un Paese civile ed una delle potenze a cui il mondo guarda. il mondo guarda. Il maxiemendamento così pasticciato che c'è stato presentato *in extremis*, su cui si chiede per l'ennesima volta la fiducia, non è sufficiente; nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica e nonostante noi eravamo disponibili a discutere ed anche disponibili ad approvarne alcune parti, non è però sufficiente. È da agosto che il Terzo Polo propone una manovra alternativa, che punta su due aspetti: rigore massimo e crescita. Se non c'è infatti questo binomio, non c'è futuro per l'Italia, per l'economia, per la finanza e per tutto il popolo italiano. Non dobbiamo continuamente rincorrere la spesa pubblica corrente aumentando le imposte e le tasse. Proponiamo di azzerare il *deficit* tagliando la spesa corrente e soprattutto puntando allo sviluppo.

colpisce, ancora una volta, chi oggi versa nelle casse dello Stato quotidianamente, cioè le piccole imprese e i consumatori che pagano alla fonte. Voi avete scelto di introdurla e non avete nemmeno ascoltato coloro che questa estate avevano dichiarato una disponibilità ad introdurre questa riforma; penso, per esempio, alle parole del segretario della CISL Bonanni, che diceva che, se si vuole affrontare questa scelta, deve essere inserita in una riforma complessiva del sistema fiscale, per passare dalle persone alle cose. Però, qui, oggi - siccome non siccome non c'è situazione peggiore di chi non vuole ascoltare, come voi non avete voluto ascoltare - voi introducete tale misura, io mi permetto di dare un suggerimento e di fare una proposta.

È indispensabile affiancare uno strumento di monitoraggio dell'andamento dei prezzi, per evitare che si indebolisca il potere di acquisto delle famiglie, già duramente provate dalla crisi occupazionale e dai tagli alla spesa sociale, e di provocare una contrazione dei consumi. Bisogna partire da strumenti efficaci e concreti, per far sì che i prezzi non aumentino colpendo i redditi delle famiglie, non provochino l'aumento del tasso di inflazione e la depressione dei consumi. È doveroso fare un confronto; ero presente in quest'Aula dal 2001 al 2006, quando voi della maggioranza criticavate ripetutamente il Governo Prodi che aveva inserito l'euro. L'allora ministro dell'economia Ciampi, divenuto poi Presidente della Repubblica, aveva previsto le commissioni provinciali di controllo, organismi che erano stati istituiti, ma che il vostro secondo Governo non ha mai reso operativi, e così i prezzi per i cittadini erano e sono tuttora quasi raddoppiati. Oggi, di fronte all'aumento di un punto dell'IVA, è indispensabile istituire commissioni provinciali di controllo e una commissione nazionale che monitori l'andamento dei prezzi che sia, al tempo stesso, dotata di poteri cogenti e sanzionatori. Non deve e non può essere la classica autorità "all'italiana" poiché la storia ci ha insegnato che le nostre autorità di controllo e vigilanza finiscono con ridursi a meri strumenti non operativi.

Serve un atto di responsabilità dei mondi economici, sociali e politici. Monti diceva che da sola una parte politica (la vostra) non riesce ad inserire la patrimoniale, così come da l'altra parte politica (il Partito Democratico e la sinistra) non riesce a formulare la riforma delle pensioni. Solo insieme, se vogliamo assumere un atteggiamento di responsabilità e di verità, possiamo ottenere questi due grandi obiettivi a cui l'Italia non può solo guardare, ma è obbligata a realizzare. «Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà». Non è una mia affermazione. Ce lo ricordava molti secoli fa Niccolò Machiavelli, ed oggi quella massima vale più che mai come massima di vita per la vita politica di questo Governo. «Un'epoca storica di straordinarie e accelerate novità porta con sé, come un fiume in piena, abbondanze e minaccia,

ricordare qui oggi perché la sua grande lezione politica serva ad «assicurare un argine» - sono ancora le sue parole - «garantire una direzione, scrutare una foce, riguarda la disponibilità di tutti e l'attitudine ordinatrice della politica... Siamo convinti» - continuava Mino Martinazzoli - «che se la politica impegnasse metà del tempo che occupa intorno alle cose impossibili» - quello che voi continuate a fare «per esercitarsi sulle cose possibili, i risultati sarebbero assai più probanti di quanto sinora non siano. non siamo all'inseguimento di una risposta totale e definitiva, ma sollecitiamo una coscienza, un'attitudine a indagare e a lavorare sui nessi e sulle relazioni che stringono drammaticamente i nodi di scelte molteplici», e, lo sappiamo,

Signor Presidente, «vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo».

continuiamo a non imboccare la strada giusta. Il Governo ha posto la fiducia su un provvedimento certamente indispensabile ma probabilmente perfettibile, se si fossero verificati alcuni presupposti e se si fosse registrata una maggior attenzione. Presidente, colleghi, se qualcuno sperava che il faticoso lavoro svolto in queste settimane dal Governo e dalla Commissione bilancio potesse servire a colmare la situazione che si era venuta a determinare dal punto di vista finanziario o che gli interventi compiuti potessero calmare la bolla speculativa che si è registrata in tutte le Borse del mondo, ebbene in queste ore ha avuto una brutta notizia. notizia. Probabilmente non erano questi i provvedimenti che ci si attendeva. Probabilmente la finanza e l'Europa volevano di più, e bene ha fatto il Governo a predisporre una manovra aggiuntiva che sommasse al lavoro svolto la scorsa settimana dalla Commissione bilancio e dal Governo ulteriori interventi in grado di mettere in ordine i conti dello Stato. che il bilancio dello Stato potesse essere messo in ordine solo procedendo con tagli orizzontali alle spese della pubblica amministrazione, senza prevedere interventi anticiclici in grado di rilanciare il sistema Paese e l'economia interna, probabilmente si sbagliava. insieme agli interventi che servono a contenere gli sprechi e a ridurre i costi impropri della pubblica amministrazione, è necessario pensare ad interventi in grado di invertire l'ordine economico vigente per consentire all'economia, che nel 95 per cento dei casi nel nostro Paese è composta da piccole e medie imprese, di vedere una luce all'orizzonte.

alla scelta che il Governo ha fatto di non avviare un percorso di recupero rispetto ai crediti che molte aziende italiane vantano nei confronti della pubblica amministrazione:

il funerale del bilancio dello Stato ma il funerale di alcune centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, e con esse

la drastica e strutturale eliminazione degli sprechi - questo provvedimento si colloca proprio nel solco degli sprechi, delle ridondanze e dei privilegi senza superare il dualismo territoriale che esiste in questo Paese, che richiede una appropriata azione politica di natura infrastrutturale, di grande e piccola dimensione, vuol dire che non vuole il bene del Paese (probabilmente non conosce il Paese). Se qualcuno pensa che i consumi di questo Paese si possano rilanciare senza sbloccare la crisi occupazionale e senza superare le incertezze del precariato, facendo sperare in un reddito costante, permanente, in grado di favorire l'utilizzazione di una parte di esso a favore dei consumi, probabilmente farebbe bene a ripassarsi Keynes e anche Smith. Se qualcuno ritiene che in un momento di recessione e di crescita esponenziale della povertà si possa abbassare il livello dei servizi erogati dagli enti locali, vuol dire che non conosce la realtà della povertà nel nostro Paese, una povertà in cui un numero sempre maggiore di famiglie italiane è costretto a dibattersi. Personalmente considero i tagli orizzontali una sorta di esercizio di socialismo reale residuo del veteromarxismo, e penso invece che uno dei compiti più importanti della politica debba essere la scelta: anche dolorosa, ma la scelta. la manovra presentata dal Governo certamente costituisce un atto che va in direzione delle scelte, che si possono condividere o meno, ma sono scelte coraggiose e importanti. Non credo che nel nostro Paese lo scontro politico possa essere limitato a chi tassa di più e a chi tassa di meno. Credo che le scelte debbano portarci a decidere chi tassa meglio e come spende meglio le tasse riscosse. Per noi, spenderle meglio significa permettere all'economia del Paese una ripresa significativa, forte,

Se qualcuno pensa che l'economia si salva screditando la politica o i politici è bene che sappia che il discredito verso la politica si trasforma molto presto in discredito verso la democrazia, il pauperismo politico e culturale nella storia prelude sempre a momenti di grande violenza, di grande travolgimento dei diritti umani, dei valori di reciproca solidarietà. Dunque, quando ci accingiamo a cavalcare il pauperismo politico e populista, che in questi mesi ha caratterizzato la stampa italiana, dobbiamo farlo sapendo che questa può anche costituire la prima mossa, ma dopo ce n'è un'altra che potrebbe travolgere e non far perdere semplicemente la partita. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente,

E dunque, orgogliosamente, rivendichiamo l'inserimento in questa manovra delle somme relative al FAS, destinato alle opere regionali, regionali, che consentiranno ai Comuni e agli enti locali di utilizzare le risorse dei vari piani di opere pubbliche attraverso uno fondo di rotazione per le progettazioni. Rivendichiamo altresì con orgoglio la primogenitura sul rilancio dei temi riguardanti lo sviluppo del Sud. Un rilancio di cui molto opportunamente - e di questo lo ringraziamo - il Presidente del Senato si è fatto carico, ipotizzando la nascita di una sorta di laboratorio per il Sud all'interno del quale - come egli ha opportunamente detto intervenendo in Commissione bilancio in apertura dei lavori

quegli steccati che fino a questo momento hanno impedito al Sud di trovare le energie necessarie per contribuire a ricomporre il dualismo cui facevo prima riferimento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Viespoli tra qualche ora annuncerà il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud alla questione di fiducia posta dal Governo, ma credo che rispetto a questo tema sia importantissimo sottolineare una questione. non abbiamo voluto sottrarci al responsabile compito di rispondere con i mezzi di cui disponevamo all'emergenza del Paese,

non è facile non cedere alla polemica politica più immediata, perché il Governo, obiettivamente, in questi ultimi due mesi si è comportato nel modo più scriteriato e approssimativo, improntando la sua azione soprattutto all'improvvisazione del caccia e metti. Del resto, la manovra licenziata l'11

dallo iato, dalla contraddizione estrema e dal paradosso che c'è e si riscontra tra il modo in cui il ministro Tremonti aveva analizzato e giudicato il sopravvenire della crisi in questi anni (tutti ricordiamo

culturale) e il modo approssimativo, superficiale e dilettantesco con cui si sono proposti i provvedimenti e le misure nelle diverse versioni di questa manovra dell'estate. Tanto acuta era stata la teoria quanto disastrosa la pratica. Ora, se non ci fossero di mezzo il futuro del nostro Paese, le condizioni del nostro debito sovrano, ci sarebbe quasi da sorridere e, forse, anche da essere soddisfatti. Ma purtroppo

La verità dei fatti sta però in altro: siamo in presenza semplicemente di coperture garantite ad una manovra che coperture Lo abbiamo detto noi nel dibattito in Commissione, l'ha detto l'Unione europea, lo testimoniano i fatti e lo dimostra purtroppo anche l'accoglienza che la manovra ha avuto in queste settimane sui mercati. Oggi, soprattutto grazie all'intervento sull'IVA, di cui dirò, questa manovra vede un tasso di copertura sicuramente più alto e più significativo di quello improbabile che aveva prima.

si scontra con un livello di pressione fiscale che non ha avuto precedenti nel nostro Paese. Infatti, tutti ormai si concorda sul fatto che la pressione fiscale sia del 44 per cento ed in aumento nei prossimi due anni. Questo è un primo elemento di diseguaglianza, che definirei trasversale, che non riguarda tanto la distribuzione dei redditi, quanto le possibilità e le opportunità anche per i ceti sociali benestanti, che vedono nell'evasione fiscale, che ancora vive in maniera fortissima, un elemento di messa in discussione della concorrenza nell'attività economica. Una pressione fiscale che si incrementa e si inasprisce in presenza di un'evasione fiscale che ha le dimensioni che tutti conosciamo diventa un gravissimo elemento

che si sono avuti in questi anni nel nostro Paese a seguito della globalizzazione e delle politiche, anche specifiche, che il Governo ha messo in campo, si è voluto, anche con questa manovra, colpire in modo unidirezionale.

Ma c'è un macigno che grava ancora, proprio nei termini dei rischi di ulteriore disuguaglianza sociale. La delega fiscale aveva in qualche modo prenotato l'incremento dell'IVA di un punto. Si diceva, e si dice nella delega fiscale, che l'IVA sarebbe stata una specie di misura di salvaguardia perché si potesse avere, dalla riforma fiscale e assistenziale, quel gettito di 20 miliardi che è atteso. Ma nel momento in cui l'IVA viene utilizzata, oggi,

se tutto graverà sulla riduzione e sulla compressione delle deduzioni, saremmo davvero in presenza di una macelleria sociale di una portata tale che nel nostro Paese non si è mai vista.

Noi abbiamo invece bisogno di tutt'altro. Avremmo bisogno di un approccio strutturale e non straordinario ai problemi. L'approccio strutturale è quello previsto da alcuni emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico. E resta comunque aperto il tema

Io resto convinto, e lo dico a titolo personale, perché non voglio in alcun modo coinvolgere il mio partito in questa valutazione, che il modo migliore sarebbe quello di avere una patrimoniale strutturale organica, leggera, sul modello francese,

ricordare una piccola ma significativa vicenda, che testimonia come nessuno voglia rinunciare in questo Paese ai propri, piccoli privilegi. E questo è tanto più grave quando riguarda noi che sediamo in quest'Aula.

che il parlamentare che si trova in questa condizione da oggi semplicemente vedrà una riduzione dell'indennità che si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 e del 40 per cento sopra i 150.000 euro. È una vergogna. è una vergogna, perché non si possono mandare segnali di questa natura *(Applausi dal Gruppo PD)* nel momento in cui chiediamo all'Italia e agli italiani di fare dei sacrifici importanti per salvare il nostro Paese.

Noi non siamo per interventi straordinari, per le gride manzoniane, per improbabili risolutivi interventi di carattere locale, che spesso diventano una sorta di delazione sociale. Siamo piuttosto per l'ordinarietà e la tracciabilità.

Perché la lotta all'evasione fiscale si fa in maniera semplice, soprattutto creando la congruenza tra reddito e patrimonio, allegando alla dichiarazione dei redditi le variazioni patrimoniali, consentendo e disponendo la comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari. cancellato la proposta iniziale di questo decreto-legge, con la quale rendevate obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi l'elenco degli intermediari finanziari con cui ciascun contribuente opera, con cui ciascun contribuente opera, la dice lunga sull'incapacità e sulla confusione totale che regnano nella maggioranza. Esiste già l'anagrafe dei conti e dei depositi, come abbiamo spiegato, anche se non ce n'era bisogno perché lo sa benissimo e meglio di noi, al ministro Tremonti in Commissione. L'importante è come si accede a quell'anagrafe e, soprattutto, come si riesce a mettere in campo un'azione di lotta e contrasto all'evasione fiscale che sia effettivamente efficace.

come di qui a fine anno circa 140 miliardi di euro del debito italiano andranno rinnovati sui mercati internazionali, e di questi quasi la metà dovranno trovare una nuova sottoscrizione nel mese di settembre. Questo significa che il nostro Paese deve presentarsi con forza e credibilità. Ecco, noi da qui vogliamo ancora dire che l'Italia è un Paese forte e credibile, e lo sarà ancora di più nel momento in cui questo Governo prenderà atto di non essere più in condizione di rispondere - se mai lo è stato - alle esigenze del Paese. Siamo una grande forza di responsabilità nazionale: diciamo alto e forte che c'è bisogno di una manovra, che vogliamo scomporre e ricomporre, ma diciamo anche che in questo modo voi state rischiando di mettere a repentaglio la nostra credibilità. Siamo qui come forza di opposizione nazionale a garantire in Italia e

erano in grado, in questo momento di grave crisi internazionale, di andare avanti tranquillamente. ad un confuso susseguirsi di decreti, di interventi che chiamiamo economici, per poter mettere un argine ad una valanga che sta travolgendo tutto e tutti. Siamo un Paese ormai non credibile, dileggiato dal mondo e tutti ormai si sentono in grado di poter riprendere, rimproverare e commentare negativamente gli interventi del nostro Governo. Di fatto siamo un Paese commissariato, anzi - se mi è consentito - abbiamo un Governo commissariato. In questa manovra c'è un unico

dove si incontravano partiti e *leader* per discutere delle questioni fondamentali della nostra Nazione. Oramai i centri decisionali della nostra politica sono diventati Arcore e Lorenzago, e purtroppo oltre il danno vi è anche la beffa: le decisioni che vengono prese sono confuse ed inefficaci, durano lo spazio di un sospiro dei vari organismi internazionali che immediatamente li bocciano e il giorno dopo si ricomincia. È quanto è successo in queste drammatiche settimane: proposte annunciate come risolutive e smentite il giorno dopo, interventi - possiamo dirlo - anche accorati del nostro Capo dello Stato che invitava alla partecipazione collettiva, all'assunzione di responsabilità in un momento difficile per tutti. Sono però inesorabilmente caduti nel vuoto. La maggioranza ha fatto, ha disfatto, ha annunciato e ha smentito se stessa. C'è stato un vortice di voci, di proposte, di controproposte, una confusione veramente irresponsabile. Alla fine, senza un minimo di credibilità, né all'interno della nostra società, né di fronte al resto del mondo, ha presentato una manovra priva di tagli di spesa, senza provvedimenti sulla crescita, che è veramente un nostro grandissimo problema, e senza interventi veri, efficaci su famiglie e aziende. L'unica cosa che ha fatto è stato prevedere un aumento della pressione fiscale per tutti gli italiani. Api-FLI, come Terzo Polo, abbiamo presentato un pacchetto di proposte alternative che non sono state prese assolutamente in considerazione. Siamo partiti dalla riduzione della spesa pubblica, quella vera, seria, da utilizzare per ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Poi abbiamo fatto la nostra proposta sul vero contrasto all'evasione fiscale con il conflitto di interessi fra chi acquista e chi cede beni e servizi. Avevamo fatto una proposta

la riduzione della pressione fiscale su tutti gli italiani, che doveva svilupparsi utilizzando le maggiori entrate della lotta all'evasione, creando un fondo che fino al 2014 servire per la riduzione del debito e dal 2014 in poi unicamente per la riduzione del carico fiscale. Questa nostra proposta è stata modificata, sterilizzata perché in sostanza sono state inserite

Questo emendamento è stato votato dalla Commissione bilancio e democraticamente il Governo l'ha escluso dal maxiemendamento su cui Questo emendamento che avevamo studiato, tecnicamente perfetto, era un aiuto alle piccole e medie imprese che hanno crediti atavici con la pubblica amministrazione;

certo che hanno con la piccole e medie aziende, e queste, in un momento di grande difficoltà economica, avrebbero avuto una garanzia in più per andare presso le banche di loro fiducia ed avere sollievo finanziario utilizzando un semplice certificato che le pubbliche amministrazioni dovevano dare. Mi dispiace

che, in un disegno di modernizzazione e razionalizzazione del nostro Stato, saremo costretti a discutere a breve: questo è indiscutibile, lo sappiamo tutti, ma nessuno ha il coraggio, il Governo *in primis*, di portare avanti un simile ragionamento.

uniformarla a quella esistente nel resto d'Europa, eliminando storture e privilegi nei confronti di tutti, poiché tutti dobbiamo dare un contributo, a cominciare da chi ha di più: anche nel sistema pensionistico, questo è il principio da cui si deve partire per una riforma seria,

stasera ci sarà l'ennesimo voto di fiducia richiesto dal Governo su un provvedimento importantissimo, determinante per tutti. Ci auguriamo tutti che i problemi vengano risolti, ma probabilmente, in maniera empirica, possiamo affermare che questo sicuramente non sarà il modo per porci al riparo dalle bufere che stanno arrivando. Tra pochi giorni o tra qualche settimana saremo ancora qui per approvare la legge di stabilità, e sicuramente vi sarà bisogno di un ulteriore intervento sulla finanza pubblica.

sarà necessario ed indispensabile ripensare alla possibilità, e soprattutto alla capacità, di un Governo che, per sottovalutazioni, temporeggiamenti, scandali e, come abbiamo visto in questi giorni, per meri interessi di bottega soprattutto elettorali, sta lentamente, inesorabilmente ed irresponsabilmente portando la nostra Patria allo sfascio più completo. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la maggioranza e il Governo si sono comportati di fronte a questa congiuntura difficilissima con un'irredimibile irresponsabilità: hanno negato la crisi e ripetutamente negato la rilevanza del momento, inaugurando una fase di manovre finte, quali l'opposizione ha dato anche prova di un senso di responsabilità forse perfino esagerato: di fronte al richiamo del Presidente della Repubblica l'opposizione ha accettato di non opporre la resistenza che pure il Regolamento permette (cioè quella pochissima che è rimasta) e ha fatto passare una manovra insufficiente, malscritta e rabberciata in soli tre giorni. Quella poteva essere l'occasione in cui un Governo degno di questo nome, poggiandosi anche su un consenso a tempo da parte dell'opposizione, avrebbe potuto perlomeno provare ad affrontare la durezza della situazione. Invece, ha preferito far passare una manovra ridicola, in cui tutti i problemi venivano rinviati agli anni successivi, e si faceva soltanto finta di prendere la misura alla situazione allarmante.

ha richiesto la convocazione delle Commissioni 1a e 5a riunite di entrambe le Camere apparentemente per discutere la proposta di modifica dell'articolo 81 con l'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio. In realtà, ha utilizzato quella occasione come una sorta di platea parlamentare informale in cui svolgere una conferenza stampa con una sua relazione scadentissima, tanto presuntuosa quanto scadente, e purtroppo i *leader* di tutti i partiti, compreso il mio, secondo me hanno fatto l'errore capitale di accettare questo tipo di scambio: di scambio: non hanno parlato i commissari, ma soltanto i *leader* politici e la cosa si è trasformata in qualcosa di tipo mediatico, totalmente insulso, senza prodotto e in un certo senso la serietà del lavoro di Commissione, se poteva esservi, è stata negata. Questo fa parte del criterio scenografico con cui si affrontano i problemi più seri. La maggioranza e il Governo hanno improntato la loro azione ad una teoria che è rappresentata dalla battuta: «Non metteremo mai le mani nelle tasche degli italiani!». In realtà, invece, il Governo non ha fatto altro. Forse non l'ha fatto estraendo direttamente con mani adunche, come quelle rappresentate dai caricaturisti classici, la moneta dalla tasca del cittadino, ma in realtà ha determinato un processo di impoverimento generale di cui oggi abbiamo purtroppo il ritratto espressivo nella realtà che ci circonda. Più di un collega un collega ha citato la questione dei crediti inesigibili da parte delle imprese, ma non c'è solo quell'aspetto: i Comuni sono stati assassinati dalla abolizione dell'unica imposta federalista presente in Italia, che era la possibilità di intervenire sull'ICI, sull'ICI, e i Comuni impoveriti si sono dovuti rivalere alzando i costi dei servizi, rinunciando ai servizi e così via; la scuola è stata avviata ad un processo di avvilimento che sembra non avere fine; l'università è ormai immersa in un lungo percorso depressivo e la ricerca è privata di risorse, questo nel momento in cui le società affluenti si difendono nella globalizzazione soprattutto accentuando la potenza del lavoro intellettuale. E certo, l'Europa e l'Italia non possono pretendere di competere competere con i mercati internazionali a basso costo del lavoro: l'unica maniera che potrebbero adottare sarebbe quella di un rinforzo straordinario, eccezionale della potenza del lavoro intellettuale e quindi di un rilancio delle risorse per la ricerca in senso lato. Invece niente di tutto questo: il Governo e la maggioranza hanno manifestato un'indifferenza patologica alle questioni del lavoro alle questioni del lavoro e non solo del lavoro giovanile. Credo che i sensori più aggiornati ci facciano conoscere un processo che oggi non è ancora quantificabile, ma che secondo me è il preoccupante processo sociale dell'immediato futuro: l'insorgenza e la diffusione di un vero e proprio campo di lavoro gratuito, soprattutto intellettuale. Nessuno oggi si sogna di chiamare un idraulico e di non pagarlo,

La diffusione del lavoro gratuito smembra anche la forza propulsiva del lavoro intellettuale, che si sente ridotto così ad una sorta di appendice trascurabile, avvilita. Come si fa a confrontarsi con una situazione di questo tipo?

è assoluta indifferenza su questo piano anche da parte delle forze che predicano un loro attaccamento al territorio. La Lega non fa che ripetere ossessivamente del proprio radicamento sul territorio; ebbene, questi soggetti così fortemente radicati sul territorio non hanno saputo né prevedere né rimediare ai ai danni di una alluvione prevedibilissima nel Veneto: quando una Regione giace in pianure che sono al di sotto del livello dei fiumi pensili, il minimo che si possa pensare è che bisogna lavorare per mantenere gli argini. E neppure questo hanno fatto, coloro che sono radicati al territorio, e poi non ci sono soldi nemmeno per rimediare ai danni: siamo in una situazione veramente tragica. La manovra è iniqua, lo hanno già detto molti colleghi. In questo contesto di iniquità totale, come si fa a protestare contro la CGIL perché fa sciopero? Chi avanza queste critiche sa cosa vuol dire davvero mettersi nei panni di chi vive con un basso reddito e che si confronta con delle difficoltà quotidiane pazzesche, da non riuscire nemmeno più a fare fronte alle necessità di mandare i figli a scuola? Ma come si fa a criticare la CGIL? Si vorrebbe forse l'unanimismo del sostegno sociale di tutti a manovre che non hanno nemmeno la percezione di un minimo di giustizia sociale? Nello stesso tempo li si schiaffeggia, dimostrando che si è del tutto indifferenti ad azioni significative ed incisive contro i redditi alti. Questo dobbiamo vedere. Si danno rabbuffi polemici alla CGIL e nello stesso tempo si fa una manovra dove i redditi alti sono sostanzialmente salvati. La manovra non incide su questo. La captazione di risorse dove più ci sono è sostanzialmente vanificata. Voglio dirlo in termini costituzionali: in Costituzione l'articolo 53 dice chiaramente che l'imposizione fiscale è progressiva. Vi farei rileggere le parole dell'onorevole Scoca, democristiano DOC, che sosteneva nella Costituente che l'imposizione non doveva essere proporzionale, per cui se uno è ricco paga di più e se uno è povero paga di meno, ma quanto più uno è ricco tanto più deve pagare e tanto meno deve pagare, se uno è povero. Ecco, la legittimità democristiana dell'articolo 53 della Costituzione è negata in modo diretto. Oggi quel che è certo è che la progressività dell'imposizione fiscale funziona al rovescio.

dall'inizio della vita alla fine ad un numero e questo numero permette di identificare l'insieme delle sue operazioni, il che impedisce l'evasione fiscale. In realtà, basta volerlo fare. In effetti il ministro Visco aveva cominciato a farlo ed era riuscito a recuperare dell'evasione fiscale: perché non si può ritornare ad un cammino di quel tipo? Poi c'è la questione di fronteggiare l'irrazionalità dei mercati. Alcuni commentatori intelligenti ed approfonditi hanno parlato di irrazionalità dei mercati, nel senso che nel momento in cui la crisi si avvita, il mercato si infiamma e può prendere dei parossismi che non sono non controllabili immediatamente; ma se c'è una maniera in cui non ci si può confrontare con l'irrazionalità dei mercati, atteso che essa esista, è l'irrazionalità del comportamento. Quando un Presidente del Consiglio si permette di dire la sciocchezza sesquipedale che i mercati sono, quando si comportano così, come l'orologio guasto che segna due volte al giorno l'ora giusta e per il resto no, dimostra chiaramente una totale mancanza di credibilità di fronte ad un fenomeno che al limite, proprio perché irrazionale, richiede un *surplus* di razionalità, non lo si può scongiurare semplicemente come si fa con Qui siamo di fronte al punto finale del mio intervento: la mancanza totale di credibilità del Presidente del Consiglio. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio ricattabile e ricattato, in preda a lenoni, meretrici e *brasseur d'affaires*, una persona di cui si può dire qualsiasi cosa, perché ormai è segnato a fuoco dalla verità conosciuta. Persino gli aspetti miserabili della sua vita, che non sono il succo fondamentale della nostra politica, incidono su questa situazione. Ma non c'è solo quello, c'è la sua totale inaffidabilità politica: il titolare del conflitto d'interessi, la persona più ricca d'Italia che sdegna qualsiasi approccio realistico alla vita associata italiana. E poi lui stesso si è auto-condannato con la sua incontinenza verbale,

signor Presidente. Lo Zapatero tanto idolatrato dalla sinistra, nel momento in cui ha capito che la sua storia era finita, ha deciso chiaramente e serenamente di non ricandidarsi. In Germania e in Inghilterra i *Premier* che sono giudicati inadeguati a continuare la loro esperienza vengono messi da parte dai loro partiti.

Signor Presidente, parto da qualche considerazione su due aggettivi che hanno connotato in queste ore l'intervento del Governo, l'intervento con cui il Governo ha cercato di rammendare la tela di Penelope con cui ha gestito l'inqualificabile percorso della manovra di correzione dei conti. Il Governo e ancora qui questa mattina il relatore hanno parlato di tempestività, di intervento tempestivo e di rafforzamento della credibilità della manovra. Non voglio commentare l'esito nel suo complesso sotto il profilo della rispondenza a questi due imperativi, peraltro imposti e incredibilmente non assunti fin da subito a vincolo di massima responsabilità da parte del Governo stesso. Mi pare purtroppo, e lo hanno già detto ampiamente i colleghi che mi hanno preceduta, che ci sia evidenza della loro inadeguatezza. Voglio limitarmi a valutarli in relazione ad un terzo analizzatore per noi fondamentale: la capacità della manovra di garantire la sua sostenibilità sociale, profondamente convinta come sono che il successo degli interventi economici e finanziari che contiene sia indissolubilmente legato alla sostenibilità sociale, anche a prescindere da ogni valutazione sulla giustizia e sull'equità, ma per mere ragioni economiche. Un primo elemento: circa la metà delle minori spese e delle maggiori entrate cui è legata la tenuta dei saldi, sono ricollegate all'attuazione della riforma fiscale e assistenziale da cui devono essere recuperati 20 miliardi in due anni, più altri 20 per il terzo. Nel caso in cui la riforma non rispetti temporalmente o quantitativamente gli obiettivi assegnati, scatterà la cosiddetta clausola di salvaguardia termine assai beffardo per commentare un risultato tecnico - consistente nel taglio lineare (prima del 5 per cento e poi del 20 per cento) di tutte le agevolazioni fiscali vigenti o, in alternativa, nell'aumento dell'IVA o delle accise. Oggi con il maxiemendamento il Governo ha utilizzato il primo paracadute: ha aumentato l'IVA, stimando da questo intervento entrate per quattro miliardi, che sono esattamente l'obiettivo assegnato per il primo anno all'intervento di riforma assistenziale. abbiamo anticipato ad oggi il primo obiettivo assegnato alla riforma fiscale ed assistenziale all'anno successivo. Abbiamo bruciato il primo pacchetto. È immaginabile, quindi, che sarà necessario porre massima portata e massima attesa di risultato agli obiettivi di riduzione di spesa assegnati alla riforma dell'assistenza, visto che il parametro fiscale è stato già utilizzato. Gli obiettivi generali contenuti nei principi di delega prevedono che la riforma garantisca protezione dei diritti sociali, adeguatezza, equità e attuazione del principio di sussidiarietà. Questi sono i quattro pilastri della riforma. Gli interventi dovranno compiersi su un *plafond* di spesa sociale di competenza statale che ammonta a circa 30 miliardi di euro, prestazioni agli invalidi civili, 9 tra assegni familiari e prestazioni per maternità e i restanti 5 suddivisi tra assegni sociali ed integrazioni al minimo delle pensioni. Su cosa interverranno allora i risparmi? Considerando non realistico che gli interventi, pur doverosi, sulle false invalidità o sulla riqualificazione dei criteri di accesso possano portare a riduzioni della spesa dell'ordine di due cifre, quali quelle che ci si dovrebbe aspettare, e considerando viceversa realistico un contenimento della spesa per non più di qualche miliardo di euro, è pressoché scontato prevedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nell'unica forma ormai disponibile, visto che l'intervento sull'IVA è stato già fatto e che immagino non si voglia attuarne un altro da qui a qualche mese, considerata la portata che l'intervento sull'IVA ha fin da ora e i possibili esiti in termini di attese inflazionistiche. Dovrà quindi essere effettuato, molto probabilmente, almeno il primo dei due tagli lineari ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che hanno come destinatari prevalenti i redditi da lavoro e da pensione: parliamo delle già scarsissime detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie, per le spese di cura ed assistenza ai congiunti non autosufficienti, delle detrazioni per la prima casa e per i mutui. Parliamo cioè in larga parte del reddito delle famiglie, della loro capacità di sostenere i propri impegni e di «tenere insieme» bisogni e prospettive di benessere e di futuro per tutte le generazioni e dei due generi che le compongono. Assisteremo, quindi, inevitabilmente ad un appesantimento ulteriore di carichi già insopportabili per le famiglie, in cui entrano redditi appiattiti dalla mancata crescita, dal progressivo divario distributivo e, da ultimo, falcidiati dalle casse integrazioni. Famiglie in cui un'intera generazione rimane a carico ben al di là del termine anagrafico per cui sono previste quelle agevolazioni fiscali, perché in tre anni di interventi devastanti sul diritto del lavoro (da ultimo l'incommentabile intervento dell'articolo 8 che vuole pervicacemente conservare quale definitivo stigma di approccio al lavoro quello dell'ingiustizia e dell'iniquità) nulla si è fatto per cambiare la condizione di milioni di giovani, esclusi dai parametri minimi di civiltà che l'accesso al lavoro retribuito deve garantire. Parliamo di famiglia in cui le donne, definite da autorevoli Ministri di questo Governo «secondo reddito» e «ammortizzatore sociale» *(Applausi della senatrice Finocchiaro)*,sono sempre più spesso costrette a scegliere di rinunciare al lavoro, perché da esso deriva un reddito non conveniente se rapportato all'aggravio di fatiche e di costi di cui debbono farsi

fin dall'inizio della legislatura: intervenendo con esclusive finalità di cassa sull'aumento dell'età pensionabile. Siamo ormai stremate dal ripetere che questo Paese spreca una risorsa fondamentale per il suo sviluppo non investendo in maniera piena e convinta nella partecipazione al lavoro delle donne, di tutte le donne. Siamo stanchi di ripetere che un intervento sul sistema previdenziale destinato esclusivamente a fare cassa, che non tenga nel contempo insieme il parametro della sostenibilità, per il sistema e per le persone singolarmente prese,

non può essere fatto se si nega alla radice la necessità della coesione sociale praticata attraverso la ricerca di patti trasparenti e attraverso il loro rispetto. La collaborazione e la solidarietà non possono essere invocate in modo ipocrita a copertura di responsabilità che questo Governo non è stato e non sarà in grado di assumersi. Non si può chiedere (non già alle opposizione, ma ai cittadini) di sostenere sacrifici ingenti e durevoli se non si ha il coraggio della verità e la coerenza dell'esempio. È questo ciò di cui questo Governo non è stato e non sarà capace. Signor Presidente, come tutti sappiamo, il nostro Paese, ormai da troppo tempo, si dibatte in una grave crisi economica, oltre che istituzionale. Dopo lo sforzo che ci ha consentito di entrare nell'euro un decennio fa, siamo tornati ad un livello del rapporto tra debito e PIL non più sostenibile. Le notizie di questi giorni riguardo l'andamento dei mercati sono sempre più preoccupanti e il timore di un brusco peggioramento della crisi economica ha affondato le borse europee, soprattutto quella italiana. I mercati, che temono l'arrivo della recessione, ancora non vedono all'orizzonte strategie per la riduzione dei debiti sovrani per i Paesi più a rischio dell'area dell'euro tra i quali, purtroppo, il nostro è uno dei principali. Le due manovre, di luglio e di agosto, si sono rese necessarie per rispondere ai gravi rischi emersi sui mercati finanziari, ma da questi provvedimenti emerge, purtroppo, un atteggiamento di politica economica del Governo italiano confuso e non ispirato a impostare riforme strutturali.

debole e inadeguato. Una manovra squilibrata sulle entrate che non contiene adeguate misure per la crescita e lo sviluppo. Siamo di fronte ad una manovra che intende fornire ad un malato grave una medicina che ha soltanto un effetto placebo, come se il medico non sia in condizione, o non sappia o non voglia somministrare delle terapie, mediche o chirurgiche, più adeguate e più proprie. Persino sulla lotta all'evasione fiscale non ci sono certezze su tempi e cifre. Questo Governo ha perso, ancora una volta, un'occasione significativa per dare un segnale concreto agli italiani sull'abolizione delle Province, per esempio, e solo il temuto intervento delle decisioni della BCE ha fatto presentare all'Esecutivo, ormai allo sbando totale, un maxiemendamento - quello su cui oggi siamo chiamati il voto di fiducia - con il quale ci vengono proposte altre tasse (mi riferisco all'aumento dell'IVA e al contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 300.000 euro). Signor Presidente, siamo evidentemente di fronte ad un provvedimento delle occasioni perdute, una manovra che non contempla investimenti né tagli, che non aiuta lo sviluppo delle nostre imprese e che tassa sempre di più gli italiani, di più gli italiani, al di là degli impegni di non mettere le mani nelle tasche degli italiani. In questo contesto così negativo, l'UDC ha tenuto fino in fondo un atteggiamento di grande responsabilità e coerenza per tentare di migliorare il testo, senza ostruzionismi, proponendo ad esempio in Commissione bilancio una modifica all'articolo 81-*bis* del codice con la quale si sarebbe finalmente avuta una tangibile velocizzazione del processo civile, in quanto si sarebbero responsabilizzati di più i giudici, gli avvocati e i consulenti e sarebbe stato più difficile usare tattiche dilatorie. Questo, con un evidente, reale risparmio di tempo e di denaro pubblico. Anche queste sono le riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno per crescere. Tuttavia, bisogna mettere al centro come obiettivi primari per la crescita economica anche l'equità sociale e e distributiva, le garanzie per la famiglia, l'equità fra giovani e anziani, l'equità fra donne e uomini e soprattutto una maggiore attenzione alle famiglie e alle fasce più deboli. Una manovra di sole tasse ha vita corta per i mercati, per la Banca centrale europea ma soprattutto dimostra la vita corta e il respiro breve che questo Esecutivo ha, in special modo nei confronti del Paese. Per questi motivi, l'UDC, senza ostruzionismo e con quel grande senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato la sua situazione politica**,** esprime ora ed esprimerà oggi pomeriggio in sede di dichiarazione di voto un giudizio negativo su una manovra che noi purtroppo dobbiamo constatare come essere, per l'ennesima volta, improvvisata ed insufficiente.

Questa estate che si avvia a conclusione è stata molto turbolenta dal punto di vista dei mercati finanziari, ma aggiungo anche dal punto di vista politico: bisogna osservare che

generale: le difficoltà del presidente Obama nel far approvare il *budget* dal proprio Congresso sono forse la testimonianza più emblematica

Il primo riguarda il fatto che l'euro senza politica ha mostrato ancora una volta la sua contraddizione di origine,

Il secondo aspetto, che si affianca a questo, è che l'Italia vive un *deficit* di autorevolezza come Paese; *deficit*

questo *deficit* di autorevolezza produce la mortificazione dei punti di forza che in Italia esistono, che ci sono ma di cui poco si parla: una mortificazione che

Ci sono poi importanti provvedimenti di riforma su cui si sta avviando la discussione nelle Commissioni parlamentari, e noi dobbiamo sempre avere un'attenzione d'insieme e di contesto. L'euro senza politica chiama il pareggio di bilancio. So che attorno a questa discussione ci sono punti di vista diversi dentro le forze politiche e tra le forze politiche. L'interrogativo che ognuno di noi si pone è: in una situazione di crisi come si fa a vietare che si possa ricorrere a un debito garantito per fronteggiare e per mettere in atto una politica anticiclica?

A noi serve che l'*eurobond* diventi una realtà il più presto possibile. questa decisione va presa con tutti i sigilli che la rendono credibile e soprattutto affidabile per chi ci osserva, perché dietro questa decisione c'è un aiuto alla battaglia perché l'*eurobond* diventi una realtà.

corra un serio rischio di *default*: è un Paese troppo grande. Mi viene in mente l'esempio delle grandi aziende sostenute dalle banche non possono farle fallire. Forse è un esempio sbagliato, ma penso che le difficoltà che in questa condizione stiamo attraversando dipendano dal fatto che il debito che costa di più produce un arretramento del sistema economico e degli investimenti. Se in Italia costa tutto di più, ovviamente la stagnazione nella quale siamo immersi rischia di essere un fenomeno

i tre quinti del mandato, ma non abbiamo visto nessuna riforma degli assetti istituzionali. Si è affermata sempre più una politica centralista, nonostante i leghisti abbiano attaccato delle targhe in qualche edificio del Nord per dire che avevano aperto i Ministeri. Per di più, è prevalso il modo peggiore per fare le riforme, perché, quando le riforme si fanno attraverso provvedimenti correttivi della spesa, come sta accadendo con il provvedimento all'ordine del giorno, e tutto il sistema della cosiddetta Italia federalista soffre in soli due anni una riduzione di spesa di quasi 30 miliardi, vorrei capire vorrei capire chi ha il coraggio di continuare a parlare di una riforma verso il federalismo. Non solo: il taglio orizzontale si abbatte su tutto, quindi su ciò che è utile come su ciò che è inutile. Lo abbiamo ripetuto alla noia.

l'emendamento del relatore ha trasformato i Comuni fino a 1.000 abitanti in associazioni Pro Loco. Sostanzialmente, il sindaco è come il presidente della Pro Loco: non decide, non si occupa più di nulla, e tutte le funzioni amministrative sono delegate all'unione. Può essere una scelta sulla quale ci misuriamo, ma attenzione, va fatta una distinzione: un conto è un Comune fino a 1.000 abitanti in aree dense di popolazione e bene infrastrutturate, altra cosa è un Comune fino a 1.000 abitanti in territorio montano o scarsamente popolato. Non è uguale fare un'unione di Comuni in un luogo e nell'altro nello stesso modo. Infine, il tema del federalismo, che è riecheggiato più volte. Noi siamo riusciti, con una iniziativa *bipartisan*,

e non debbano concorrere come le altre Regioni allo sforzo che il Paese nel suo insieme sta facendo, ma semplicemente perché è necessario discutere aprire una relazione. Ed è la stessa accusa che viene dalle Regioni ordinarie, che si sentono mortificate da un Governo che aveva iniziato la legislatura dicendo che avrebbe cambiato il Paese attraverso una pluralità di soggetti, ignorando però del tutto la riforma del Titolo V della Costituzione,

soffermiamo su cose marginali, ignorando l'effetto coesivo necessario. Concludo, Presidente. Per tutte queste considerazioni e per altre che sono state fatte da chi mi ha preceduto, in particolare contenute nella relazione di minoranza, capace di contrastare con efficacia i tentativi sempre attivi, anche nel contesto europeo, di governare la crisi del modello di crescita che i Paesi occidentali hanno conosciuto fin qui, scaricandone il peso in modo sbagliato, perché non equo tra i diversi Paesi. Questo è quello che sta accadendo, e quindi serve un Governo autorevole perché prevalga una linea diversa. Chi vive soprattutto di finanza è in crisi forse più di noi

La fiducia che manca in questo momento nei confronti dell'istituzione, nei confronti del Governo, la ritroveremo solo con un altro Governo, capace di produrre quella coesione necessaria che serve perché l'Italia sia una protagonista attiva, al pari degli altri Paesi, in

una decisione diversa, come quella che è stata presa o portata avanti da altra parte politica, che secondo noi rappresenta il peggio, non sarebbe ben posta. Ma questo non significa che noi siamo il meglio.

contributo alla politica economica del nostro Paese. In questo senso dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. La mia critica è che questa non è una manovra anticiclica.

Tra le manovre che si stanno realizzando oggi in Europa, quella migliore e di maggiore successo sarà certamente quella francese, perché è anticiclica. Non lo è quella spagnola, non lo è quella tedesca, non lo è quella italiana. infatti, un *mix* di interventi che vanno dai tagli alle minori spese, ma non c'è niente che rilanci la congiuntura: c'è molto poco, ben poco. Qualche emendamento in tal senso è stato introdotto e qualche

il raggiungimento dei mancati risparmi, oltre ad essere coperto dalla Robin *tax,* avrebbe potuto essere coperto dal FAS; avrebbe significato cioè che le deliberazioni

Questo è stato ottenuto, ma contemporaneamente non c'è nessuna certezza che questo accada. Infatti, contemporaneamente, avendo mirato alla competenza non abbiamo la sicurezza della cassa. E c'è una cosa di cui ci dobbiamo rendere conto: non possiamo fare l'errore dei tedeschi, i quali hanno voluto varare delle manovre rivolte al rigore della spesa, ai tagli, e si sono ritrovati con un PIL che negli ultimi tre mesi non è cresciuto affatto. Abbiamo introdotto nella ricerca del rigore il teorema inverso a quello che in economia si usa per spiegare la domanda e l'offerta raccontando la favoletta dell'isola con dentro la miniera d'oro: ma se l'isola è deserta avere la miniera d'oro non serve a nulla. Così noi abbiamo la miniera d'oro, la miniera d'oro, ma la stiamo chiudendo. Ragion per cui con un'offerta notevole di prodotti vendibili, avendo chiuso la miniera d'oro non abbiamo l'oro per poter comparare e sviluppare la domanda;

la loro struttura dello Stato, con un «re» di Francia eletto per tutto il periodo presidenziale, stanno riuscendo a varare delle manovre

di Maastricht perché la loro capacità e la loro autorevolezza sono salvaguardate dalla forma di Stato e della forma di governo. E ritorniamo sempre lì, ad una scarsa capacità di rappresentanza e a delle manovre che vengono varate più per essere comunicate che per la loro azione. ricordare che i grandi Governi non dicono le cose che debbono fare ma la fanno. Noi abbiamo cominciato a parlare delle cose che dovevamo fare sotto Ferragosto. Abbiamo fatto diventare

un errore di comunicazione, visto che le feste che a quel punto si sarebbero potute eliminare erano soltanto tre. Il Ministro a Cernobbio ha detto che non se ne era accorto. No, non è che non se ne fosse accorto, in quanto gli era stato detto da Casini e Bersani - tanto per non citare la nostra parte - ma non ne ha tenuto conto, perché la politica in quel momento ha ritenuto di volersi riscattare dalla propria capacità dalla propria inefficienza, comunicando le cose da fare e cominciando a parlare di quelle che, l'abbiamo visto, sono state giudicate dal mercato non di riscatto rispetto al mancato perseguimento del rigore che la politica della nostra parte aveva fatto

l'articolo 8 dove è scritto «nel rispetto della Costituzione». Tutti sappiamo che, quando si scrivono le leggi e i decreti, all'inizio si mette «vista la Costituzione». Quindi, scrivere all'interno dell'articolato «nel rispetto della Costituzione» non capisco che cosa significhi.

Signor Presidente, intervenire in discussione sul testo del cosiddetto maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, offrendoci finalmente la dimensione compiuta di questa ulteriore manovra per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, vuole essere il segno di una responsabilità di ruolo in un periodo di così palese confusione istituzionale, del quale è auspicabile la fine, con il ripristino di modalità di rapporti politici e di comunicazione più consone alla gravità della situazione. Di questo dobbiamo in quest'Aula, credo, preoccuparci: la informazione fra Governo e Parlamento è stata ed è completa e veritiera? La comunicazione alle italiane e agli italiani è stata ed è altrettanto corretta e veritiera? Noi qui rappresentiamo il popolo che, in larghissima parte, non è composto di accademici, di economisti, di analisti finanziari e nemmeno di ricchi. Incombe quindi su chi governa il grave compito della verità. L'indecoroso susseguirsi di dichiarazioni, smentite, azzardi e quant'altro, al quale, impotenti, abbiamo assistito in queste ultime tre settimane ha conseguito il risultato di un palese declassamento (purtroppo ulteriore) della credibilità italiana nel multiforme scenario internazionale e di una diminuzione del ruolo del Parlamento e -in questa occasione - proprio del nostro Senato, che si è con grande diligenza impegnato nella redazione dei pareri da parte delle diverse Commissioni; poi nelle necessarie audizioni e quindi nella elaborazione, discussione e votazione di emendamenti nella 5a Commissione, per approdare in Aula in questo modo. Ma, soprattutto, il comportamento della classe politica di governo in queste tre settimane ha contribuito a disorientare la cittadinanza: o la situazione è veramente grave, ed allora occorre che, con un recupero di senso della responsabilità istituzionale lo si dica, lo si espliciti con evidenza di dati e prospettazione delle questioni e si chiamino tutti al necessario, ma equo, sacrificio; oppure la situazione non è veramente grave: ma allora ci si evitino le penose esibizioni dei troppi che sono intervenuti a proporre correzioni ad un testo che, per essere stato decretato d'urgenza, una qualche motivazione e interna coerenza avrebbe pur dovuto manifestare di per sé. Ad un Paese che sta vivendo oltre le proprie possibilità e alla sequenza di soggetti pubblici, statali e locali che stanno spendendo più di quanto possano, occorre forse che il Governo attualmente in carica dica che non si può andare avanti così e proponga modifiche radicali nei comportamenti effettivi e quotidiani, anzitutto della classe politica (dobbiamo recuperare Già questo però è difficile, direi impossibile da accreditare a chi non ha dimostrato capacità selettive nei cosiddetti tagli da tre anni a questa parte. Ma peggio è per ciò che viene pervicacemente evitato: offrire, cioè, una prospettiva di futuro ai giovani. Ma veramente questo potrebbe essere, fra gli altri, l'obbiettivo dell'articolo 8? Non solo precarietà assoluta, ma consegnare un destino all'arbitrio dei titolari di aziende piccole e piccolissime, dove la tutela sindacale può faticare ad esprimersi. Del resto, abbiamo presente la situazione odierna? O facciamo finta di non sapere lo stato di vera prostrazione dei diplomati e dei laureati costretti a scelte di sussistenza, demotivanti per il percorso già compiuto e frustranti verso la formazione di una famiglia e - quindi - un consolidamento di vita? E tutti i giovani che si danno per vinti ancora prima, senza completare gli studi e senza cercare lavoro? Cosa c'è per i nostri giovani in questa manovra? Nulla. Dobbiamo fare cassa, dobbiamo tutelare un elettorato potenziale, salvare il salvabile di un percorso di governo che in questi tre anni si è sempre più arroccato attorno ad un Presidente del Consiglio a sua volta ripiegato sui suoi interessi, sui suoi svaghi, sulla sua autostima, sul suo sostanziale disinteresse per l'Italia. Ecco perché, in questo momento che riteniamo essere veramente drammatico, assolviamo con dignità al nostro ruolo parlamentare. Erano presenti altre proposte molto incisive, che potevano essere integrate nella manovra e sono state neglette perché provenienti da un'opposizione che pure ha preso molto seriamente atto della crisi. Doveva essere detta alle italiane e agli italiani un'amara verità e si è preferito riferirsi solamente al quadro di crisi internazionale. Occorreva agire con equità, esplicitando una necessaria gradualità nell'imposizione fiscale di vario tipo attivata in questa emergenza e si è scelto invece di aumentare qua e là, di colpire qua e là. Non c'è niente da fare: piaccia o non piaccia, sono i ricchi che devono pagare di più. E questo - in manovra - non c'è strutturalmente. Soprattutto, in questa emergenza, insieme a tanto chiedere alle italiane e agli italiani, occorreva inserire in manovra anche un dare. I tecnici e i mondi economici dicono che mancano elementi strutturali per la crescita. Mi permetto di dire che mancano elementi di fiducia, di positività, di sguardo al futuro: ma questo non si può proprio chiedere a un Governo e a una maggioranza che sono privi di visione strategica per le nuove generazioni e per il sistema Italia. Per questo, il voto sarà conseguente al giudizio.

un passaggio delicato, anche controverso, che ha trovato comunque una lodevole intesa tra i parlamentari di entrambi i Gruppi (in realtà possiamo dire di tutti i Gruppi), nello spirito di salvaguardare il patrimonio

Alludo all'articolo 19-*bis*, che è stato inserito sia nell'emendamento presentato in Commissione bilancio, sia ora in questo nuovo emendamento: si tratta delle disposizioni finali che, appunto, riguardano le Regioni a statuto speciale e le due Province autonome. Potrebbe apparire persino pleonastico dover ribadire ogni volta che una legge dello Stato viene applicata nel rispetto delle autonomie speciali. Va sottolineato, come dicevo in precedenza, che non c'è nessuno spirito particolaristico o difensivistico in questo, ma soltanto il tentativo di ricordare che le autonomie regionali e quelle delle due Province autonome di Trento e di Bolzano non sono privilegi, come a volte qualcuno vuole lasciare intendere o ironicamente afferma, ma rispondono a normative con rango costituzionale: per modificare la disciplina che riguarda l'attività e le funzioni di queste due Province autonome, oltre che delle Regioni a statuto speciale, occorre modificare la Costituzione. Anche in questo passaggio, ringrazio il Governo, che ha saputo aprire un dialogo per evitare *a posteriori* sgradevoli ricorsi, che avrebbero potuto anche portare ad un blocco di tutta la manovra, chiaramente con un grave disagio e con un altrettanto preoccupante svantaggio per tutto il Paese. Il dialogo ha consentito di inserire invece questa clausola di salvaguardia delle prerogative autonomistiche delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, che consente loro di negoziare ora con il Governo posizioni indubbiamente diverse non privilegiate, ma semplicemente diverse - rispetto alle altre Province. L'intento principale, signor Sottosegretario, era quello di ricordare che il Patto di stabilità esiste per le due Province autonome di Trento e di Bolzano dal 2009, anno nel quale a Milano fu stipulato un accordo tra le due Province autonome e il Governo per aprire una fase di contributo per la riduzione delle spese dello Stato in termini di minori erogazioni, ma anche di aumentate competenze, che hanno prodotto tra l'altro un onere annuale per ciascuna di tali Province di 528 milioni di euro, che sono pagati dal 2010 sia da Trento che da Bolzano e saranno pagati ancora per un paio d'anni: si tratta, in particolare, di 320 milioni come rinuncia alla somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, 280 milioni come rinuncia sulla cosiddetta quota variabile, e di 100 milioni in termini di assunzione di nuove funzioni finora a carico dello Stato e ora delegate alle due Province. Tenendo conto di altri passaggi, che vi risparmio per non rendere troppo indigesto il mio intervento richiamando troppi numeri, diciamo che questo contributo di solidarietà si trasforma in 923,8 milioni in un anno. equivale al 27 per cento del bilancio del Trentino del 2010, esclusa la parte riguardante la sanità; se si inserisce poi anche la sanità, che in Trentino e in Alto Adige è competenza diretta delle due Province autonome, la quota di rinuncia è pari al 20 L'intento ed il comune impegno dei parlamentari di queste due Province nel ricordare al Governo questa posizione era solo quello di chiedere quando da adesso in poi si incomincerà a negoziare la quota ulteriore con la quale le due Province, che non si sottraggono all'impegno nazionale, dovranno contribuire, ci si ricordi che esiste già questo impegno e che sono già state pagate delle somme. Quindi, non è che le due Province di Trento e Bolzano invochino lo statuto speciale delle autonomie come grimaldello o *escamotage* per non sobbarcarsi una certa parte di onere per la riduzione del debito complessivo, ma vogliono solo rammentare - ma il Governo sicuramente non lo ha dimenticato - che sono già impegnate in quest'azione da almeno un paio d'anni. Non è facile parlare di queste di queste due Province come anche delle Regioni a statuto speciale davanti a tanti colleghi che vivono in Regioni a statuto ordinario, dove sappiamo che le condizioni di vivibilità sono magari meno facili.

un impegno ulteriore, una grande responsabilità. Le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza diretta ed esclusiva su molte materie che per le altre Regioni ancora sono deleghe dello Stato. Hanno una competenza che significa soprattutto rispondere ai cittadini dell'efficienza, dei costi di servizi che appunto in altre Regioni sono addebitabili all'organizzazione generale dello Stato. Quindi, ripeto ancora una volta che non è che si tenda ad essere diversi o peggio ancora unici, unici, come a volte potrebbe apparire, ma soltanto a ricordare che questa particolarità, legata ad un patto originario fra De Gasperi e Gruber, deriva dal fatto che nella nostra Regione convivono, ora fortunatamente in maniera pacifica, etnie diverse, situazioni particolari che anche a livello internazionale hanno, e rivendicano e ottengono delle valutazioni differenti rispetto alle altre Regioni. Tutto questo ha un costo un costo che le due Province sanno sobbarcarsi grazie alla responsabilità con cui finora in questi oltre cinquant'anni di storia hanno saputo interpretare in senso politico la delega amministrativa e democratica dello statuto speciale di autonomia. Grazie ancora al Governo perché anche in questa circostanza ha ribadito che questa responsabilità, oltre ad essere garantita dalla Costituzione, finora è stata saggiamente interpretata da parte di coloro che hanno retto i destini amministrativi e politici di queste Regioni e non hanno un colore politico perché in questo concorre sicuramente la responsabilità di tutti, indipendentemente e al di là dei partiti. che è nata una filosofia, una forma mentale: sapersi amministrare in maniera autonoma e saper distribuire saggiamente le risorse nel nome di tutti. Direi che potrebbe essere un cartello da indicare per ogni spinta di tipo federalista.

dopo l'annuncio del voto di fiducia. Porre la fiducia in questa occasione è stato particolarmente grave e ha contraddetto tutti gli impegni alla collaborazione assunti da questo Governo e dalla maggioranza in sintonia con le ripetute raccomandazioni del Capo dello Stato. Ancora una volta si calpestano i diritti del Parlamento. Questa non è una novità per questo Governo. Se non che, queste sono giornate di portata storica, gravide di conseguenze per il futuro dell'Italia e dell'Europa, così come le decisioni che prenderà questo ramo del Parlamento, che avranno un effetto sull'economia e potrebbero rappresentare veramente un pericolo reale in ordine all'impoverimento di tanta parte della popolazione, così come è avvenuto dopo una successione di manovre e come vediamo - ahimè - in Grecia. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico dopo l'enorme lavoro di agosto in Commissione bilancio (a questo proposito mi lasci dire che sono veramente molto sorpresa, senza nulla togliere alla presenza qui del sottosegretario Giorgetti, che segue sempre i lavori della Commissione bilancio, che questo dibattito non sia stato seguito da un Ministro di questo Governo), era pronto ieri a venire in Aula, rendendo essenziali i nostri emendamenti. Lo abbiamo fatto anche in Commissione bilancio, dove la maggioranza e non l'opposizione si è presentata divisa al suo interno e con oltre 700 emendamenti al decreto. Gli appelli accorati al senso di responsabilità e al superiore interesse del Paese del presidente Napolitano per noi del PD sono stati una guida per l'azione. Nella nostra condotta parlamentare li abbiamo tradotti in proposte essenziali, che mettevano al centro obiettivi di rigore e disciplina di bilancio, insieme alla elaborazione di quelle proposte di riforme che ci caldeggia l'Europa e liberalizzazioni per la crescita e per l'occupazione, sempre nel segno dell'equità e di una ripartizione dei sacrifici che innanzitutto faccia pagare chi non ha mai pagato e abbia rispetto per i più deboli. Signor Presidente, tutto questo nostro contributo è stato vanificato dalla maggioranza e dalla richiesta della fiducia e dal maxiemendamento del Governo. È bene che il presidente Napolitano sappia tutto questo. Con un colpo di mano la manovra è stata ancora una volta cambiata, aggiungendo confusione a confusione e negando al Parlamento la possibilità di dire la sua. Tutto questo è molto grave. Ci sarebbero state tutte le condizioni per rafforzare questa manovra, così come ha chiesto il Presidente della Repubblica, con una imposizione sui grandi patrimoni. Questa proposta, che è stata presentata con un emendamento del Partito Democratico, è una proposta largamente condivisa nella società italiana, è una proposta in maggioranza. In minoranza è la posizione del Governo. Non è una proposta solo della sinistra. Questa proposta avrebbe anche potuto consentire di eliminare la prospettiva di aumento dell'IVA e orientare invece il risparmio fiscale, così come tante volte ci ha suggerito Bankitalia, in direzione della riduzione della pressione fiscale, che oggi ha superato il 45 per cento, in particolare orientandolo al cuneo fiscale sul lavoro. Un provvedimento di questo genere avrebbe avuto una ricaduta certa sulla crescita. Invece la manovra, alla sua quarta versione, quella di oggi con fiducia, prevede l'IVA al 21 per cento, un contributo di solidarietà del 3 per cento per i redditi superiori a 300.000 euro e un anticipo al 2014 dell'aumento dell'età di pensione per le donne Sull'aumento dell'IVA, non è tanto la sua proiezione depressiva e inflazionistica sui consumi ad interessarmi in questo momento, quanto piuttosto le sue implicazioni in ordine alla delega fiscale e assistenziale. Ne ha parlato poc'anzi anche la senatrice Ghedini: i complessivi 20 miliardi di euro che dovrebbero essere recuperati in tre anni attraverso la riforma fiscale ed assistenziale sono evidentemente un obiettivo del tutto irrealistico (in tal senso era stata prenotata in qualche modo l'IVA). Si prefigura in realtà un drammatico taglio sul sociale, con conseguenze molto gravi; o viceversa, se scattasse la clausola di salvaguardia, un azzeramento di tutto il sistema delle agevolazioni, che si scaricherebbe anche questo ancora una volta sulle fasce più deboli del Paese, esasperando ulteriormente l'effetto depressivo e recessivo della manovra. Parliamo - lo diceva la senatrice Ghedini - di assegni familiari, di prestazioni per maternità, di assegni sociali d'integrazione al minimo pensionistico, parliamo cioè delle fasce più deboli della nostra società. Ecco allora chiarito, una volta per tutte, chi è che dovrà pagare i costi sociali di questa manovra. E quando si tratta di tagli di questa portata dobbiamo sapere che a livello territoriale è il Sud che paga il prezzo più alto: un prezzo che il Meridione d'Italia ha già pagato, e salato, appena mitigato dall'accoglimento, in Commissione bilancio, dei nostri emendamenti per sottrarre i FAS regionali dal finanziamento dei Ministeri centrali, mentre resta ancora del tutto irrisolto il tema di cui tanto si è discusso del finanziamento degli investimenti nel Mezzogiorno, anche di quelli già progettati e deliberati sul territorio utilizzando i fondi europei ma in realtà bloccati dalle regole del patto di stabilità, che insistono anche sulle quote di cofinanziamento degli enti locali. È questo un tema cruciale che il maxiemendamento del Governo affronta solo dal punto di vista ordinamentale, senza in realtà prevedere alcun finanziamento. In realtà si tratta di decidere se aprire qualche spiraglio e una prospettiva di crescita, consentendo di impiegare legittimamente i fondi europei che sono dedicati al Sud o viceversa condannare definitivamente all'impoverimento vaste zone del Paese e fasce amplissime della popolazione italiana. È una risposta che il Governo fin qui non ha dato e che invece deve dare alle popolazioni meridionali, insieme a molte altre a proposito di settori strategici (a cominciare da quello dei trasporti, dove ha operato con tagli che sono rilevantissimi e senza nulla aver previsto per il trasporto pubblico locale) piuttosto che di politiche per l'occupazione, che mancano del tutto, lì dove (e penso alla mia Regione, la Campania) si stanno vivendo drammatiche crisi occupazionali, come quelle di Alenia, Fincantieri e Fiat Irisbus, che stanno gettando nella disperazione migliaia di famiglie, intere comunità e città, come Castellammare e Avellino. Questa manovra pessima, sbagliata, ingiusta rischia di essere il punto di avvio di una tragedia sociale, che nel Mezzogiorno troverà il suo epicentro, ma che non si fermerà al Mezzogiorno. Per finire, e come ultima provocazione a chi tanto ha già pagato fino ad ora il prezzo della crisi, il Governo ha voluto pensare e dedicarsi alle donne. Come senatrice di opposizione, ma ancora prima come cittadina e lavoratrice dipendente del settore privato, io mi sento offesa dalle parole che nei giorni scorsi il ministro Brunetta ha rivolto alle donne. Il Ministro, per caldeggiare la proposta di equiparare l'età pensionabile ed innalzare l'età pensionabile delle donne del settore privato, non ha trovato argomento migliore di quello che si poteva fare perché tanto si era già visto che innalzare l'età pensionabile per le donne del pubblico si era fatto in due giorni e in due anni si era portata a 65 anni senza un'ora di sciopero, garantendo che anche le donne del privato avrebbero fatto la stessa cosa. È una schifezza! Come se i diritti delle donne potessero essere pesati sulla base delle ore di sciopero e, comunque, pesino di meno i diritti delle donne di quelli degli uomini o di chiunque altro. Si tratta di una provocazione inutile, una provocazione sbagliata dopo avere escluso interventi sulla previdenza, come quello, altrettanto sbagliato, dell'annullamento del riscatto degli anni di laurea e del servizio militare. La verità è che anziché operare considerando l'equilibrio e la sostenibilità del sistema pensionistico, in tre anni - lo voglio ricordare - sono stati fatti ben dieci interventi sul sistema previdenziale, di cui il più rilevante sulla previdenza delle donne del pubblico, senza risolvere nessuno dei problemi di fondo del sistema, e prima di tutto quello che riguarda l'assenza di prospettiva previdenziale per i giovani precari, e senza restituire nulla del risparmio previdenziale al sociale e alle donne, così come la legge prevedeva. Anche sulla previdenza si può e si deve fare di più e si deve fare meglio. costruendo da subito e per tutti, uomini e donne, il passaggio al contributivo. In questo contesto, anziché ragionare in chiave restrittiva per le donne e di taglio di diritti e di benefici, si dovrebbe restituire flessibilità a tutte le persone, uomini e donne, nella scelta del pensionamento, e premiandole in modo adeguato se decidono di continuare l'attività. Ma, per far questo serve dialogo sociale, capacità di fare coesione, serve ascoltare i sindacati e le proposte delle opposizioni. Quello che non serve sono i Ministri scassatori: non è il loro tempo; l'Italia non ha bisogno di loro. E per le donne serve rispetto politico e sociale, perché le donne continuano ad essere il pilastro fondamentale del sistema sociale, facendosi carico di compiti che altrove sono svolti dalle strutture pubbliche, con effetti enormi sulle ore di lavoro che gravano sulle donne stesse. donne stesse. Invece, la maggioranza ha respinto in Commissione bilancio persino un emendamento che non costava proprio niente, ma che aveva un grande significato: quello che avrebbe ripristinato una legge, già approvata dal nostro Parlamento, con la quale s'impediva ai datori di lavoro di ricattare le neoassunte obbligandole a firmare le dimissioni in bianco da utilizzare in caso di maternità. Una legge cancellata nel 2008, il primo atto di questo Governo, perché, spiegò allora l'ineffabile ministro Sacconi, di burocrazia si muore. Non ci sono parole, signor ministro Sacconi. Ha ragione Susanna Camusso: il Paese non merita questa manovra, era possibile farne un'altra più giusta, più equa e chi ci ha portato fino all'orlo dell'abisso deve fare una cosa sola: fare un passo indietro, o forse un passo in avanti, ma senza portare nell'abisso il Paese tutto intero.

si era parlato della norma cosiddetta manette agli evasori, alcuni giornali avevano pubblicato la notizia la notizia che, tra le diverse questioni che riguardano il nostro Presidente del Consiglio, vi era anche quella di una contestata evasione per 16 milioni di euro, cifra abbondantemente al di sopra della soglia individuata di 3 milioni di euro. Ma come: Berlusconi si fa una norma che lo può danneggiare?

le cosiddette manette agli evasori, con la soglia dei tre milioni di euro, ossia faccia feroce a chi evade più di tre milioni di euro

prevedeva che «qualora l'imposta evasa non versata sia superiore a tre milioni di euro non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena»;

«per i delitti previsti (...) l'istituto della sospensione condizionata della pena non trova applicazione

rimediato a quell'imperdonabile errore che esponeva Berlusconi ad una condanna a pena non sospesa. È stato subito trovato il rimedio. milioni di euro, oltre ad un altro elemento che congiuntamente deve concorrere per escludere l'applicazione della sospensione della pena e cioè che comunque l'evasione 30 per cento del volume di affari. Questa è una norma che premia i grandi evasori;

perché chi evade ruba - «non ha diritto a benefici di legge». Noi avevamo proposto una norma diversa.

che doveva essere affrontato, e viene affrontato. Si afferma che si possono accorpare i tribunali ricorrendo a criteri oggettivi: dimensionamento, sopravvenienze, distanze chilometriche, bacino di utenza e così via. Vi sono criteri oggettivi inseriti nella delega, se non fosse nella delega è prevista la possibilità di accorpamento degli uffici di procura senza individuazione di criteri oggettivi, cioè senza alcuna indicazione. afferma: «ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti con la possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali». non vi sono criteri oggettivi di riferimento. Ciò significa che avremo tribunali senza procure, perché vi sarà un ufficio accorpante che gestirà più territori, più circondari. Conosciamo per esperienza viva il grande problema delle procure distrettuali che hanno competenza territoriale a livello di distretto di corte d'appello: esse lamentano sempre il problema della presenza sul territorio, ma comunque possono appoggiarsi alle procure della Repubblica. Con gli accorpamenti avremo procure per più tribunali, ossia diminuirà il controllo di legalità sul territorio, quella possibilità di acquisire notizie di reato da parte del procuratore del Repubblica, degli uffici di procura a livello circondariale, e quel rapporto stretto con la polizia giudiziaria. Vi sarà un ufficio accorpante che dovrà gestire anche il resto

malissimo) che l'ufficio di procura accorpante potrà svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Noi sappiamo che gli uffici di procura sono sono cosiddetti bifasici, ossia hanno una fase inquirente ed una fase requirente: la fase inquirente è quella

che l'ufficio accorpante di quei circondari ormai privati da procura possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali pone il problema di chi svolge le funzioni inquirenti; infatti,

Mi auguro francamente che il buonsenso e l'equilibrio del Ministro della giustizia

al tentativo di far soldi prevedendo raccolta da gioco attraverso l'introduzione indicendo nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottando nuove modalità di gioco del lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale. Sappiamo che il prelievo per cento. Prevedere un aumento di un miliardo e mezzo dei giochi significa aumentare di 20 miliardi la raccolta. Negli ultimi sette anni la raccolta da gioco, cioè i soldi presi dalle tasche dei cittadini, è stata di 309 miliardi di euro. Questa è un'altra forma di tassazione. Qui si incentiva la raccolta, nell'ultimo anno per 70 miliardi, e si prevede che bisogna offrire altri giochi, altre occasioni a chi è malato da gioco da gioco per sottrarre quei 20 miliardi da cui verrà poi fuori il ricavo erariale intorno a un miliardo e mezzo. Sono queste tre delle tante ragioni (tre delle quali io mi sarei dovuto occupare) per farci dire no a questa manovra e, quindi, no alla fiducia al Governo.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, finalmente oggi si può parlare di una cosa certa, la cosa più certa della quale parliamo da tempo, cioè della richiesta di fiducia da parte del Governo. Della manovra, invece, forse è bene non dire quasi più nulla, dal momento che tutto quanto è stato detto in questi giorni è stato spesso e volentieri rivisto. Mi ero permesso di fare un esempio, che ha suggerito qualche gesto apotropaico da parte del Presidente della 5a Commissione. Mi sembra, però, che abbiamo lavorato come avessimo un paziente in sala operatoria, per il quale abbiamo prima sbagliato la diagnosi, poi non avevamo le lastre e, infine, abbiamo avuto le lastre sbagliate. Adesso, parliamo della fiducia. della fiducia. Il Governo chiede la fiducia ai parlamentari, ma a me pare che vi sia un problema di fiducia da parte dei cittadini nel sistema governato da questo Esecutivo, che ha la ventura di esprimere la propria responsabilità nel governo del Paese in questo tempo. Tra i molti dati che sono stati pubblicati in questi giorni, sono stato colpito da che avrebbe dovuto suggerire qualche titolo ai giornali, titoli del tipo: ma ci sono i comunisti al Governo? Gli italiani, infatti, nel mese di giugno hanno chiuso conti correnti per 23 miliardi di euro,

nelle cassette di sicurezza alcuni e sotto i materassi altri. Questo la dice lunga sulla fiducia del Paese nelle istituzioni e in chi lo governa. Per tale motivo, diventa imbarazzante parlare di questa cosa certa, cioè della fiducia.

Nella scena centrale, nodale, di quel film, il protagonista, James Stewart, si si pone dietro il bancone di una banca che il cattivo di turno aveva fatto precipitare. Ai cittadini che chiedono di ritirare i soldi, dice che bisogna fidarsi del Paese, che bisogna fidarsi di lui, che in quel Paese era restato anche se avrebbe sempre voluto andare via. Ecco,

penso che avrei dato volentieri la fiducia al Governo del mio Paese se in questo momento quel Governo avesse saputo coinvolgere fino in fondo tutti in in maniera credibile, riconoscendo magari qualche errore per tirare fuori l'Italia da una vicenda così difficile e complicata. Avrei voluto che qualcuno da dietro i banchi

più di una volta ieri nelle piazze italiane. Piacerebbe anche a me interrogarmi su come mai, signor Sottosegretario, anche questa volta si va alla fiducia. Tuttavia, vorrei porre qui l'argomento

Come mai, a fronte di tagli tanto virulenti portati da questa manovra e rivolti a diverse classi sociali, non si è preso seriamente in esame l'emendamento proposto da noi, a prima firma della presidente Finocchiaro, e condiviso dall'Italia dei Valori e dai colleghi del Terzo Polo con un emendamento omologo: con un emendamento omologo: l'opportunità di mettere a disposizione di un'asta competitiva le frequenze per la televisione digitale, quella parte che riguarda il cosiddetto dividendo interno, cioè i *broadcaster* televisivi. In verità, un'asta c'è; è in corso ed è anche molto fruttuosa, per quello che viene chiamato nel gergo il dividendo esterno, ovvero per la parte telecomunicazione. Dai previsti 2,4 miliardi di euro, si sta arrivando ben oltre i 3 miliardi. miliardi. Perché si è scartata una simile procedura per il campo televisivo? Perché si è fatta una scelta chiamata, con una terminologia mutuata elegantemente dal keynesismo (Keynes si rivolterà nella tomba), *beauty contest*, un modo per dire che non si fa un'asta? Uso le parole di un commentatore importante del «Corriere della sera», Edoardo Segantini, di qualche giorno fa: «Il cosiddetto *beauty contest* (concorso di bellezza) per le frequenze televisive è, a dispetto del nome, l'ennesima bruttura italiana nel campo dell'etere». Con lui, tanti altri commentatori e anche tanti gestori, che già hanno fatto ricorso ai TAR e alla magistratura su una procedura assolutamente anomala. L'asta avrebbe portato all'erario pubblico da uno a due miliardi di euro.

che stiamo parlando di cose molto concrete. denaro importante per lo Stato democratico. Perché tutto questo non si è fatto, scegliendo la strada, già prevista tanti anni fa

perché in Italia c'è il conflitto di interessi. Se il Presidente del Consiglio non si chiamasse Silvio Berlusconi, ma in un altro modo, e fosse anche di centrodestra, e non avesse un immediato interesse a non pagare le frequenze per le sue aziende Mediaset, sicuramente avreste fatto l'asta competitiva, perché nessun Governo

Joyce in «Gente di Dublino». Epifania, cioè quel fenomeno che fa apparire chiaro ciò che c'è dietro ed è più grande di quello che la parola stessa dica. È una storia antica. I canoni di concessione televisiva in Italia costano pochissimo. Rinvio alla lettura di un materiale della Fondazione Bordoni, quindi un'entità neutra, del dicembre 2008, dal titolo «*Gli Administered Incentive Prices*».

del ripristino del Fondo per l'editoria. 100 testate rischiano di scomparire il prossimo anno davanti, invece, all'Epifania del conflitto di interessi. Guardate, massimo del del clamore in questa vicenda, che pure fu esaminata dalla Commissione europea e discussa, con un'accesa votazione, dall'Autorità per per le garanzie nelle comunicazioni, a farne le spese sono anche le emittenti locali, che rischiano di chiudere in molti casi la loro attività. rappresentante del Governo, vorrei concludere questo amaro intervento ponendo la questione di fondo: l'Italia può continuare a sopportare un Governo che, persino in una vicenda come questa, mette i suoi interessi, in particolare quelli del Presidente del Consiglio, prima di ogni altro interesse degli italiani? Possiamo avere un sistema radiotelevisivo, che nel passaggio al digitale aveva l'opportunità di cambiare, e che invece rischia di essere peggiore di quello della stagione analogica? Non è più possibile! Andatevene prima che davvero sia troppo tardi.

sommessa, anche se, me lo consenta, intellettualmente appassionata. Tre sono gli assi portanti del pacchetto lavoro della manovra, che si materia principalmente nell'articolo 8. Il primo asse è quello della convinzione secondo la quale le relazioni industriali, che per tutta la storia economica repubblicana sono state zavorra, impedimento e inibizione allo sviluppo competitivo delle nostre imprese, oggi possano possano diventare un formidabile vettore competitivo. Lo dimostra limpidamente la vicenda FIAT, insieme alla vicenda di tante aziende medie, posizionate nei settori tradizionali, a forte innovazione di prodotto, a significativa trazione comunitaria, a marcata propensione all'*export*, che stanno declinando una splendida storia di successi, tanto che in larga parte del Paese oggi abbiamo già recuperato i livelli dell'*export* del 2007, riposizionandoci nei Paesi a più alta densità di sviluppo, nei mercati emergenti. Valorizzando e intensificando l'autonomia delle parti sociali noi non garantiamo soltanto una maggiore coesione sociale, ma creiamo anche le condizioni per agevolare, supportare e sostenere quel colossale processo di riposizionamento competitivo in cui si sostanza la chiave della rinascenza economica del nostro sistema manifatturiero e dei servizi. Oggi la sfida cui tutto il Paese è chiamato è quella di andare a presidiare i segmenti più elevati dei mercati internazionali concentrando il sistema delle proprie competenze distintive sui prodotti, non più sui processi (storico errore dell'industria italiana); prodotti che tanto più significativamente possono ottenere riconoscibilità e remunerabilità in quanto siano espressione di grumi autentici e dispiegati di storie, di esperienze e di verità secolarmente radicate; il che consente loro di diventare a tutti gli effetti compiutamente l'uscio contemporaneo dove quel che conta non è l'esclusività del prezzo, ma l'esclusività della storia incorporata nel prodotto. Ma il prodotto è figliato da risorse umane, da sistemi integrati di intelligenza, esperienza e competenza regolati nella loro vocazione comunitaria da nuove relazioni industriali. Il terzo asse, colleghi, è evidentemente quello della liberazione, dell'affrancamento di giacimenti competitivi che oggi giacciono e che oggi risiedono in contiguità al punto del fare nella compiuta, concreta qualità dell'esperienza competitiva quotidiana delle nostre imprese nei nostri distretti; giacimenti competitivi che non possono essere sfruttati da un modello regolatorio burocratico, centralizzato, malamente e asfitticamente concentrato nella dimensione della prospettiva della legge del contratto nazionale. Serve invece per liberarne le energie. Una prossimità contrattuale data dal contratto aziendale, dal contratto territoriale come nuova, audace dimensione della liberazione competitiva, delle vocazioni delle nostre imprese. Questo, soltanto questo, vuol dire l'articolo 8. Significa dare ai sindacati più rappresentativi la possibilità di modellare e modulare la regolazione contrattuale sulla specificità irriducibile del modello competitivo che si realizzi lì, in quella impresa, in quel territorio, consentendogli di esprimere tutta la sua forza. In Italia, checché se ne dica, nella compiuta catena del valore, il valore del lavoro è ancora il 50 per cento, è governato dal contratto di prossimità. Il resto è prigioniero, occluso da un contratto nazionale che ha esaurito ogni propulsività nella sua spinta. Cito tre esempi molto semplici, ruvidi e franchi sulle deroghe che sono consentite. Parto subito da tre esempi sull'articolo 18, perché non abbiamo nessuna paura a ragionare su questo tema. Se un grande gruppo internazionale farmaceutico si accorge che a Bari c'è un'eccellente facoltà di medicina che produce eccellenti laureati il cui costo, tra l'altro, è del 35 per cento inferiore alla media europea dei laureati in medicina, e decide di portare il suo centro di ricerca a Conversano, o a Ceglie Messapica,

sarà licenziato, e, anche laddove quel licenziamento fosse ritenuto da un giudice non giustificato, può sostituire la fisicità del reintegro, con l'inevitabile disordine organizzativo che esso arreca, con un congruo risarcimento? Oggi per quasi tutti i lavoratori italiani e per quelli delle imprese sotto i 15 dipendenti sono previste due mensilità e mezzo, sei al massimo: può quell'accordo di quella grande multinazionale prevedere 24 mesi di risarcimento? Invece sì, caro senatore Passoni, perché questo rispetta la Costituzione, la normativa europea, ed è in linea con le migliori esperienze internazionali. Questo può essere fatto. E allora, senatore Passoni, le chiedo un'altra cosa, a lei che con me ha governato tanti accordi pieni di sano, vitale e virtuoso pragmatismo. Se una azienda della logistica del meridione,

parasubordinati e pararegolari, a tempo pieno e a tempo indeterminato, potrà negoziare con lei, sindacato maggiormente rappresentativo, che il centoventottesimo di quel gruppo, se non funzionale, se licenziato anche ingiustificatamente per riconoscimento dal giudice, anziché

Parlo della mia Treviso dove, anche nel pieno della crisi, il tasso di disoccupazione è del 5 e mezzo per cento e dove è stato appena sottoscritto, da CGIL, CISL e UIL, un patto con Confindustria per lo sviluppo.

attingendo dalle similari esperienze germaniche e baltiche questa forma di regolazione attiva del mercato del lavoro. Dentro quel patto, per qualunque lavoratore che perda il posto, è previsto un percorso di riqualificazione, di riconversione, di formazione, un percorso di restituzione alla vitalità

Se arrivasse in Italia, per il meccanismo con il quale è costruita la norma sul lavoro ordinario e su quello straordinario, avrebbe grosse difficoltà a implementare quel modello organizzativo, anche se questo fosse accompagnato da investimenti colossali, di decine di milioni di euro. di milioni di euro. Rispettando sino in fondo la direttiva europea, che giustamente l'articolo 8 richiama come non eludibile, la quale prevede 48 ore medie settimanali (straordinari compresi), potrebbe per davvero la compiuta realizzazione dell'equilibrio economico, gestionale ed organizzativo tra la sua tipologia di orari, ideale per quel tipo di investimento in impianti, e la concreta positiva difesa degli interessi dei lavoratori, garantita dalle grandi organizzazioni sindacali. Non affronto neanche i troppo facili esempi, amici e colleghi, relativi all'articolo 4, una norma che è stata fatta nel 1970 quando per la prima volta abbiamo visto a colori sul televisore le partite del mondiale messicano. Credo che sia lecito poter modificare quella piattaforma tecnologica. norma folle, una norma che pietrifica le mansioni. Se una persona vuole fare una ristrutturazione salvando il posto di lavoro degli impiegati e consentendo loro di essere impiegati, giustappunto come

culture e tradizioni che nell'articolo 8 si ritrovano, come la cultura del personalismo cattolico che ha generato l'economia sociale di mercato; o le scelte fondative dell'identità della CISL, come la contrattazione articolata, sin dagli anni Cinquanta. Guardo esponenti del socialismo patriottico e riformista. Guardo esponenti nel FLI, della destra sociale nazionale. Guardo persino, nella sinistra più autenticamente audace, l'esperienza morandiana dei consigli di gestione. Vogliamo davvero e trascurare quindi questa esperienza concreta e compiuta di innovazione solo per assecondare la furia anabattista, fosca e febbrosa della FIOM?

Signor Presidente, la crisi internazionale del 2007, come noto, è stata la conseguenza dell'esplosione di una bolla speculativa nel mercato immobiliare

«non ha dovunque cancellato gli effetti della crisi, né ha eliminato le fragilità che l'hanno determinata»: concetto, questo, espresso dal Governatore della Banca d'Italia. L'Italia, d'altro canto, rispetto ad altri Paesi colpiti dalla crisi, grazie all'azione del Governo che era riuscito nell'obiettivo della tenuta dei conti pubblici, anch'essa subito un rallentamento economico, pur essendo un Paese quasi privo di *asset* tossici o illiquidi e con un basso grado di indebitamento delle famiglie. In sintesi, la crisi del 2007 - una delle più gravi dal 1970 ad oggi - ha evidenziato le carenze del sistema economico europeo e mondiale e la poca trasparenza del mercato dei derivati, che dovrebbero essere sottoposti ad una sorta di tracciabilità che individui l'origine e il percorso di ciascun contratto, tutelando così i risparmiatori e lo stesso mercato. Oggi, ancora una volta, a livello europeo e globale, ci ritroviamo di fronte ad una situazione analoga, caratterizzata da instabilità economica, incertezza e sfiducia nei mercati, calo dei consumi, mancata crescita economica e strutturale. Le cause di questa nuova crisi si possono ricondurre principalmente ai seguenti fattori: speculazione finanziaria, conseguente inadeguatezza dei sistemi di regolamentazione e vigilanza, debolezza delle politiche economiche europee, cali dei consumi e degli investimenti che hanno generato una contrazione del PIL e debiti pubblici elevati. La risposta delle istituzioni europee a seguito della recente crisi del debito sovrano greco, come noto, ha portato, tra l'altro, nel corso del 2010, all'approvazione da parte del Consiglio ECOFIN delle modifiche al codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita correlate all'introduzione del cosiddetto semestre europeo. nel nostro Paese il Governo, con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, approvato dal Senato, ha introdotto importanti e sostanziali riforme in materia di semplificazione burocratica e aiuto alle imprese e ai privati, volte ad avviare politiche di sviluppo e sostegno dell'economia e, quindi, al superamento della crisi decreto sviluppo ha rappresentato un importante tassello per la ripresa economica dell'Italia e il decreto-legge che andiamo ad approvare ne è la naturale continuazione. 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», aveva introdotto significative disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, attraverso la riduzione dei costi della politica, la riduzione delle spese dei Ministeri, la soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici, il contenimento e la razionalizzazione in materia di impiego pubblico e spesa sanitaria e previdenziale e, infine, aveva previsto il pareggio di bilancio per il 2014. Il provvedimento in esame ha proprio lo scopo di superare la crisi, attraverso una serie di interventi tesi principalmente al raggiungimento del pareggio di bilancio già nel 2013. Il testo del provvedimento proposto dal Governo, comprensivo delle modifiche introdotte in Commissione e ulteriormente modificato dal maxiemendamento, presenta norme che per la loro natura dovrebbero anche essere condivise dall'opposizione. Mi riferisco, nello specifico, a quelle in materia di rafforzamento della lotta all'evasione, di riduzione dei costi della politica, di contenimento dei costi della pubblica amministrazione e di riduzione degli oneri amministrativi e procedimentali che limitano la libertà di impresa. In particolare, questo ultimo tema della sburocratizzazione e liberalizzazione per le imprese è la naturale continuazione dell'azione governativa annunciata per l'approvazione della riforma costituzionale di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, contenuta nell'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento. Tale azione di modifica dell'articolo 41, a mio avviso, deve poi essere attuata con leggi ordinarie ed è di fondamentale importanza per il nostro Paese, tenuto conto che le piccole e medie imprese rappresentano la forza trainante e il motore dello sviluppo del sistema economico italiano e che in un periodo economico negativo, come quello che stiamo vivendo, appare necessario eliminare quelle rigidità del sistema economico rappresentate, appunto, dalla burocrazia e dagli oneri connessi, che limitano la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle straniere. In sintesi, risulta chiaro che è imprescindibile la semplificazione amministrativa ed un maggior senso di responsabilità da parte della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire la crescita ed incentivare gli investimenti esteri. Come più volte sottolineato, la riduzione degli oneri burocratici determinerebbe un incremento del PIL, oggi particolarmente in sofferenza. Rispetto al testo originario, inoltre, il Governo ha successivamente e opportunamente introdotto delle modifiche, e tra gli aspetti che mi stavano più a cuore vi erano quelle riferite alla soppressione delle Province e le norme sui Comuni e anche i trasferimenti agli enti locali. Per ciò che concerne le disposizioni sulle Province, per le quali ho presentato un emendamento soppressivo dello stesso articolo, appare doveroso sottolineare la necessità di un progetto di riforma costituzionale per procedere alla loro soppressione, tenendo conto del bisogno di individuare un soggetto sostitutivo, sicuramente più snello, che assolva i compiti delle Province stesse. A mio avviso, la norma soppressiva rischiava di creare negatività, soprattutto per quelle Province caratterizzate da un territorio prevalentemente montano. Inoltre, per ciò che concerne i Comuni, a mio parere, è stata enfatizzata ingiustamente la norma che prevedeva la soppressione di 54.000 poltrone, tenendo conto che il risparmio che ne derivava era veramente limitato; mentre un fattore importante è che le piccole realtà devono essere riorganizzate per ciò che attiene ai servizi, accelerando la costituzione delle unioni, per la gestione comune dei servizi. Le unioni restano essenziali per le piccole realtà, sia per l'applicazione del federalismo fiscale, sia allo scopo di rendere i servizi efficienti, adeguati e celeri ai cittadini. Appare altresì opportuna e voluta da più parti, e da me condivisa, la richiesta di una rappresentanza democratica e non monocratica della piccola amministrazione comunale. In questo senso le proposte maturate mi sembrano giuste, e colgo l'occasione per ringraziare per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti tende, tra l'altro, a cogliere l'esigenza di quelli che intendono attuare la fusione. Tale operazione di fusione, a mio modo di vedere, potrà essere considerata ed attuata esclusivamente attraverso *iter* democratici, come quello del *referendum* a livello comunale, a cui è demandata la decisione in materia. Bisogna sottolineare che, in generale, le proposte dell'opposizione politica, dei *media* e dei diversi esponenti politici qualche volta sembrano essere ricette poco credibili: si pensi, infatti, alle proposte di tassare addirittura i beni della Chiesa, alle proposte di dismissione del patrimonio, i cui esiti già nel passato non hanno dato risultati rilevanti dal punto di vista economico, alla vendita dei cosiddetti gioielli italiani (Cassa depositi e prestiti, Poste e così via), proposte che appaiono inopportune e non tengono conto dell'attuale ridotto valore delle società quotate in borsa. Appare del resto chiaro che le innumerevoli pseudosoluzioni e le critiche senza fondamento più che risolvere hanno contribuito ad animare la confusione dei mercati in un momento in cui l'Italia, più che mai, necessita di una coesa e coerente politica economica.

appare chiaro che le decisioni prese sono state graduali, sofferte e ponderate, non per incertezza o ripensamento da parte del Governo, ma in considerazione della preoccupazione nell'applicare misure rigorose a carico dei cittadini e del sistema economico. La decisione di porre la fiducia e di modificare il provvedimento è la conseguenza della mutata situazione dei mercati finanziari europei e delle indicazioni arrivate sia dal presidente Napolitano che dall'Unione europea, la quale ha accolto positivamente il nuovo testo e auspica che la manovra sia approvata il più presto possibile. possibile. A tal proposito, si evidenzia che già nella giornata di oggi per Piazza Affari vi è stato un avvio brillante e quindi un segnale positivo di apprezzamento per il nuovo testo della manovra. In conclusione, il provvedimento in esame, a seguito delle nuove proposte del Governo e del dibattito

Presidente, quello che stiamo facendo e dicendo in queste ore era scritto in quello che abbiamo fatto e detto nei giorni e nelle settimane passate.

il 22 agosto, che sintetizzava il percorso seguito dall'economia greca nell'ultimo anno e mezzo. È facile arguire che di quel percorso ne abbiamo già fatto una buona parte. Per la verità, in alcuni casi l'abbiamo fatto anche a tappe forzate. Mancavano solo due ingredienti a quella ricetta: l'aumento dell'IVA e il *downgrating* del debito. Al primo ci stiamo pensando in queste ore. Del secondo i mercati finanziari si sono cominciati a preoccupare e ad occupare fin da ieri. La richiesta che ci era arrivata dai mercati finanziari e dall'Europa nelle ultime 48-72 ore era solo una ed era di ripristinare un po' della nostra credibilità.

ad una maggiore e non ad una minore rigidità nei confronti dei Paesi membri che devono tenere in ordine le loro finanze pubbliche. Questa è la strada che ormai stiamo seguendo. È una strada in cui la Germania si assume progressivamente quote crescenti di responsabilità, ma le condiziona in maniera molto pressante e crescente ad una disciplina sempre maggiore da parte degli Stati membri. E la credibilità è fatta non solo e non tanto di maggiori entrate e di minori spese. In realtà, è fatta soprattutto di un riconoscimento senza riserve dell'esistente

del contribuito di solidarietà, ciò di cui discutiamo oggi è sostanzialmente una sola cosa: è l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21 per cento. A questo incremento - ed è questo il punto - si chiede di fare molte cose e ho l'impressione che siano anche troppe. Si chiede di offrire una copertura più certa di quella offerta dalla lotta all'evasione in presenza di una cancellazione del precedente contributo di solidarietà, di anticipare ad oggi la parte della manovra, ancora piuttosto vaga ed incerta, connessa alla delega fiscale ed assistenziale e di precostituire la possibilità di rispondere alle conseguenze della minore crescita che io credo più o meno il 20 settembre in quest'Aula finiremo per certificare nella Nota di aggiornamento. Va da sé che è un po' troppa roba da chiedere ad una sola cosa. L'incremento dell'IVA era già previsto a garanzia dei risultati derivanti dalla delega. Sebbene oggi utilizzato per sostituire coperture incerte, non potrà più essere utilizzato domani. E questo si vede abbastanza facilmente. E se venisse utilizzato domani per evitare di prendere atto della conseguenze sul bilancio pubblico di una minore crescita, allora non lo si può presentare oggi come un rafforzamento della manovra.

Una risposta credibile si sarebbe dipanata in maniera completamente diversa. Avrebbe cominciato innanzitutto con il non cifrare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e avrebbe chiuso, anche se malamente a mio modo di vedere, le le coperture della manovra di agosto con altre maggiori entrate, quelle appunto derivanti dall'aumento dell'IVA. Simultaneamente avrebbe preso atto che alla manovra di agosto dovrà - temo - far seguito inevitabilmente una manovra di settembre

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, i dati allarmanti dei mercati e delle borse, che si sono ulteriormente aggravati in questi ultimi giorni e a cui ha fatto seguito anche l'appello del Presidente della Repubblica a rafforzare immediatamente la manovra

Voglio ringraziare a questo punto tutti i colleghi componenti la Commissione bilancio per l'intenso lavoro svolto in queste difficili settimane, e confermo che siamo convinti della necessità dei sacrifici, ma mi preoccupano sinceramente diverse misure previste nel presente decreto, in particolare la disposizione che porta l'aliquota IVA al 21 per cento, in quanto colpisce direttamente il consumo di tutti i cittadini e sicuramente avrà ripercussioni negative sul consumo in generale. Mi soffermo brevemente sulla questione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne: adeguamento inevitabile e richiesto più volte dall'Europa, ma invito in proposito, ancora una volta e con insistenza, come ho già fatto diverse volte, il Governo ad affrontare in modo più approfondito la politica della famiglia, a tenere conto della grave carenza dei servizi sociali e del ruolo della donna lavoratrice nella famiglia e del ruolo della donna come madre, riconoscendo ai fini pensionistici dei periodi figurativi almeno di un anno per ogni figlio educato e cresciuto. Devo aprire anche una piccola parentesi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che preoccupa molto gli operatori ed in particolar modo i piccoli imprenditori, che trovano insuperabili difficoltà di adeguamento tecnico ed organizzativo al nuovo sistema. Mi auguro che il termine di entrata in operatività, previsto per il 9 febbraio del 2012, consenta veramente ai competenti Ministeri di approvare tutte le dovute modificazioni volte alla semplificazione delle disposizioni attuali. delle disposizioni attuali. Per quanto riguarda le autonomie speciali, voglio ringraziare il Governo e i colleghi del Senato per avere accolto la nostra richiesta, avanzata insieme a tanti nostri colleghi, riguardo all'inserimento nel testo del decreto della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Grazie a questo inserimento abbiamo avuto la conferma di una grande serietà da parte del Governo e la dimostrazione di voler proseguire nel cammino intrapreso verso nel cammino intrapreso verso il federalismo fiscale e lo sviluppo delle autonomie speciali nel pieno rispetto degli statuti dell'autonomia, delle norme di attuazione e in particolar modo dell'articolo 27 della legge sul federalismo e, di conseguenza, del patto Signor Presidente, avendo a disposizione solo questi pochi minuti, concludo ribadendo che nel complesso ritengo che il decreto, così come da ultimo modificato, abbia le potenzialità per ridurre il

all'approvazione delle riforme previste. Sarà compito del Governo applicare le misure previste in questo provvedimento in modo corretto ed uniforme su tutto il territorio dello Stato e nei tempi stabiliti dalla manovra stessa per essere credibile.

potremmo essere in qualche modo anche soddisfatti, se non altro del lavoro che è stato svolto in Commissione, in particolare per l'approvazione dell'emendamento riferito al comma 2 dell'articolo 1, che riguarda i fondi FAS, siamo riusciti in qualche modo a salvare i fondi per la programmazione regionale, anche se credo che finalmente dovremmo fare una riflessione molto più seria su questo punto. Nel maxiemendamento troviamo infatti nel piano per il Sud che, con che, con un meccanismo abbastanza contorto, di fatto si salvano soltanto i fondi FAS per la programmazione nazionale che potrebbero sforare il Patto di stabilità interno.

Se il meccanismo continuerà a rimanere questo, quei fondi rimarranno inutilizzati, li restituiremo all'Unione europea, le aree sottoutilizzate rimarranno tali e tutto ciò mentre Potremmo essere abbastanza soddisfatti per il fatto che si sia data attenzione anche ai Comuni, se non altro perché i Comuni possano trattenere il 100 per cento dei proventi della lotta all'evasione. Anche qui però, Sottosegretario, non credo che la lotta all'evasione debbano farla semplicemente i Comuni. Proprio oggi ho presentato un'interrogazione molto articolata sull'evasione o elusione - non so come vogliamo definirla - delle grosse aziende petrolifere, che versano molto poco allo Stato in termini di accise, con dei meccanismi veramente infernali che, a conti fatti, producono un'elusione - la definisco

D'altra parte, non siamo soddisfatti neanche del fatto che sia stata eliminata la possibilità per le aziende di vedersi riconosciuti i crediti vantano nei riguardi della pubblica amministrazione perché, purtroppo, questo è un problema che ci stiamo trascinando da tempo. Un altro fatto positivo che abbiamo annoverato è il riconoscimento del Fondo per per la progettazione, che indubbiamente è un notevole passo avanti, soprattutto per quegli enti locali cosiddetti di periferia, che non si possono consentire un lusso del genere.

Questi grossi operatori usufruiscono di servizi con costi pagati da noi, dalla collettività e, poi, pagano le loro tasse - quando e se le pagano - all'estero, non contribuendo minimamente in termini di solidarietà

i fitti per gli uffici giudiziari, finanziari e, in genere, per gli uffici che vengono garantiti attraverso i Comuni con rimborsi dati *a posteriori*, quando vengono dati, con un riconoscimento

lo Stato, da un lato, o l'ente locale, dall'altro, o *pro-quota* l'uno e l'altro, quanto meno possono patrimonializzare ed avere una maggiore capacità d'indebitamento, o quanto meno

per legge e non per invenzione, all'emittenza locale. Mantenere l'emittenza locale non è un fatto assistenziale, ma un fatto di grande democrazia, specialmente in un sistema dell'emittenza radiotelevisiva

pagando a rate il loro debito nei riguardi della previdenza sociale. Non si riesce a venire a capo di una situazione del genere. Eppure, se facessimo il conto di quante multe paghiamo all'Europa, altro che debito pubblico! Basterebbe rimanere nella legalità

che non prevede solo l'abolizione delle Province, cosa che potrebbe sembrare quasi un fatto politico punitivo nei riguardi di chi non vuole l'abolizione delle Province. Noi consideriamo tutto l'insieme: le unioni dei Comuni, gli ambiti territoriali

Mi avvio a concludere, signor Presidente.

che questi ed altri argomenti che abbiamo posto all'attenzione del Governo vengano esaminati con grande volontà di procedere, soprattutto nei riguardi di quelle zone d'Italia come il Mezzogiorno nelle quali si può maggiormente investire per determinare sviluppo

giacché il completamento della manovra, nel bene o nel male, a seconda dei giudizi, è avvenuto solo questa mattina. Oggi, pertanto, ha senso svolgere una valutazione complessiva rispetto a quello che ci troviamo di fronte.

i suoi contenuti ed i suoi possibili effetti occorre avere chiaro a cosa deve rispondere. Sappiamo tutti che essa deve rispondere ai mercati finanziari che hanno messo l'Italia sulla graticola della cosiddetta speculazione, sulle montagne russe, soprattutto per ciò che riguarda lo *spread* nei confronti dei titoli tedeschi,

In entrambi i casi, i mercati e le autorità europee si aspettano che l'Italia realizzi riforme strutturali che consentano un aggiustamento e quindi un azzeramento del *deficit* pubblico (nella manovra di luglio era stato indicato come termine il 2014 ed in quella ora

con tagli di spesa pubblica corrente, almeno per due terzi, con possibili aggiustamenti dal lato delle entrate per non più di un terzo, ma con un'operazione che liberi più risorse di quelle necessarie al puro azzeramento contabile del *deficit* pubblico nel 2013, per poter spostare le risorse a sostegno della crescita economica.

Il picco dei 400 punti base di differenziale tra titoli italiani e titoli tedeschi è stato raggiunto dopo la manovra di luglio, e non prima. Quindi, evidentemente, gli operatori, in tutto il mondo, hanno dato un giudizio molto netto

la risposta adeguata, sia ai mercati, sia alle autorità europee: ai mercati, per evitare che ricomincino, nel giro di pochi giorni, o anche di qualche settimana, a mettere i titoli italiani sulle montagne russe; alle autorità europee, e in particolare alla Banca centrale europea, per convincerle che gli eventuali interventi di acquisto di titoli italiani sul mercato da parte della BCE andranno a buon fine, cioè

Questa è la questione, che non è una questione semplicemente del Governo; non è una questione semplicemente della maggioranza; non è una questione delle opposizioni, ma è una questione di 57 milioni di cittadini, di 21 milioni di famiglie e di 5 milioni di imprese. imprese. La cosiddetta classe politica ha la responsabilità di assumere in sé le decisioni per rispondere in modo adeguato

anche se avvenisse in tempi rapidissimi, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Devo dire che avevo tentato personalmente, in Commissione bilancio, nella seduta di giovedì della settimana scorsa, di invitare tutti i colleghi, Governo, maggioranza e opposizione, a ragionare su questi argomenti, magari per un quarto d'ora o per mezz'ora, e a non passarci sopra come fosse acqua fresca, solo perché alcune proposte, chiaramente alternative a quelle del Governo, venivano da una parte piuttosto che da un'altra. Avevo avvertito in Commissione bilancio che purtroppo, alla riapertura dei mercati di lunedì, sarebbe potuto succedere ciò che è avvenuto, tanto che il Governo si è convinto questa notte ad aggiustare ulteriormente la manovra. oppure, se tali turbolenze dovessero emergere tra un paio di settimane, faremo un altro aggiustamento in sede di legge di stabilità. Questo è lo scenario, e mi permetto di richiamare veramente ad un minimo senso di responsabilità collettiva. Vengo allora all'analisi della manovra per capire se è la risposta giusta ai mercati e alle autorità europee. Certamente, di fronte a queste situazioni di emergenza, occorre far presto e dare una risposta rapida, ma l'esperienza di luglio ci dice come palesemente dimostrato, se la risposta è rapida, si fa presto, ma si fa male e anche peggio. Quindi, la richiesta è duplice: bisogna fare presto, ma bene, perché se si fa presto e male la situazione peggiora.

che nascondono aumenti di spesa effettivi, ma generici e nascondono il cuore della politica, che è quello di scegliere. Il taglio di spesa orizzontale o il taglio di trasferimenti generico agli enti locali è la rinuncia a fare politica e, se mi permettete, non è neanche quella nobile professione del ragioniere, perché almeno questi sa fare di conto e qualche volta deve rifiutarsi di firmare conti palesemente falsi. palesemente falsi. Mercato e autorità europee - signor Presidente, lo dico anche per esperienza diretta e conoscenza di molti di questi soggetti operatori, persone fisiche

la manovra di aggiustamento modifica questi numeri e, quindi, nel 2013 quanto sarà la spesa pubblica, quanto saranno le entrate e quanto sarà il *deficit*. Non guardano i tagli sui tendenziali, gli aumenti di imposte che ci sono la sera e non ci sono più la mattina, ma questi numeri. Facendo come loro l'analisi della manovra, emerge emerge che la manovra che il Senato dovrebbe approvare stasera con la fiducia da qui al 2013, dopo la sua approvazione, determina un aumento di entrate totali di 100 miliardi di euro

sono i numeri della Tabella del Documento di economia e finanza del Ministero dell'economia e delle finanze che loro guardano. Questi 100 miliardi serviranno

con un taglio nominale di investimenti pubblici di 11 miliardi, per un netto di spesa complessiva di +25 miliardi.

Allora, da domani mattina, tutti gli analisti si chiederanno: con una manovra di più tasse, più spesa corrente e meno investimenti, anche se, *ex ante*, a bocce ferme, si raggiunge contabilmente il *deficit* zero nel 2013, quali effetti si produrranno sull'economia italiana da qui a

che l'obiettivo di *deficit* zero nel 2013 questa manovra non lo raggiungerà, nonostante peraltro la pressione fiscale salga dal 42 al 45,2 per cento, se si considera

è evidente che la pressione fiscale salirà di tre punti in tre anni. Nonostante questo, dicevo, l'obiettivo di zero *deficit* non viene raggiunto. La settimana scorsa il Fondo monetario internazionale ha reso note le nuove previsioni sull'economia italiana e la sua crescita, che non incorporavano però ancora gli effetti di questa manovra, visto che non era stata ancora approvata. Le differenze sono le seguenti. Tutti i conti che ha presentato il Governo sulla finanza pubblica dipendono dall'ipotesi, confermata dal Governo stesso, di crescita dell'1,7

che fa il Governo, avevo fatto una stima molto, molto prudente. Ora qui siamo tra intimi, quindi possiamo anche dirci certe cose, ma non possiamo illuderci che operatori ed autorità europee

titoli di Stato italiani e ad evitare che lo *spread* balzi di nuovo sopra i 400 punti? Ma soprattutto, sino a quando quando durerà questa finestra di opportunità che c'è stata concessa dagli acquisti della Banca centrale europea? E ancora: questa manovra che state per varare

con una proposta alternativa, nel senso di quello che chiedono i mercati e l'autorità europea, cioè tagli di spesa e sostegno alla crescita e allo sviluppo.

dei provvedimenti mi rimetto agli interventi dei colleghi del mio Gruppo che sono già intervenuti in modo preciso. Chiedo formalmente in quest'Aula, come ho fatto più volte, come sia possibile e presumo la risposta del Governo, che non ha dato un emendamento approvato in Commissione, quello relativo ai pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazione alle medie e piccole imprese, che non ha niente a che vedere con il debito pubblico, che riguarda un'operazione privata tra un'impresa e una banca che, bontà sua, a libera scelta della banca potrebbe anticipare il pagamento di quelle fatture, *pro solvendo*; mi aiutino i giuristi, non sono un esperto; ma ciò vuol dire che non cambia nulla rispetto a chi è il debitore e chi è il creditore: è la banca che fa un'operazione di anticipo su una fattura, come fa normalmente tra imprese private.

che balzi in alto il debito pubblico attraverso le regole della contabilità SEC e che vada messo tutto in indebitamento netto. Francamente su questo tema prego il Governo e la Ragioneria di smetterla di prendermi personalmente in giro, perché la ritengo un'offesa personale.

che eventualmente avete impedito al Governo di inserire quell'emendamento nel maxiemendamento per quelle motivazioni tecniche vi vergognate o no di bollinare come entrate certe anche nella relazione tecnica che sta nell'ultimo emendamento del Governo un miliardo e mezzo di entrate da una lotta all'evasione, che è il motivo per il quale i mercati lunedì scorso hanno fatto saltare gli *spread*?Infatti, appena hanno letto che c'erano quelle entrate da lotta all'evasione lo *spread* è andato a 380. E allora in questa relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria come si fa a firmare che ci sono un miliardo e mezzo di entrate certe dovute alla lotta all'evasione?

più gettito per 169,7 milioni di euro nel 2012, 226,3 milioni di euro nel 2013 e così via nel 2014.

perché queste cose non solo non le crediamo noi (e nemmeno un piccolo ragioniere di campagna come il sottoscritto), ma sui mercati internazionali sono cose devastanti! La prova l'abbiamo avuta lunedì

necessaria per garantire il pareggio prima previsto per il 2014 e poi - come è noto - anticipato al 2013. Dopo aver concordato in sede europea, sin dal marzo scorso, la necessità di raggiungere tale obiettivo, unito a quello della progressiva riduzione dell'incidenza del debito sul PIL, e dopo aver acquisito l'atto di indirizzo parlamentare, il DEF, ai primi di maggio, che prevedeva la necessità di un intervento correttivo di 40 miliardi, il Governo italiano ha provveduto - nel modo che sappiamo - con una approssimazione, confusione e inadeguatezza senza precedenti. Durante tutti i numerosi passaggi dal mese di giugno ad oggi, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia hanno sempre inutilmente affermato che le misure erano efficaci, che i saldi erano assicurati, che il pareggio sarebbe stato conseguito. Il diluvio di incidenti, dichiarazioni, errori, conflitti interni al Governo e alla maggioranza, marce indietro e cambiamenti repentini sono impressionanti. Cito a titolo di esempio le dichiarazioni di queste settimane, a partire dall'iniziale incidente, che molti hanno già dimenticato, contenuto nel primo decreto di giugno sulla norma "salva Mondadori", poi stralciata,

«Ne siamo totalmente convinti», disse il Ministro dell'economia il 30 di giugno, quando la manovra era di 25 miliardi. Il 4 agosto, intervenendo in Parlamento, il Presidente del Consiglio ribadì la certezza - cito testualmente - "di centrare l'obiettivo del pareggio di bilancio con le misure già adottate" e parlò di mercati - lo ricorderete - quali orologi rotti. Disse sostanzialmente di non sentire i mercati in quanto orologi rotti. Il 26 agosto, dopo quelle giornate turbolenti, il ministro Tremonti dichiarò che occorrevano invece scelte di maggiore rigore. Il 30 agosto, dopo la riunione di Arcore, di cui non è rimasto praticamente nulla, il Presidente del Consiglio assicurò, con i toni esaltanti che ricordiamo, che i saldi erano invariati, che tutto era a posto. Fino ad oggi, con le scelte che conosciamo, tutte consistenti in un aumento d'imposta, quelle dichiarazioni sono totalmente smentite. Non si contano inoltre, sempre in questo arco temporale, signora Presidente, i richiami del Presidente della Repubblica, della BCE, della Banca d'Italia

il vice direttore della Banca d'Italia, durante la sua audizione in Commissione bilancio, ha dichiarato espressamente che non vi erano ostacoli a rendere nota quella lettera, ma che ciò doveva essere fatto da parte del destinatario della lettera, ovvero il Governo delle autorità europee, di alcuni Capi di Stato di Paesi europei, di moltissimi autorevoli commentatori, tutti concordi nel ritenere deboli, non strutturali molti degli interventi, non certi - per cui incerti - i saldi e quindi l'obiettivo del raggiungimento del bilancio; tutti concordi, proprio tutti, comprese le istituzioni e le parti sociali audite in Commissione bilancio; tutti, tranne il Governo e la maggioranza che lo sostiene, isolati come mai prima era accaduto. Dunque, all'origine delle gravi e ripetute turbolenze sui mercati finanziari, degli attacchi ai nostri titoli di debito, con una insostenibile lievitazione del differenziale del tasso di interesse rispetto al titolo di riferimento, il *Bund* tedesco, ci sono certamente fattori di crisi internazionale, i mostri della speculazione che vede il nostro Ministro dell'economia. Ci sono però anche, in misura rilevante, l'incertezza, la scarsa credibilità e la confusione generata dalle decisioni del Governo. è ormai una verità storica riscontrabile, che determina il permanere dei fattori di rischio per il nostro debito pubblico e per l'affidabilità del Paese. Basti guardare

durante l'esame a luglio in Senato, con l'integrazione della cifra della delega fiscale; la cifra si accresce poi di 7,4 miliardi (sempre a regime) con il decreto che stiamo discutendo nella sua versione originaria aumenta - ancora - di 4,3 miliardi con il maxiemendamento di oggi, arrivando quindi al totale necessario per ottenere - forse - il pareggio di bilancio nel 2013 e nel 2014, per un ammontare complessivo di 59,6 miliardi. parlo dell'effetto della manovra a regime nel 2013 e nel 2014, perché la sommatoria degli interventi dei singoli anni dà ovviamente una cifra molto superiore. Perché si è verificata questa lievitazione di quasi 20 miliardi, ossia dai 40 originari a 60 a regime? A quali ragioni è da ricondurre uno scostamento di tali proporzioni? Si tratta di un quesito serio, signor Presidente, perché il Parlamento agisce per espressa previsione della legge di contabilità, sulla base del quadro programmatico e macroeconomico fissato annualmente nel DEF e nelle note di aggiornamento. Quello è il quadro di riferimento: il Parlamento e, tanto più, il Governo non possono dare i numeri. Come è noto, fissava in 40 miliardi la manovra per ottenere il pareggio di bilancio; noi oggi, sotto la spinta dei mercati e delle più alte istituzioni italiane ed europee, ne approviamo una di più ampie dimensioni.

alla prima, manca un documento presupposto: noi, cioè, non siamo nelle condizioni di valutare l'adeguatezza di questi numeri, ovvero il DEF, l'aggiornamento del DEF o un documento simile, come avevamo tempestivamente richiesto all'inizio dei lavori della Commissione, non ottenendo alcunché dal Governo. Ciò rende queste previsioni incerte. luogo, la manovra non incorpora gli effetti recessivi ad essa correlati (aggravati dagli effetti depressivi sui consumi derivanti dall'aumento dell'IVA oggi disposta), così come le variazioni in diminuzione dell'andamento del prodotto, di recente stimate dal Fondo monetario in misure di molto inferiori a quelle programmatiche, nei termini e con i contenuti cui si è diffusamente riferito il presidente Baldassarri poco fa. Permane nella pancia della manovra l'enorme punto interrogativo sugli effetti stimati della delega fiscale e assistenziale. Come sappiamo, si prevede di ricavare 20 miliardi ma senza dire come,

della vostra politica economica. Dunque, anche il rafforzamento finanziario di oggi non ci mette al riparo dai rischi per il prossimo futuro. Speriamo fortemente di sbagliarci, ma abbiamo il dovere di segnalare questa seria preoccupazione. La manovra era e rimane iniqua, colpisce lavoratori e famiglie ed è poco credibile, oltre che recessiva. Essa è recessiva più di quanto sia fisiologico attendersi da una qualunque manovra restrittiva. Si introducono - inoltre - tagli pesantissimi senza averne valutato l'impatto e gli effetti *ex ante*: mi riferisco al taglio di 8,5 miliardi a carico dei Ministeri, che i Ministri di questo Governo ritengono non sostenibile, a partire dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa. inoltre, un taglio micidiale per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, che sono sul piede di guerra. Per fortuna, è stato approvato il nostro emendamento sulla *spending review*: una norma serissima, che ha un carattere programmatico ma per la cui attuazione occorrerebbe una forte determinazione del Governo a lavorare da subito per poter percorrere quella strada. Pochissime nostre proposte hanno trovato accoglimento, anche se esse rappresentano una sia pur lieve mitigazione del carattere sconclusionato delle misure. Molte altre potevano trovare una più favorevole apertura da parte del Governo, ma ciò non è accaduto.

Nel mese di settembre il nostro Paese dovrà collocare sui mercati finanziari internazionali titoli di Stato, per la sostenibilità del nostro debito, per un importo di circa 45 miliardi. Entro la fine dell'anno, poi, sempre il nostro Paese dovrà collocare titoli del debito sovrano per un importo complessivo di circa 148 miliardi. Dalle dimensioni ci si rende facilmente conto che ogni passo, ogni ritardo ed ogni indecisione da parte di questo Governo e di questa maggioranza determineranno effetti devastanti,

trovo sia estremamente critica l'assenza del Ministro dell'economia in un momento in cui il Parlamento sta decidendo del futuro del Paese. Questa assenza può avere un duplice significato:

oppure l'assenza del Ministro dell'economia non fa altro che confermare la scelleratezza politica di questo Governo e di questa maggioranza, oltre che l'accanimento nella dissipazione dei conti pubblici. Questa è la fotografia che viene in questo momento dai banchi vuoti del Governo e dall'Aula semivuota. È un dato politico. Lo stesso Presidente della Repubblica è stato costretto nell'ultimo mese ad intervenire più volte con appelli importanti, nell'ultimo dei quali ha chiesto che venissero adottate all'interno di questa manovra misure efficaci ed immediate. A questo appello possono rispondere solo il Governo e la maggioranza, perché rientra nel loro ruolo e nella loro responsabilità, o meglio nella loro irresponsabilità.

rappresenta un quinto della quarta manovra, quella che era uscita dall'incontro ad Arcore. Rappresenta un quarto della manovra del 13 agosto, la quale a sua volta era una manovra correttiva nei confronti di quella del mese di luglio, bocciata nei tempi - anche qui dobbiamo dire la verità

perché non era credibile per l'assenza totale di interventi sulla crescita del Paese, ma bocciata anche nella credibilità di un Governo che doveva affrontare questa situazione critica. E la manovra di luglio, a sua volta,

ma qualcuno sa che fine ha fatto il credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione che doveva essere assegnato alle imprese in attività con le università o gli enti pubblici, che doveva essere assegnato per le nuove assunzioni dal Meridione? Sono rimaste tutte lettera morta. Allora, questa manovra di agosto - arriviamo a questa manovra che oggi è in Aula - cosa fa? Agisce sulle maggiori entrate. Il collega Legnini parlava di un aumento negli ultimi 12 mesi della pressione fiscale, da parte di un Governo che aveva detto che non metteva le mani

perché la manovra - si dimentica - stabilisce anche una anticipazione della possibilità di attuazione del federalismo fiscale - federalismo avvelenato che stanno producendo questo Governo e questa maggioranza - per cui le Regioni con le aliquote IRPEF e i Comuni con l'anticipazione degli effetti della tassazione con l'IMU saranno saranno costretti ad un aumento della pressione fiscale che alcuni economisti hanno già quantificato intorno al 52-53 questa manovra determina anche una sovrastima degli effetti per far quadrare i conti. E come lo fa?

un imbroglio legalizzato che va a colpire le fasce più povere e più deboli del nostro Paese e che va a colpire la dignità di un Parlamento che solo pochi mesi fa ha approvato all'unanimità una risoluzione

un presunto, fumoso contrasto all'evasione fiscale. Ma il primo a non credere a questo provvedimento è proprio il Governo. E lo dimostra in due esempi molto semplici: il primo, il recupero delle risorse delle entrate non pervenute del condono del 2002. Era stato quantificato dalla Corte dei conti in quattro miliardi di euro che erano stati persi dalle casse dello Stato, perché evasori ed elusori avevano pagato la prima rata e poi erano scomparsi nel nulla. l'Agenzia delle entrate ha detto che di questi quattro miliardi, due miliardi e mezzo sono già dimenticati, irricevibili, irrintracciabili. sulle altre risorse il Governo giustamente non ha neppure cifrato, quantificato l'entrata nelle casse dello Stato, perché è il primo a non credere nel recupero di questo condono. questo condono. In Commissione bilancio abbiamo assistito ad un ministro Tremonti che ci ha elogiato gli effetti benefici dell'obbligo

nella relazione tecnica come entrata) 145 milioni di euro, e poi all'improvviso questa norma scompare. Scompare anche la norma sulla soppressione degli enti inutili, che è stata tanto decantata e tanto annunciata dal ministro Calderoli; scompaiono le liberalizzazioni, che sono diventate solo dei principi astratti. astratti. L'unica liberalizzazione che troviamo in questa manovra è la liberalizzazione al licenziamento, perché si è fatto credere che l'incentivazione al sistema industriale non avviene attraverso un impulso alla ricerca, all'innovazione di prodotto, di sistema, di processo, ma avviene attraverso lo smantellamento dello statuto dei lavoratori e del contratto collettivo nazionale. E allora, signora Presidente, l'Europa ci chiedeva effetti immediati, perché gli annunci non fanno altro che danneggiare ulteriormente la credibilità del Paese; ci chiedeva che i risultati fossero quantificabili (e sappiamo che, se la crescita del Paese è stimata in ribasso rispetto a quanto quantificato dal Governo, non otterremo neppure questo effetto); questo bisogna essere particolarmente attenti, che ci sia la credibilità nella gestione di questa manovra, e questo Governo e questa maggioranza in queste settimane hanno dimostrato l'incapacità di orientamento da parte del Capo del Governo. Ciò è giustificato per i guai ed i problemi che ha, ha dimostrato di avere incapacità di coordinamento di questa maggioranza, che sta pensando più alle lotte interne di potere che non agli interessi generali del Paese. signora Presidente, mi consenta: questa maggioranza e questo Governo, in termini di aggiustamento dei conti pubblici, passerà alla storia perché l'unico aggiustamento che sarà stato capace di fare in questi tre anni è quello dell'aumento del costo della spigola.

un articolo fortemente voluto da tutti gli autonomisti che lo hanno votato all'unanimità in Commissione bilancio anche in modo trasversale, viene giudicato da noi in modo positivo. Da più parti infatti oggi si alza, e anche da parti per noi inaspettatamente contrarie, una richiesta di tagliare fondi alle Regioni a statuto speciale, istituzioni che per questi osservatori, mi si permetta, spesso superficiali, vogliono solo difendere privilegi ottenuti a danno delle Regioni ordinarie. La specificità delle nostre Regioni riconosciuta dalla Costituzione ha invece una ragione reale e tuttora esistente in particolari situazione storiche, geografiche, culturali e linguistiche. Gestire infatti i servizi in Regioni montane o insulari è obiettivamente diverso e più costoso: si pensi alle piccole scuole di montagna, alla sanità, ai trasporti, alla stessa energia e a come portarla, a mandare i giovani in università fuori dalla nostra valle. In modo contraddittorio e quindi non chiaro, però, insieme a questo giusto articolo 19-*bis* rimane il comma 8 dell'articolo 1, che prevede, per il raggiungimento del patto di stabilità, una somma per le autonomie speciali addirittura superiore a quella prevista per le Regioni ordinarie: 8 milioni di abitanti di queste cinque Regioni a statuto speciale pagano il 65 per cento di quanto previsto per tutte le Regioni. Questo mi sembra più che ingiusto e non equo. Come si accorderà questo articolo 1 con l'articolo precedentemente citato, che richiama appunto l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009? Che questi importi vengano invece concordati tra Regioni e Governo, tanto più se vengono già fissati gli importi e ci viene detto continuamente che bisogna arrivare al pareggio di bilancio. Noi siamo d'accordo, signora Presidente, su una riorganizzazione e sulla necessità di ottimizzare e risparmiare, ma vogliamo che il prelievo sia equo per i tutti i cittadini italiani, che hanno tutti gli stessi diritti. Nel bisogno di fare cassa, non vorremmo che anche qui si colpissero i più deboli, i cittadini delle Regioni autonome, numericamente meno influenti e condizionanti sulle grandi scelte che oggi bisogna prendere, ma portatori di necessità particolari e, quindi, di diritti che ora non si vorrebbe più riconoscere e rispettare. Il nostro voto, proprio per questa ambiguità del testo, ma pur con il senso responsabilità che ci ha sempre caratterizzato, non può essere che quello di astensione.

Governo, colleghi, sono già intervenuto ieri nella fase di discussione di quello che era il testo del decreto prima del deposito da parte del Governo del maxiemendamento. In tale intervento intervento ho evidenziato tutte le caratteristiche positive del decreto ed anche i messaggi importanti di stabilità che dobbiamo dare al Paese, al sistema europeo

Grazie

è arrivati all'aumento dell'IVA, la decisione più scontata, meno coraggiosa, meno efficace nel rapporto con le opinioni pubbliche che in Europa e fuori dall'Europa interverranno su questi temi,

Può essere questo un punto sul quale attaccare. E nel Governo, e nel nostro dibattito, questo problema non c'è. Il PD, rispetto

infatti pensare ai servizi esterni alle imprese, alle infrastrutture che non ci sono e al fatto che siamo dietro ai più forti Paesi europei. Quelli sono problemi e inadempienze che incidono sul rapporto con l'investimento estero. C'è anche la politica industriale

Salario e produttività del lavoro legati, in un sistema industriale e produttivo come quello italiano, così differenziato, non potete gestirli con il contratto nazionale, che non va però cancellato.

Ciampi nel 1993, che compì un passo avanti rispetto ai ritardi su questo problema, e andò avanti per diversi anni. Poi intervenne un tran tran che rallentò la possibilità di lavorare con i contratti aziendali. un contratto del 2008, parziale, e nel 2009, alla fine, si arrivò alla rottura tra le organizzazioni sindacali, proprio su questo tema. due anni difficili, di contraddizioni, due anni di conflitti tra i sindacati che hanno ridotto la possibilità di applicare questa contrattazione decentrata in maniera più massiccia (vi è stata la vicenda FIAT, che tutti conosciamo). Poi, il 28 giugno scorso, è stato compiuto di nuovo uno sforzo straordinario, innanzitutto delle parte sociali, comprese le controparti padronali, che sono riuscite a realizzare una svolta, straordinaria e inaspettata, su questo problema, tutti insieme. Quell'accordo, sui contenuti e su quali materie affrontare (dallo sviluppo alla gestione delle crisi, ai rapporti di lavoro, alla produttività), quello spazio che ci si aspettava proprio da Giugni (che sorriderà da dove si trova), perché, finalmente, tale accordo ha creato le condizioni per andare avanti. E questo è uno dei punti

Il Ministro del lavoro, il 29 giugno, rispetto a questo accordo, fortemente innovativo, afferma che «l'intesa raggiunta ieri tra sindacati e Confindustria sulle contrattazioni porterà, in primo luogo, un vantaggio per la credibilità del Paese nel suo insieme e un segnale di coesione sociale, e gli stessi analisti dei mercati finanziari lo apprezzeranno». Il 29 giugno, Si può dire che dentro una fase conflittuale, complicata, dura e difficile, che ha messo in difficoltà le organizzazioni, c'è stata una svolta anche da parte della CGIL e lo dico io che per lo sciopero

a gamba tesa con il decreto che riapre la discussione di principio, che ha sempre un valore, e che con l'introduzione della territorializzazione della modalità della contrattazione apre un problema che non può essere più gestito a livello generale. C'è bisogno per queste materie di una linea comune e di un punto di riferimento generale. Il

il dialogo ed è intervenuto, dopo un accordo faticoso che li ha visti tutti coinvolti, in una materia dove tradizionalmente le parti sociali sono sempre state autonome la legge è intervenuta molte volte come legge di sostegno. Se c'è l'obiettivo di amplificare l'elasticità e i poteri anche diversificati dentro l'azienda, si cerca di sviluppare l'accordo del 28 giugno 2011 e di far camminare in avanti questa posizione perché è rilevante e giusta ai fini della ripresa, degli investimenti esteri in Italia e di una flessibilità maggiore. Noi ci siamo trovati dinanzi a un fatto

Per poter sviluppare i contratti aziendali di produttività in maniera significativa c'è bisogno di un rapporto disteso tra gli attori,

guardano certamente a quello che abbiamo fatto, ai numeri, alla capacità di risposta finanziaria alle difficoltà che abbiamo, ma vi è innanzitutto il problema del nostro debito e nei rapporti dentro l'Europa della credibilità politica e sociale del nostro Paese.

una difficoltà maggiore all'interno anche dei rapporti sociali nel nostro Paese possa esserci. A chi serve? All'Italia? Certamente no. Alla politica? No,

finestra"). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

in Commissione bilancio del Senato sono state rilevate alcune questioni sulle quali il Governo

Con riferimento all'articolo 1-*ter* (pagina 7 del testo) il Governo ritiene di specificare la decorrenza di efficacia della disposizione. Quindi va aggiunto il seguente comma 2: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

all'articolo 2, comma 2-*quater* (pagina 8 del testo), il riferimento al comma 2 è errato e va inteso come riferito al comma 2-*ter*.

il Governo ritiene opportuno sostituire le parole:

17, commi 1 e 2 (pagina 25 del testo), il Governo ritiene necessario sostituire la fonte normativa presente Copertura finanziaria. Il Governo riformula l'articolo 19 sulla copertura finanziaria.

maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280 milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto 1.330 milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

che l'enumerazione vada un po' oltre quanto avevamo annotato in Commissione. Ma comunque ci riserviamo di verificarlo. Le chiedo soltanto la possibilità di farlo da qui al voto

riguarda la responsabilità penale tributaria. Il Sottosegretario ha parlato di refuso, ma io vorrei chiarire che si tratta di un intervento che va ben oltre il refuso. Infatti,

che rende la fattispecie penalmente rilevante sotto il profilo del non obbligo di concessione della sospensione condizionale della pena una fattispecie amplissima. In pratica si può evadere fino a cifre esorbitanti con l'introduzione della soglia del 30 per cento senza per questo veder revocato

i Repubblicani hanno giudicato e giudicano la manovra tardiva e insufficiente per far superare al Paese la grave crisi che attraversa, anche per l'assenza nella stessa di riforme strutturali e di misure capaci di consentire la crescita, e temono che fra qualche tempo sarà necessario adottare altri e più incisivi provvedimenti. Tuttavia, non ritengono di assumersi la responsabilità di negare il voto al provvedimento di fronte alla crisi dei mercati europea, il cui intervento è essenziale per evitare un aumento dello *spread* fra i nostri BTP e i *Bund* tedeschi: elemento, questo, che aggraverebbe ulteriormente il nostro già pesantissimo debito. Certo, la questione è resa più complessa dal fatto che, avendo posto il Governo la fiducia sul maxiemendamento, secondo il nostro Regolamento il voto a favore della manovra si identifica con quello sulla fiducia al Governo. Per questo vogliamo dire alto e forte che il nostro sì non significa fiducia al Governo, che ha prima sottovalutato la gravità della crisi, abbandonandosi a un immotivato ottimismo e ha tenuto poi un atteggiamento incerto e contraddittorio sulle misure da prendere. E comunque noi attendiamo dall'Esecutivo il mantenimento dell'impegno all'abolizione con norma costituzionale delle Province, una richiesta, questa, avanzata da Ugo La Malfa nel lontano 1970 e che ha rappresentato sempre una costante programmatica dei Repubblicani. Per questo il nostro sì è ispirato oggi solo alla fiducia nell'Italia e a quel senso di responsabilità nazionale che ha sempre caratterizzato la storia del PRI,

sarebbe troppo facile indugiare ancora sull'approssimazione e sull'inadeguatezza dell'azione posta in essere dall'Esecutivo con questa manovra. Peccato, però, che queste percezioni siano ormai diffuse nell'opinione pubblica nazionale e internazionale, rischiando di assestare un altro colpo alla credibilità di tutto il sistema della democrazia rappresentativa, inducendo ancora altri a cavalcare l'onda dell'antipolitica,

Alla fine la manovra è stata varata nella sua compiutezza; i saldi terranno, perché l'intervento sull'IVA in qualche modo mette la toppa a un buco sempre più largo, se dietro questa toppa le difficoltà dell'Esecutivo sono gravissime e conclamate. Esse hanno impedito di affrontare i temi veri, quelli che il collega Del Pennino poco fa evocava, i nodi strutturali che stanno mettendo in grave difficoltà il nostro Paese, sia per quanto riguarda la finanza pubblica, che il sistema economico nel suo complesso.

confronti del nostro Paese, senza che noi riusciamo a reagire con una manovra seria, che affronti le questioni di fondo. Ma quali sono le questioni di fondo, signor Presidente, signori del Governo? Sono quelle che riguardano l'alleggerimento del peso della spesa pubblica e della pubblica amministrazione nel nostro Paese. L'emendamento sulla *spending review* può essere un'occasione: speriamo che sia utile. È un contributo dell'opposizione, come dall'opposizione è venuta la proposta sul tema della riforma della giustizia, che è stata inserita nel provvedimento.

la mancata previsione di un'imposta patrimoniale di impatto limitato sul piano percentuale, ma strutturale e non *una tantum*, che avrebbe garantito maggiore equità. Avrebbe garantito un cespite certo e, incrociata con altri meccanismi, avrebbe aiutato la lotta all'evasione perché avrebbe fatto individuare alcuni cespiti immobiliari molto rilevanti. Considero un errore non aver mantenuto un credibile contributo di solidarietà per redditi non così smisuratamente alti - oltre i 300.000 euro - con una pressione del 3 per cento, che è davvero una foglia di fico e che non produrrà alcun gettito se non salvare la coscienza a qualcuno. In ciò c'è davvero la cultura politica che impregna questa maggioranza, non è quella degli italiani, perché in essa prevale e domina un sentimento di iniquità sociale che è il segno distintivo di questa manovra. E quando avete utilizzato la lotta all'evasione come strumento tecnico per la copertura della manovra, la non credibilità di questo Esecutivo e di questo meccanismo ha reso quella scelta davvero infelice, perché per fare della battaglia all'evasione fiscale la scelta di fondo di un Governo occorre essere credibili, occorre che la *leadership* del Governo sia credibile attorno a questo tema. Per carità di Patria, non voglio evocare gli ultimi episodi che sono sulle pagine dei giornali ma che indicano costumi e comportamenti - personali, pubblici e privati - che tutto sono tranne che rigorosi ed eticamente corretti. Per fare simili scelte, per combattere la battaglia all'evasione fiscale occorre che l'esempio venga da chi governa questi processi, ma così non è stato. Ma la cosa più grave è la mancanza di scelte attorno alla crescita. Questo provvedimento manca di qualsiasi politica per la crescita, se non vogliamo limitarci ad evocare il tema delle liberalizzazioni accennate e delle privatizzazioni. Attorno a questo tema - che non può essere disatteso - ed alla dismissione del patrimonio pubblico,

il Paese e la sua comunità civile, e che invece aiutino qualcuno, ripercorrendo vecchie strade, magari quelle dell'inizio degli anni '90, in cui, sotto la pressione di una situazione economico-finanziaria difficilissima, quel processo di privatizzazione, piuttosto che favorire grandi *player* nazionali di tipo privato, ha determinato un indebolimento del nostro sistema produttivo, nonché la fragilità di alcune grandi strutture economiche che oggi sono oggetto

di far ritrarre lo Stato e la spesa pubblica corrente da quelle aree, garantendo in tal modo l'emergere di una società civile economica vitale e innovativa. È giusto così ma, dove è più debole la società civile economica, lo Stato deve fare un'opera virtuosa di accompagnamento e di stimolo all'innovazione ed allo sviluppo attraverso meccanismi seri come

in quelle condizioni sociali di debolezza, ove lo Stato ha spesso svolto il ruolo di ammortizzatore, ove questo ruolo oggi non può più essere svolto, lo Stato abbia una funzione di stimolo e di sviluppo attraverso criteri nuovi di virtuosità. Per concludere, la virtuosità che oggi ispira molti meccanismi di erogazione di risorse pubbliche agli enti locali non può essere il dato storico che registra dato storico che registra una differenza drammatica tra le zone del Paese. Occorrono meccanismi che invece premino le *performance* di miglioramento e che stimolino in modo educativo alla virtuosità. Queste iniziative vanno intraprese. Non le ha fatte l'Esecutivo. Andranno fatte. Forse dovrà farle un altro Esecutivo. A questo noi neghiamo la fiducia.

mi consenta innanzitutto di esprimere apprezzamento per l'impegno dei colleghi del Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud del Sud in sede emendativa e di confronto e di dibattito in Commissione; un impegno che ha portato ad affrontare e a migliorare alcuni interventi importanti e significativi. Mi riferisco a quelli ai quali hanno fatto riferimento nel corso del dibattito i senatori Fleres e Poli Bortone, che appunto sono intervenuti in discussione generale, e hanno ricordato l'obiettivo raggiunto, in convergenza con la maggioranza e con il Governo, di intervenire a tutela del Fondo per le aree sottoutilizzate, in particolare per le risorse destinate alla programmazione regionale, non per un rivendicazionismo meridionalista di maniera, ma per tutelare e difendere un interesse nazionale su cui c'è stata convergenza con il Gruppo della Lega, in direzione degli interventi e degli investimenti in termini infrastrutturali finalizzati allo sviluppo e alla crescita. Penso agli interventi su alcune misure sgradevoli, oltre che espressione di una cultura sbagliata rispetto alla pubblica amministrazione, e cioè all'intervento sulle tredicesime, che abbiamo sostituito, con un nostro emendamento, ferme restando le risorse, con un intervento mirato sulla responsabilità dei dirigenti. all'intervento sui Comuni e al Fondo per la progettazione per accompagnare i piani triennali dei Comuni, determinando quella capacità di fare banca-progetto che molte volte è fondamentale per attrarre investimenti e finanziamenti in direzione qualitativamente significativa. Penso al sistema di tracciabilità, al SISTRI, che è stato reintrodotto con il contributo fondamentale del nostro Gruppo. Ciò detto, doverosamente, per sottolineare e ribadire l'impegno dei senatori, di tutti i colleghi del Gruppo, signor Presidente, vorrei motivare il voto di fiducia che noi esprimiamo oggi attraverso alcune considerazioni ed alcune riflessioni molto pacate e serene, finalizzate innanzitutto a riportare una sorta di processo di verità nel dibattito e nel confronto che stiamo svolgendo e sviluppando da qualche settimana. Ricordo innanzitutto a me stesso che noi ci siamo trovati di fronte e ci troviamo ancora a vivere dentro un percorso di crisi con il quale dovremo fare i conti (è il caso di dirlo, di sottolinearlo e di ribadirlo), non soltanto dal punto di vista economico-finanziario, per lungo tempo, perché siamo dentro il tempo della crisi e dentro il tempo della crisi dobbiamo individuare quelle risposte, quell'innovazione, quella creatività per recuperare alla politica la capacità di rispondere ai nuovi problemi epocali che scandiscono il nostro tempo. allora ci siamo trovati, dentro questo percorso, ad un primo *step* fondamentale con la manovra di luglio, e qui vorrei ricordare ancora una volta il ruolo del Presidente della Repubblica, che sta sviluppando una funzione alta in termini politici, per quello che la politica significa in termini alti, non nella banalizzazione quotidiana che molte volte si determina. Il Presidente della Repubblica, di fatto, intervenne nel dibattito, lo ricordiamo tutti, quando alla presentazione della prima manovra emerse la polemica a proposito della spalmatura dei pesi e degli interventi concentrati essenzialmente nel 2013 e nel 2014. Il Capo dello Stato intervenne per dire, più o meno testualmente, che era sorpreso della sorpresa di una spalmatura temporale degli interventi, perché quella spalmatura temporale accompagnava la richiesta che in sede europea veniva al nostro Paese, che aveva già sviluppato una capacità d'intervento che comportava nel breve periodo solo un'esigenza di vigilanza e, nel periodo più lungo, cioè nel 2013 e nel 2014, la concentrazione degli interventi necessari a raggiungere l'obiettivo fondamentale del pareggio di bilancio. Dopo quella manovra si è innestata un'accelerazione formidabile che ha posto il traguardo, alzato l'asticella, ha determinato che l'obiettivo del pareggio di bilancio si configurasse e si anticipasse al 2013 e, in quell'ambito, si è sviluppata una nuova manovra che è restata sostanzialmente dentro il perimetro

di disorientamento rispetto alle scelte e all'assestamento della manovra. In particolare, quando si è prefigurata quella misura che era sostanzialmente una misura di classe che interveniva su quelli che erano i laureati e su quelli avevano assolto il loro dovere nei confronti dello Stato, vi è stato sicuramente un elemento di comunicazione sbagliato che ha creato disorientamento. Sarebbe però altrettanto intellettualmente, prima ancora che politicamente, disonesto non riconoscere che la manovra che oggi arriva al Senato è sicuramente una manovra rafforzata e migliorata rispetto alla credibilità circa il raggiungimento degli obiettivi e dei saldi. Questo anche perché è una manovra che interviene su alcuni elementi che determinano, nel caso dell'IVA, una capacità finanziaria forte e considerevole; nel caso del contributo e nel caso dell'intervento sul processo pensionistico delle donne, interventi di minore impatto dal punto di vista finanziario, ma altrettanto significativi ed importanti dal punto di vista simbolico. Che cosa è infatti accaduto in queste ore in termini politici? È accaduto che c'è stata una capacità di risposta rispetto alle esigenze che sono state poste in maniera autorevole dalle massime istituzioni nazionali, e non solo, che andavano nella direzione di intervenire - lo ricordo a me stesso - su due questioni

prima ancora che il tema di carattere finanziario, vorrei sottolineare il tema di carattere politico: di fronte alla sfida della sovranità, il Governo e la maggioranza hanno dato una risposta, a mio avviso, positiva e utile, che serve a dire con chiarezza che qualcuno sbaglia se pensa di far coincidere la via giudiziaria e la via finanziaria per ottenere non la salvezza dei conti e l'interesse della Repubblica, ma un modo per contrastare e mandare a casa un Governo che esprime, ancora oggi, la sovranità popolare e la maggioranza in Parlamento. Non è una questione solo di carattere finanziario, ma di carattere politico significativo e rilevante. Vorrei infine dire una cosa per

perché è legittimo il contrasto ed è legittimo il dissenso. Tuttavia, se ciò è sbagliato, lo è in entrambe le direzioni. È altresì sbagliato personalizzare la vicenda dell'articolo 8 8 e criminalizzare chi la pensa diversamente da chi legittimamente ha scioperato. È però altrettanto legittimo che ci sia un sindacato riformatore e che ci siano forze politiche che capiscono che la via della coesione sociale passa attraverso relazioni industriali improntate alla cultura della collaborazione e della partecipazione e non al tempo del conflitto e dell'antagonismo. finestra"). Vorrei richiamare molti di voi a una maggiore compostezza in Aula. Quest'Aula non è una zona di incontro per chiacchiericcio. È un'Aula del Parlamento. Mi spiace dover fare questo richiamo, in particolare modo perché siamo in diretta televisiva. E si continua....

siamo nel mezzo di una delle crisi economiche più gravi della storia della nostra Repubblica e il Governo si è presentato con la seconda manovra di emergenza in due mesi, e l'ha modificata almeno cinque volte. La domanda che ci poniamo, e che si pongono tutti gli italiani, è semplice: dopo tanta confusione, dopo tanti litigi nella maggioranza e nel Governo, tanti annunci e marce indietro, questa nuova manovra è all'altezza di ciò che sarebbe necessario? La nostra risposta negativa la esprimeremo con il nostro voto tra pochi minuti. Nel dibattito il senatore Baldassarri ha spiegato, da par suo, con quale serietà noi abbiamo avanzato una proposta di manovra fondata su misure responsabili, strutturali, capaci di rispondere in modo credibile a questa crisi che colpisce i conti pubblici, le imprese, le famiglie, tutti gli italiani: con misure serie di tagli della spesa per acquisti di beni e servizi e per i fondi perduti, da trasformare in crediti di imposta; con più impulso coraggioso per la crescita, a partire dalle liberalizzazioni nei servizi pubblici; con proposte efficaci per creare quel contrasto di interessi che permetta di ridurre l'insostenibile evasione fiscale; con misure europee sulla previdenza, da tradurre a vantaggio dei giovani e della conciliazione di lavoro ed esigenze familiari per le donne; con un taglio vero e immediato delle Province inutili. C'è però un tema colossale, politicamente colossale, che domina questa manovra e che il Governo vorrebbe nascondere. Il mio intervento vuol cercare di far capire anche agli italiani che ci ascoltano che con questo decreto si è definitivamente la lunghissima stagione delle vostre promesse sul taglio delle tasse. Gli infiniti ritornelli: taglieremo le tasse; ci saranno meno tasse per tutti; riformeremo subito (e finalmente) un fisco troppo pervasivo, con tasse troppo alte per chi le paga e un'evasione tanto diffusa da essere un sistema immorale. Ed ancora: ridurremo le aliquote, porteremo la pressione fiscale sotto il 40 per cento. È tutto finito, e per sempre. Solo nelle due manovre di luglio e agosto il Governo Berlusconi ha fatto ricorso a un diluvio di maggiori tasse: l'imposta di bollo sul deposito titoli, l'aliquota IRAP per banche e assicurazioni, i coefficienti di ammortamento, le nuove tasse sui giochi, le accise sulla benzina e sui tabacchi, le maggiorazioni sulle rendite finanziarie, un'ulteriore delega sui giochi e le accise sul fumo, gli studi di settore, l'addizionale IRES sul settore energetico, la tassa sul *money transfer*, il cosiddetto contributo di solidarietà. Adesso, arriva il colpo grosso dell'aumento dell'IVA: un'imposta sui consumi è quanto di più vecchio esista. Colpisce in modo regressivo le fasce sociali più deboli e, ancora una volta, quelle piccole imprese, quei commercianti e artigiani che pagano le tasse. A proposito, perché non avete accolto il nostro emendamento, pur approvato dalla Commissione bilancio, che prevedeva che alle piccole imprese si consentisse di recuperare con accordi con le banche i crediti che vantano verso le pubbliche amministrazioni? È stato un errore grave, è stata una mancanza imperdonabile. Continuo: c'è una fantascientifica previsione di 1,5 miliardi di euro in più dalla lotta all'evasione. Certo, se la mano sapiente del Tremonti fiscalista si applicasse, come ha fatto per la raffica di condoni e di scudi fiscali, ad esempio per ridimensionare l'uso del contante - ma, ahinoi,

Non è finita qui, signor Presidente. Il Governo del "meno tasse per tutti" ha deciso di tagliare una forte componente della spesa per gli enti locali; consapevole dell'insostenibilità di questa scelta per i servizi che ogni cittadino, nella sua vita, deve ottenere nel proprio Comune, ha sbloccato le imposte addizionali. vuol dire che avremo altri miliardi di tasse locali, oltre a tariffe più salate, da parte di enti che devono in qualche modo evitare la bancarotta. Non è finita, ancora. Se la delega sull'assistenza sociale - tagli per 4, più 16, più altri 20 miliardi nel triennio - non andrà in porto, porto, tutte le risorse saranno ricavate da tagli su agevolazioni e deduzioni fiscali (che colpiranno i redditi più bassi in modo drammatico),

L'effetto recessivo di queste manovre, senza misure strutturali, complicherà ancora di più il cammino della Nazione, perché tutte le cifre, a partire da quelle della crescita economica, sono destinate a far saltare le previsioni e ad imporre nuove manovre, nuovi sacrifici inutili, nuove riduzioni della crescita, in una terribile spirale. Questo è il fallimento conclusivo del vostro Governo. Certo, il *Premier* ha ingannato gli italiani per lunghi ed estenuanti anni. Oggi lo *slogan* preferito della maggioranza è «così fan tutti». Per cercare di tenere buoni gli italiani, voi amate dire che «la crisi c'è dappertutto», «le misure sono dure allo stesso modo in mezzo mondo». Non è vero: la crisi è più grave in Italia, come noi invano sosteniamo da molto tempo. Per questo avevamo previsto che le vostre manovre sarebbero state inadeguate e, dunque, dannose. Abbiamo proposto misure serie, credibili, e ve le abbiamo messe a disposizione, ma voi non le avete volute accogliere, in questo purtroppo aiutati da opposizioni di sinistra che anch'esse temono misure impopolari sui tagli di spesa o sulla previdenza. Noi vi diciamo che non sarebbero state impopolari, perché gli italiani sanno benissimo che, a partire dal taglio dei costi impropri ed ingiustificati della politica, su cui abbiamo presentato proposte doverose e giuste, fare dei sacrifici ben studiati oggi può permettere di salvare il Paese, di ricreare sviluppo Gli italiani sanno che rinviare le misure per la crescita economica, per tagliare interessi non trasparenti e sprechi inaccettabili, significa aggravare la situazione, lasciare a chi verrà dopo di voi un fardello terribile da far portare

Da qui, con l'effetto di queste manovre, l'Italia sarà seconda solo al Belgio, al massimo della pressione fiscale di tutta l'area dell'euro. Presidente, questa è la definitiva rottura delle promesse fatte da Berlusconi agli italiani. Proprio noi, del Gruppo Per il Terzo Polo, formato dai senatori di ApI e FLI, possiamo dirlo a testa alta, perché si incontrano in questo Gruppo i senatori che hanno seguito il presidente Fini nella formazione di Futuro e Libertà, che avevano aderito all'idea di un centrodestra coerente con un'idea liberale, ancorata ai principi di uno Stato di diritto fondato su legalità e responsabilità, assieme a noi senatori di Alleanza per l'Italia. Il nostro è un Gruppo che guarda oltre alla stagione di queste promesse mancate. Noi, insieme a UDC e MPA, vogliamo costruire un Governo di larga responsabilità, che affronti la crisi il concorso di tutte le migliori energie della politica, della società civile e produttiva: un Governo politico. Domani, costruire coalizioni di Governo che dicano la verità agli italiani e che si concentrino non sulle esigenze della propaganda, ma sulle soluzioni per far tornare a crescere l'Italia. Non avete voluto votare i nostri emendamenti. Io sono convinto che molti senatori del PdL, la parte critica che condivide queste riflessioni, avrebbero potuto votarli, perché perché oggi i problemi la maggioranza li ha al suo interno rispetto alle proposte razionali,

Dovrete presentarne un'altra, dopo che avrete bruciato miliardi, dopo che avrete depresso il Paese, dopo che avrete mandato a picco, colleghi della Lega, l'illusione di un federalismo ormai ridotto a tagli selvaggi per gli enti territoriali, con più burocrazia, più imposte e tariffe più alte. Presidente, si conclude qui qualcosa di più: una stagione politica. Il Governo è senza guida. L'economia è senza guida.

a meno di due mesi dalla precedente dimostra che avete sbagliato tutto. Ed oggi volete curare un malato sotto la tenda ad ossigeno con l'aspirina! *(Applausi il Presidente del Consiglio rassicurava la Camera sulla solidità dei fondamentali economici dell'Italia, salvo poi smentire se stesso, come d'abitudine, appena due mesi più tardi.

economico-finanziario, senza che la maggioranza abbia provato, insieme al Governo di riferimento, se non a risolvere un problema, almeno ad avviarlo a soluzione.

L'Italia dei Valori aveva presentato degli emendamenti puntuali che partivano dalla riduzione del 20 per cento dell'indennità parlamentare, dalla soppressione immediata dei vitalizi, che costituiscono dei privilegi che gli italiani ormai mal sopportano. Avevamo presentato, ancora una volta, l'emendamento per la soppressione delle Province. Adesso si rinvia ad un disegno di legge costituzionale, quando il PdL ha affossato alla Camera un analogo disegno di legge che l'Italia dei Valori aveva presentato. l'adozione di misure eque e strutturali per la riduzione del debito pubblico che, lo ripeto, durante la vostra gestione, signori del Governo, è aumentato. ci sono misure per la crescita, né misure per contrastare efficacemente la corruzione e l'evasione fiscale. D'altra parte, cosa potevano aspettarsi gli italiani da un Presidente del Consiglio imputato per frode fiscale e corruzione? Questi sono i dati e non si può più imbrogliare il Paese; non potete promettere cose che sapete non manterrete mai. Vi siete inventati manovre usa e getta, annunciate e strappate, le manovre cosiddette a tempo determinato, buone al mattino e scadute la sera come gli yogurt. Vi siete certamente coperti di ridicolo, ma quello che mi preoccupa è che ci siamo coperti e che avete coperto gli italiani all'estero di ridicolo agli occhi del mondo. Siete fuori rotta per questo ponete per la quarantanovesima volta la questione di fiducia, quando il segretario del PdL soltanto lo scorso 4 settembre l'aveva il Ministro degli affari esteri l'aveva ritenuta fuori dall'orizzonte, lo stesso collega capogruppo del PdL aveva dichiarato che la manovra sarebbe stata approvata entro mercoledì e che all'orizzonte non vi era una questione di fiducia.

avete detto che non avreste mai messo le mani nelle tasche degli italiani, ma è quello che state facendo, come ci ricorda la Corte dei conti e come ci ricordano le proteste delle Regioni e degli enti locali. Bugiardi, in malafede? Questo non spetta a me ma agli italiani capirlo. Certo, ve la prendete sempre con gli stessi colpendo i lavoratori, le famiglie, i pensionati ma lasciando al riparo evasori, speculatori, truffatori. Date la colpa agli speculatori, ma gli speculatori internazionali sono solo l'effetto; la causa di questo disastro è il Governo Berlusconi-Bossi-Tremonti, e gli italiani lo stanno capendo sulla loro pelle. La vostra inutile sicumera, il vostro immobilismo, il vostro agire tardi e male ci hanno portato a questo livello. Adesso grandina e voi avete aperto un ombrello di carta. credibilità è ormai inesistente e irrecuperabile. Un Governo, dicevo prima, che cambia la sera quel che aveva deciso la mattina. Come ci si meraviglia se nel mese di giugno i depositi dei conti correnti bancari sono scesi di 23,4 miliardi? È la conseguenza della paura e

il problema è che il Governo è inadeguato. Noi lo diciamo da tempo che è arrivato al capolinea. Non bastano endovene di chiacchiere. Il Paese ha bisogno di fatti e voi non siete nelle condizioni di realizzare alcunché nell'interesse degli italiani. Voglio chiudere ricordando la manifestazione di ieri. Noi abbiamo deciso di sfilare, dicendo no alla fiducia che il Governo ha chiesto, con lo Statuto dei lavoratori in mano.

che dovrà venire subito dopo di voi, toccherà invece infondere passione, voglia di realizzare, serenità, mandando fuori dal Parlamento e dal Paese inquisiti, condannati, truffatori e cricche

Signor Presidente, colleghi senatori, noi siamo decisamente contrari a questa ennesima e tardiva manovra economica, e ancora una volta vi negheremo la fiducia. Per senso di responsabilità e per la credibilità internazionale dell'Italia non ci siamo opposti né ci opponiamo ai tempi rapidi che sono stati imposti per la sua approvazione e non contestiamo l'ennesimo ricorso al voto di fiducia, perché sappiamo che domani si terrà un incontro importante della Banca centrale europea, dal quale può dipendere molto del futuro economico dell'Italia. Facciamo così, anche se abbiamo tanti buoni motivi per polemizzare con voi, sia per i metodi che avete usato che per le scelte che avete fatto. Metodi e scelte che hanno portato la politica italiana al punto più basso di credibilità e di autorevolezza mai raggiunto negli ultimi anni. Solo grazie agli interventi autorevoli del Capo dello Stato teniamo ancora botta e noi, da opposizione leale, ci assumiamo la responsabilità di assecondare questo modo di procedere solo ed esclusivamente per il bene del Paese. Se siamo accondiscendenti nel metodo, non lo siamo, però, nel merito, perché questa è e resta una manovra sbagliata; una manovra fatta in fretta, come ha detto il ministro Tremonti, e male. In fretta, perché, anche in presenza delle oggettive difficoltà politiche ed economiche dell'Europa e degli Stati Uniti, è frutto della sottovalutazione della crisi operata dal Governo e dalla maggioranza. Basti pensare alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che, fino a due mesi fa, escludevano categoricamente ogni problema per l'Italia. Fatta male, perché risolve più i problemi della maggioranza che quelli dei cittadini italiani. Le misure che essa contiene sembrano, infatti, una strana specie di *puzzle* dalle forme confuse, che cerca di evitare accuratamente di colpire gli interessi di questo o quel partito del centrodestra. Basta dare un'occhiata alla corsa ad ostacoli che avete fatto dal 12 agosto fino ad oggi, che vi ha costretto a cambiare il testo della manovra almeno cinque volte. Siete partiti con un forte taglio di risorse agli enti locali, con l'abolizione delle Province al di sotto dei 300.000 abitanti, salvando però quelle politicamente vicine alla Lega e simpatiche al ministro Tremonti; con la soppressione dei piccoli Comuni il taglio di 54.000 poltrone, scaricando ingiustamente sui sindaci e sugli amministratori delle piccole comunità i tagli dei costi della politica, quasi che fossero loro la casta. Siete arrivati ad una riduzione dei tagli, al mantenimento di tutte le Province (perché sappiamo tutti che quando non si vuole fare una cosa si rinvia ad un disegno di legge costituzionale) e al mantenimento di tutti i Comuni. Siete partiti colpendo ingiustamente il ceto medio italiano (e in modo particolare le famiglie monoreddito con più figli) con il cosiddetto contributo di solidarietà per chi guadagna più di 90.000 euro l'anno e siete arrivati ad alzare la soglia del reddito a 300.000 euro con un'aliquota però abbastanza irrisoria. Sicché il ministro Tremonti dovrà rassegnarsi, perché anche questa volta i ricchi non piangono. Grazie alle nostre proteste e alle battaglie parlamentari dell'UDC e del Terzo Polo è stata cancellata questa tassa odiosa che colpisce solo chi le tasse le paga fino in fondo, anche se l'avete mantenuta, ingiustamente, per i pubblici dipendenti e per i pensionati. Non sapendo cosa inventarvi, vi siete sbizzarriti nel sopprimere le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, salvo poi fortunatamente ripensarci. Siete partiti con l'idea (sbagliata) di non intervenire sulle pensioni; in corso d'opera ci avete ripensato e volevate colpire i lavoratori che con i propri risparmi si sono riscattati gli anni di laurea ed il servizio militare, allungando loro il periodo di anzianità. Dopo aver abbandonato nottetempo questa proposta oscena, siete arrivati ad un minianticipo del pensionamento femminile, che fino al 2015 non produrrà alcun effetto positivo sul bilancio dello Stato. In poche parole, tra una dichiarazione solenne dell'onorevole Alfano sul fatto che occorreva intervenire sulle pensioni per salvare gli enti locali e una pernacchia di risposta dell'onorevole Bossi, siete riusciti nel miracolo di inserire il capitolo pensioni nella manovra senza alcun effetto positivo e concreto. Siete partiti con l'idea che non bisognava aumentare l'IVA (perché questo Governo mai avrebbe messo le mani nelle tasche degli italiani; perché l'aumento dell'IVA avrebbe ridotto i consumi danneggiando le imprese e commercianti; perché avrebbe aumentato l'inflazione; perché - dice la Lega - è una tassa contro la Padania; perché doveva essere l'ultima carta da giocarsi per fare una buona riforma fiscale) e siete arrivati ad aumentarla di un punto, non per favorire la crescita riducendo le tasse sul lavoro e sull'impresa, ma perché non vi sono tornati i conti dopo la soppressione del contributo di solidarietà. A questo riguardo, signor Presidente, mi dispiace dover sottolineare che un Governo che mente sui conti pubblici, un Governo che fa il gioco delle tre carte con le coperture di spesa, un Governo che un giorno sostiene in Commissione bilancio che i quattro miliardi che mancano per la soppressione del contributo di solidarietà sono coperti con le nuove norme contro l'evasione fiscale e il giorno dopo propone in Parlamento l'esatto contrario, aumentando l'IVA dell'1 per cento e diluendo le pene per gli evasori, non è un Governo serio, e non è un Governo del quale, prima ancora dei mercati e delle principali istituzioni finanziarie europee, si possano fidare i cittadini italiani. Perché gli italiani sono persone serie e sono pure disponibili a fare sacrifici. Li hanno sempre fatti nei momenti più difficili della storia del nostro Paese, ma vogliono sapere come e per cosa li fanno. Se un Governo non ha il coraggio e l'onestà di spiegarlo in maniera chiara e trasparente, non ha titolo morale, prima che politico, per guidare un Paese. Avete avuto il coraggio di colpire le cooperative per un miope calcolo politico e non perché ve ne sia un reale vantaggio fiscale, non comprendendo che in un momento di crisi economica e sociale, in un momento in cui la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è ai più alti livelli in Europa queste strutture possono offrire opportunità di lavoro e di solidarietà sociale, oltre ad essere uno strumento di sostegno alla nostra economia. In poche parole, nel tentativo di rimediare ai ritardi e alle inadempienze con cui avete affrontato la crisi, avete messo su in fretta e furia una manovra confusa e disordinata, che certamente - nessuno lo nega - potrà garantire il pareggio di bilancio nel 2013, ma che non consentirà all'Italia di uscire dalla crisi e di migliorare la propria condizione economica e sociale. Signor Presidente, il Fondo monetario internazionale sostiene ancora oggi che il nostro Paese non cresce e che il prossimo anno crescerà ancora meno del previsto. I principali problemi che abbiamo sono legati alla crescita lenta della nostra economia e all'enorme debito pubblico, che condiziona pesantemente la compravendita dei nostri nostri titoli di Stato sui mercati finanziari. Se non incidiamo profondamente su questi due problemi non solo non saremo nelle condizioni di garantire in maniera stabile il pareggio di bilancio dopo il 2013, ma rischiamo di aggravare la condizione economica e sociale del Paese. L'UDC e il Terzo Polo hanno fatto proposte chiare e nette su questi problemi, che però avete ritenuto, sbagliando, di non prendere in considerazione. Se ci aveste prestato attenzione - come avete fatto per alcune misure in materia di giustizia civile, di tassazione delle rendite finanziarie, di cancellazione del contributo di solidarietà per il ceto medio, probabilmente questa manovra sarebbe stata più equa, perché non avrebbe colpito così violentemente le famiglie italiane, che pagheranno più tasse statali e locali e avranno meno servizi e avrebbe rilanciato la crescita economica del Paese. Pensiamo alle nostre proposte sul Mezzogiorno, sulla banda larga, sulla velocizzazione della spesa regionale legata ai fondi per le aree sottoutilizzate, alle nostre proposte sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali, alle dismissioni del patrimonio immobiliare per l'abbattimento del debito, alla riduzione della spesa corrente in rapporto al PIL, alla vera lotta all'evasione fiscale attraverso il contrasto di interessi, alla riscrittura di un nuovo patto generazionale tra vecchi e giovani perché, senza toccare i diritti acquisiti, un padre e una madre accetterebbero volentieri di andare in pensione a 65 anni o con quarant'anni di contributi pur di vedere il proprio figlio disoccupato prendere un posto di lavoro o, se precario, vederlo sereno con una vera e propria pensione. La paura e la miopia in realtà vi hanno paralizzato. Tutto questo ci preoccupa e non poco, perché il Paese ha bisogno di riforme strutturali e di una classe politica generosa e coraggiosa. Di fronte ad un'aggravarsi della crisi, che non ci auguriamo, di fronte alla necessità di dover fare quelle scelte che, per paura, avete fino ad oggi irresponsabilmente rinviato, siamo convinti che voi non sarete nelle condizioni di farcela, perché o realizziamo condizioni di unità e di solidarietà tra le forze politiche responsabili, di maggioranza e di opposizione, oppure quei provvedimenti che sono necessari all'Italia per farla crescere, per rendere i nostri conti pubblici credibili in Europa e tra gli investitori internazionali, per collocare senza difficoltà i nostri titoli di Stato, non vedranno mai la luce. Con la vostra sindrome di autosufficienza non si governa più il Paese. Cambiare è necessario. Prima ve ne rendete conto e meglio sarà per l'Italia.

è in atto una crisi mondiale che coinvolge tutte le grandi democrazie occidentali e che ha portato una drammatica instabilità sui mercati. È una crisi senza precedenti. In questi mesi abbiamo visto cose impensabili fino a poco tempo fa. La crisi ha colpito tutti, anche quei Paesi che ci venivano portati ad esempio per la loro crescita economica, come la Spagna e l'Irlanda, ora in ginocchio e in piena recessione. La Francia, la Gran Bretagna e la Germania hanno dovuto varare manovre economiche aumentando le tasse. Gli Stati Uniti d'America sono stati sull'orlo del fallimento, evitato all'ultimo momento dal presidente Obama. Non solo. Le Borse di tutto il mondo hanno perso miliardi di capitalizzazione. In questo drammatico contesto si è trovato anche il nostro Paese, con l'aggravante di avere fra l'altro il più alto debito pubblico d'Europa, il terzo nel mondo. Nonostante questo, finora siamo riusciti a resistere, a tenere, anche grazie - è giusto ricordarlo - ai provvedimenti di contrasto alla crisi fatti dal Governo, sostenuti dal ministro Tremonti che, fin dall'inizio di questa legislatura, ha pensato in maniera lungimirante e prudente a tagliare sprechi e spese dello Stato come mai nessuno in passato. Oggi siamo chiamati ad approvare una nuova manovra economica e siamo anche consapevoli che questo politicamente non ci farà certo guadagnare consensi. Sarebbe tutto più facile stando all'opposizione, ma non potevamo certo lasciare alla sinistra o a qualche Governo tecnico il compito di far quadrare i conti di questo Paese luogo perché non ci sarebbero mai riusciti e poi perché sicuramente avrebbero penalizzato ulteriormente il nostro territorio. Stando al Governo e soprattutto grazie alla determinazione di Umberto Bossi, siamo riusciti comunque a non toccare le pensioni di anzianità, evitando di penalizzare soprattutto i lavoratori del Nord. il decreto, a reperire quasi due miliardi a favore degli enti locali. Siamo riusciti ad evitare ulteriori tasse, imponendo un contributo a chi utilizza i cosiddetti *money transfer*. Abbiamo chiesto e ottenuto un contributo di solidarietà per i ricchi, per chi ha un reddito superiore ai 300.000 euro all'anno. Per quanto ci riguarda, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, chi più guadagna più aiuta. *(Applausi

introdotto norme antievasione contro chi, negli anni, si è arricchito senza pagare le tasse, intestando auto, *yacht* e immobili di lusso a società di comodo. Abbiamo così colpito i grandi evasori, che sono i veri nemici dello Stato, e non certo i piccoli artigiani, i commercianti e gli imprenditori che con fatica tengono aperte le loro attività. Siamo intervenuti sui costi della politica, raddoppiando il contributo di solidarietà per i parlamentari e tagliando migliaia di poltrone. Nessuno ci era mai riuscito in passato. Lo ricordo soprattutto ai ai colleghi dell'opposizione, che hanno occupato poltrone prestigiose nel Governo Prodi 2006-2008, rimasto alla storia non per quello che ha fatto, ma per il *record* di poltrone che aveva al Governo, con 103 tra Ministri e Sottosegretari. Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? In un contesto meno conflittuale forse sì, ma non si poteva certo fare più velocemente. La prima cosa che gli investitori internazionali ci chiedevano erano tempi rapidi per l'approvazione. In tre settimane, in pieno agosto, siamo riusciti a fare una manovra che in altri tempi avrebbe richiesto mesi e mesi di tempo. In questo senso voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio per il lavoro fatto in Commissione. un altro tema. Gli investitori internazionali, che sono poi coloro che comprano i nostri BOT e sostengono - dunque - il nostro sistema economico, ci chiedevano un minimo di coesione nazionale. Un Paese serio, in un momento di difficoltà, dovrebbe smetterla con le polemiche interne e unirsi intorno al proprio Governo, dando consigli e aiutandolo. Questo, purtroppo, non è avvenuto. I giornali nazionali hanno fatto a gara nello sparare contro il Parlamento, alimentando l'antipolitica. Confindustria e sindacati sono stati capaci solo di lamentarsi, ognuno impegnato a difendere il proprio orticello, incurante dei problemi degli altri.

massimo è stato raggiunto ieri, con tutti i vertici del Partito Democratico in prima fila ai cortei di protesta della CGIL, insieme a Nichi Vendola e a Rifondazione Comunista. Bersani e cara senatrice Finocchiaro, i problemi di questo Paese non si risolvono cantando «Bella ciao» dal palco! Se si volevano rassicurare i mercati, peggio di così non si poteva fare. La speranza, comunque, è l'ultima a morire e io spero che nei prossimi giorni il senso di responsabilità di tutti prevalga sulla ricerca di visibilità e che in Parlamento si possa trovare più unità e coesione almeno sui temi più rilevanti, anche perché lo scontento nella popolazione è ormai generalizzato e colpisce tutti. Per fare un esempio, sempre ieri a Genova, durante un corteo della CGIL, l'Inno d'Italia è stato sommerso dai fischi dei partecipanti. Hanno dovuto interromperlo.

Il disagio nei confronti di questo Stato è sempre più forte e abbraccia tutte le classi sociali. Al Nord, in Padania - ve lo posso assicurare - ormai è incontenibile.

vogliono vedere annientato il centralismo romano e le cricche di Stato, ed è quello che noi dobbiamo fare in Parlamento. Dobbiamo procedere con le riforme istituzionali, dobbiamo modernizzare il Paese, dimezzando il numero dei parlamentari, superando il bicameralismo perfetto con l'istituzione del Senato federale e, allo spesso tempo, dobbiamo decentrare i Ministeri per collegare e avvicinare lo Stato al territorio. I tempi per approvare queste riforme prima della fine della legislatura ci sono e vedremo in Parlamento chi sarà disposto ad accettare questa sfida. Oggi il Gruppo della Lega Nord Padania approverà questa manovra. Il nostro è un voto convinto.

serviranno a non far saltare anche il sistema economico del nostro Paese, mettendo a rischio risparmi delle famiglie, imprese e posti di lavoro. Una cosa, però, deve essere chiara a tutti. A Nord, in Padania, tutti sanno che questa crisi non ci avrebbe colpito così duramente, se le altre Regioni italiane negli anni si fossero comportate come le nostre. *(Commenti dai banchi del PD).* La Padania, che è l'area più produttiva d'Europa, oggi soffre per colpe non sue

Con la norma che il Governo intende inserire in Costituzione, che impone l'obbligo del pareggio di bilancio, e con il federalismo fiscale, ognuno dovrà fare la propria parte, faccio degli esempi: se a Napoli non saranno in grado di raccogliere i rifiuti, non ci penseremo più noi; se le Regioni del Sud sforeranno i loro bilanci sanitari, dovranno ripianarli usando le proprie risorse; se la città di Roma farà ulteriori debiti, dovrà arrangiarsi. Questo varrà per tutti. *(Commenti dai banchi del PD).* Tutti, al Nord, al Centro e al Sud, saranno costretti a spendere quanto hanno in cassa: in questo modo elimineremo gli sprechi e le spese inutili del passato. Cari colleghi, e concludo, il mondo è cambiato e lo deve fare anche il nostro Paese. Ora serve serietà e rigore, e tutti ci dobbiamo rimboccare le maniche.

signori senatori, permettetemi di non tener conto di questo "comizietto" della Lega Nord sulla Padania. invece di ricordare che nessun italiano, nessun cittadino europeo ha mai visto nulla di così grave quanto ciò che sta accadendo in Italia in questi mesi, mai visto un Governo e una maggioranza affrontare con tanta incapacità, tanti annunci e tante retromarce una crisi che mette a fortissimo rischio il nostro futuro. Sul contenuto caotico di questa manovra resta poco da dire che non sia già stato detto in discussione generale dai senatori del Partito Democratico, che hanno illustrato carenze e contraddizioni in materia di riforme di equità, crescita, Mezzogiorno, evasione fiscale e licenziamenti. Né c'è nulla da aggiungere a quel che è stato scritto dai giornali italiani e stranieri. Abbiamo persino sentito un Nobel americano per l'economia chiamare «buffone» il nostro Presidente del Consiglio prestigiose testate definire «una buffonata» la manovra, mentre da parte della maggioranza non c'è stata nessuna reazione, nonostante fosse stato offeso il nostro Paese. Adesso aspettiamo di conoscere il giudizio del presidente Schifani su questo ennesimo voto di fiducia, visto che nelle ultime settimane tante volte lo aveva escluso, addirittura lo aveva demonizzato. La decisione di porre la fiducia è del Governo, ma coerenza vorrebbe che il Presidente del Senato ribadisse pubblicamente la sua contrarietà. Presto ci accorgeremo - è stato già ricordato - che questa manovra non basta e che per l'insipienza del Governo l'Italia sarà costretta ad un'altra manovra, purtroppo più dura e più feroce. In un saggio recente sulla crisi il professor Guarino ha chiesto di conoscere quale livello di crescita del PIL sia previsto dopo le manovre di luglio e di Ferragosto. Quella del professor Guarino è una domanda retorica, perché egli sa bene che l'effetto delle due manovre sulla crescita sarà nullo. Il Governo italiano sta impiegando 90 miliardi senza nessuna misura strutturale, strutturale, senza investire sullo sviluppo, senza nessuna strategia. E la crescita quindi sarà pari a zero. Non c'è quindi da stupirsi del panico di quegli economisti ed imprenditori che a Cernobbio hanno constatato l'indifferenza di molti Ministri italiani per la gravità dei rischi che l'Italia sta correndo. Purtroppo qui in Senato non ci meravigliamo, perché è stato Berlusconi a sostenere un mese fa in Parlamento che la nostra economia è solida e che la colpa è tutta dei mercati. E questa manovra è figlia di quest'assenza di consapevolezza. È figlia delle tensioni con Tremonti, degli egoismi di Bossi e degli scontri dentro la maggioranza. I mercati lo hanno capito. Hanno capito che l'Italia è molto malata e non riesce a crescere perché da troppo tempo non è governata. I mercati sanno che senza crescita il nostro debito, di cui ha parlato poco fa il presidente Marini, non diminuirà mai. I Governi europei, le opinioni pubbliche, i mercati, i grandi banchieri internazionali conoscono i comportamenti e la natura di Berlusconi e sanno che le sue follie sono un pericolo per l'Europa e per l'euro, e hanno deciso di opporsi come possono a questo disastro. Ed è questo diffuso giudizio politico negativo che fa dell'Italia l'area di maggior rischio per l'Europa. I mercati ci mandano a dire che le manovre senza riforme non possono risolvere i problemi. I continui tonfi delle borse e le continue impennate dello *spread* non sono né episodi isolati, né frutto della cattiveria della speculazione. Sono il segno che a furia di tener buoni Bossi e Scilipoti si sopravvive per qualche settimana, ma si uccide l'Italia. L'Italia è l'anello debole di una crisi che ha colpito l'Occidente. E la ragione di questo cataclisma non è quell'orologio rotto dei mercati di cui ciancia Berlusconi, ma la miopia delle azioni dell'uomo. Non siamo stati capaci di comprendere i pericoli di una crescita fondata sul troppo debito e su mercati senza regole. La globalizzazione non governata ha portato nel mondo non solo ricchezza, ma anche squilibri e tensioni. Ed allo stesso modo l'illusione di un mercato senza regole che ci facesse crescere di più ha prodotto quell'economia del debito che ci sta strozzando. E l'idea del Governo di riscrivere nell'articolo 41 della Costituzione che d'ora in avanti è tutto permesso è la prova provata che nemmeno la gravità della crisi è riuscita a mettere nella testa di Berlusconi che il mercato, se ben regolato, può essere un grande motore di sviluppo, ma senza regole e controlli è uno strumento di distruzione. D'altra parte, Berlusconi ha spesso coltivato i suoi interessi personali proprio dietro lo schermo dell'ideologia fondamentalista e fallimentare di un mercato senza regole. Quella che stiamo attraversando, signor Presidente, è molto più di una gravissima crisi finanziaria. È l'inizio di una fase di grande cambiamento dei nostri modelli di vita e dei nostri ritmi di sviluppo. È un cambiamento epocale, forse il più profondo nella storia dell'uomo. Al termine di questo processo ci saranno nuovi equilibri tra gli Stati, grandi mutamenti nel pensiero politico e nelle relazioni sociali e il mondo comprenderà che lo strapotere della finanza creativa deve cedere il passo ad una forte rivalutazione del mondo del lavoro e dell'economia reale. Se vogliamo benessere e sicurezza sociale per i nostri figli, leviamoci dalla testa di poterli ottenere con l'economia di carta dei *subprime* e dei derivati. Il futuro si costruisce con il sapere, con il lavoro, con le fabbriche e con la terra. *(Applausi il punto centrale del processo in atto. Il Partito Democratico lavora per unire il nostro Paese e Berlusconi ha lavorato finora per dividerlo e per spaccarlo. Con le gravi lesioni allo Statuto dei lavoratori imposte con l'articolo 8 della manovra, il Governo ha mostrato di non aver compreso che senza una forte coesione nazionale noi non usciremo mai dalla crisi. I danni di una politica di divisione sarebbero molto pesanti anche in tempi normali, ma oggi alimentare le fratture del mondo del lavoro è una provocazione irresponsabile. Negli ultimi tre anni non c'è stato un solo atto del ministro Sacconi che avesse come obiettivo la coesione e l'unità; al contrario, non si contano gli atti e le iniziative tutti di divisione e di rottura. Chiamiamola con il suo vero nome, questa vicenda dell'articolo 8: è una risposta maligna alla firma unitaria del 28 giugno. È un atto che serviva a cancellare gli effetti di una unità così faticosamente ritrovata. Sono tantissimi i parlamentari della maggioranza di centrodestra che hanno capito in quale baratro l'Italia sta sprofondando, sono veramente tantissimi, e anche loro, come noi dell'opposizione, sanno che nessuna manovra, qualunque ne sia il contenuto, può rassicurare i mercati se il Presidente del Consiglio è giudicato inaffidabile, ricattabile e addirittura inavvicinabile. Quella mondiale è una crisi di debito e di mercati non regolati, ma quella italiana è tutto questo ma, come ha ben detto questa mattina il senatore Morando, è anche crisi di fiducia, e di questo pesante sovrappiù di sfiducia la responsabilità è tutta del Presidente del Consiglio. L'Italia non è quel Paese che Berlusconi, parlando con Lavitola, ha definito con volgarità: siamo un grande Paese, siamo un grande popolo e se saremo capaci di restare uniti, se non permetteremo a nessuno di dividerci, ce la possiamo fare. Ma se vogliamo iniziare la ricostruzione, se vogliamo liberare le nostre energie positive, c'è un ostacolo che va rimosso, e mi appello ai parlamentari che sinora hanno sostenuto il Governo, ma che vogliono bene all'Italia. Ad un grande italiano morto nei giorni scorsi, Mino Martinazzoli *(Applausi)* capitò di dire qualcosa capitò di dire qualcosa che descrive perfettamente la condizione dell'Italia di oggi. Diceva Martinazzoli: «La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è la rotta, ma ciò che mangeremo domani». Signori senatori, cacciamo il cuoco di bordo.

il valore complessivo delle manovre attuate durante l'estate dal Governo, considerando le misure attive e quelle nelle deleghe, è probabilmente intorno ai 100 miliardi di euro. L'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 è da considerare storico. Per trovare un precedente analogo dobbiamo risalire al 1876. Possiamo dire che il pareggio di bilancio è il vero modo per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia con i fatti e non soltanto con le parole. L'obiettivo è il bene comune. L'impatto di manovre di questo tipo, in altri tempi, avrebbe costretto alla resa qualsiasi Governo, noi stiamo invece superando queste prove,

Per affrontare prove di questo tipo serve un Governo con una maggioranza coesa e non confusa, dove le contraddizioni avrebbero impedito ogni decisione. Nel mondo tutti fanno manovre; non so se sia anche questa colpa di Berlusconi. Negli Stati Uniti, nei giorni scorsi, le agenzie di *rating* hanno bocciato in maniera clamorosa le politiche economiche del presidente Obama e, a dimostrazione di quanto il mondo sia preda di sconvolgimenti, il presidente Obama ha deciso di portare davanti alla Corte federale J. P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank e tutti gli altri istituti per la responsabilità della crisi che tre anni fa vide il fallimento di Lehman Brothers. Lo stesso Obama ha dovuto rinunciare alle politiche ambientaliste, che gli avevano prodotto così tanto consenso, a dimostrazione che molti cambiano l'agenda del mondo e non è certamente colpa

il presidente Sarkozy è rientrato dalle ferie e ha rivisto i conti pubblici francesi. In Germania il PIL nel il PIL nel mese di agosto si è fermato e quella che era la locomotiva europea vive giornate molto difficili. Voglio anche consigliare a molti la lettura di un articolo pubblicato oggi sul «Corriere della Sera», che spiega come quella che è una specie di Cassa depositi e prestiti tedesca non fa calcolare il suo debito con le modalità previste dal Trattato di Maastricht. Se le regole di Maastricht fossero applicate in Germania a quella struttura, il debito pubblico tedesco salirebbe dall'80 al 98 per cento del PIL. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Quindi, in Europa le cose vanno forse diversamente da come alcuni Noi, per la nostra Cassa depositi e prestiti, quei debiti li calcoliamo e, se potessimo fare come i tedeschi, 100 miliardi di euro dal debito sparirebbero. Vorrei dire che i Governi consociativi farebbero crescere quel debito perché, nella mancanza di assunzioni di responsabilità, tutti scaricherebbero le richieste di ogni parte e, in Italia, proprio i Governi consociativi hanno fatto crescere notevolmente il nostro debito. A conferma di quanto la crisi sia planetaria e paradossale, mi ha molto colpito l'11 agosto leggere che la Banca centrale cinese in un comunicato ha detto che la Cina è disposta ad

La Cina ci chiede riforme liberali! Evidenzio il paradosso di questa crisi che attraversa il mondo; chi nega la democrazia al proprio interno - che è certamente molto ricco perché sfrutta il prossimo, non ha regole sociali ed inquina l'ambiente - ci esorta alle riforme. Noi le stiamo facendo e le faremo, ma anche a Pechino consigliamo una riforma: si chiama democrazia. La facciano anche loro in casa loro. I saldi di questa manovra sono stati rafforzati anche nelle ultime ore e consideriamo positivi i giudizi e le valutazioni di tanti organismi europei ed internazionali e abbiamo considerato con grande rispetto le valutazioni del Presidente della Repubblica. Voglio ricordare all'opposizione che il segretario del Partito Democratico l'11 luglio disse che bisognava accantonare quel primo decreto del Governo, trasformarlo in un disegno di legge e il Partito Democratico s'impegnava a garantirne l'approvazione entro la fine di settembre. Se avessimo seguito l'agenda di Bersani, oggi l'Italia sarebbe al collasso. Questa è la verità dei fatti. Abbiamo varato un decreto per il pareggio del bilancio nel 2014 seguendo le indicazioni europee e, nel mezzo di una grave crisi mondiale, l'Europa ha cambiato le sue valutazioni e noi a metà agosto, con rapidità, abbiamo condiviso le nuove valutazioni europee. È cambiata l'agenda

Il partito dei no blocca l'Italia e questa manovra serve anche a far ripartire il motore della crescita e dello sviluppo *(Applausi dai

consentitemi di ringraziare i senatori della maggioranza per la loro disponibilità, il loro spirito di sacrificio e la responsabilità nel condividere ogni scelta. *(Applausi dal Gruppo* è stata prudentemente valutata dal Governo zero; voi del Partito Democratico dite che vale 10 miliardi di euro di minori spese. Se sarà così i saldi della manovra saranno ancora più forti. Abbiamo accolto la vostra proposta di riaprire i termini di condono del 2002. Noi l'abbiamo valutata prudentemente zero, voi dite che porterà quattro miliardi di euro. Vuol dire che i saldi della manovra saranno ancora più forti. Abbiamo rivisto le decisioni sulle festività, sui Comuni, sulla tassazione delle rendite finanziarie. Il decreto-legge ha introdotto misure importanti

che anche noi avremmo voluto si evitasse, è dovuta alle scadenze internazionali, all'urgenza di assumere ulteriori misure e agli altissimi richiami che sono arrivati al Parlamento, che hanno portato il Governo a decidere che oggi il Senato approvasse in prima lettura queste misure per difendere i conti la credibilità dell'Italia sui mercati internazionali. Abbiamo deciso di modificare tante decisioni perché ci siamo confrontati con tutti. Se la manovra avrà saldi ancora migliori di quelli che sono stati indicati noi ci auguriamo - lo dico al Governo - che il capitolo della crescita possa trovare in futuro ulteriori risorse. però vogliamo rinforzare i saldi per affrontare in maniera forte e credibile i mercati internazionali, ma vogliamo anche che poi con i proventi della lotta all'evasione, affrontata con un coraggio che non ha precedenti, attraverso le misure per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, l'impegno che dovrà perseguire nella riforma della previdenza, si possano portare ulteriori risorse per la crescita e l'occupazione. Sul versante dei costi della politica domani il Consiglio dei ministri varerà ulteriori norme costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari, per l'abolizione di tutte le Province (ricordo, peraltro, che proposte di questa natura sono già in discussione al Parlamento). Sono state poi ridotte di migliaia di unità le cariche degli eletti. Noi vogliamo dare l'esempio, ma non vogliamo la morte della politica e della democrazia per lasciare il posto a governi eterodiretti da qualche banchiere che ha messo a repentaglio i soldi dei propri risparmiatori *(Applausi in Parlamento la democrazia e daremo l'esempio nel combattere i costi della politica. Credo che abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte anche con riferimento all'articolo 8 perché la politica di questo Governo è stata per la coesione sociale, per introdurre nelle fabbriche il dialogo tra le forze responsabili. Se

sono un'ulteriore dimostrazione di senso di responsabilità per il futuro dell'Italia, il futuro che questo Governo, questa maggioranza garantiranno per affrontare una crisi epocale dalla quale usciremo a testa alta.

quale ci viene presentato dalla Commissione competente comprensivo degli emendamenti presentati dal Governo, ne aumenta in qualche modo, rispetto a precedenti formulazioni, la credibilità e l'efficacia. Ciò è stato riconosciuto oggi dalle competenti istanze europee. Avrei perciò desiderato esprimere un voto favorevole, nello spirito delle preoccupazioni e sollecitazioni espresse dal Capo dello Stato e dalle stesse istituzioni europee, pur non nascondendomi la fragilità di alcune norme, l'ineguale distribuzione degli oneri, l'assenza di una visione complessiva proiettata anche verso la crescita economica e perciò verso un'effettiva graduale riduzione del debito. Ma il Governo ha deciso di giungere all'approvazione del testo apponendovi il voto di fiducia ed io non ritengo di poter votare la fiducia. Consapevole delle diversità di posizioni nell'ambito del Governo stesso, che trasudano dalla stessa elaborazione e scelta degli emendamenti e della complessiva situazione politica, la convinzione che qui desidero esprimere è che l'attuale composizione del Governo debba lasciare il posto ad una coesione più ampia, ad una attenuazione delle profonde contrapposizioni che emergono nel Paese, ad una posizione di politica interna ed estera che ridia all'Italia una presenza più credibile ed efficace nella politica europea ed internazionale. Per queste ragioni, esprimerò il mio dissenso attraverso il voto di astensione, non partecipando al voto stesso. 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, con le precisazioni al testo illustrate dal rappresentante del Governo e con la conseguente modifica del titolo del disegno di legge di conversione, inerente l'introduzione di una delega legislativa.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 Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Onorevoli colleghi, alla Presidenza sono

Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio,

D'Ambrosio

Matteoli, Mauro, Mazzaracchio,

Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli,

La violenza è sempre un gesto contro la democrazia. Protestare è garantito dalla Costituzione, così come lo sciopero e tutte le forme pacifiche Quando si manifesta però in forma violenta davanti ai Palazzi delle istituzioni ma contro lo convivenza civile, e in ogni momento, ciò rappresenta naturalmente un *vulnus* per la nostra democrazia e per il nostro Paese. Voglio ringraziare nel contempo le forze dell'ordine che, da quanto ho appreso, si stanno impegnando, rischiando anche la loro incolumità, per evitare che queste manifestazioni possano arrivare nelle immediate prossimità del Senato.